L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

che è previsto dalla riforma della *governance* economica europea quale strumento per la definizione del quadro programmatico di finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale. Il quadro di riferimento esposto dal Piano include un orizzonte temporale che si estende dal 2025 al 2029. La disciplina transitoria stabilita dalla nuova normativa europea prevede la presentazione alle istituzioni europee del primo Piano entro il 20 settembre 2024, salvo proroghe concordate con la Commissione. Il Governo italiano ha comunicato alla Commissione l'intenzione di posticipare la trasmissione del Piano al fine di poter disporre della revisione dei dati di contabilità nazionale pubblicati dall'Istat lo scorso 23 settembre. L'invio del Piano alle istituzioni europee dovrebbe avvenire entro la metà di ottobre, in concomitanza con la trasmissione del Documento programmatico di bilancio. Sulla base delle condizioni previste dalla normativa europea e dello scambio tecnico avvenuto con il Governo, il 21 giugno scorso la Commissione ha trasmesso all'Italia la traiettoria di riferimento della spesa netta. Nel mese successivo si è svolto un dialogo tecnico tra il Governo e la Commissione europea, per discutere i principali contenuti del Piano, tra cui il sentiero di spesa netta, le prospettive economiche e fiscali e il programma di riforme e di investimenti. Il 26 luglio il Consiglio dell'Unione europea ha avviato una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia e di altri sei Stati membri. A settembre, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze i propri rilievi relativi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio del Piano strutturale di bilancio 2025-2029 e, in data 25 settembre 2024, sempre l'UPB ha inviato una lettera di conferma della validazione del quadro macroeconomico tendenziale aggiornato alla luce delle stime diffuse dall'Istat, relative alle revisioni generali dei conti economici nazionali. Il 25 settembre il Governo ha presentato alle parti sociali lo schema di Piano strutturale di bilancio. La proposta di Piano è stata quindi deliberata dal Consiglio dei ministri e trasmessa al Parlamento il 27 settembre. Dopo l'esame di oggi, il Governo dovrà inviare il piano alle istituzioni europee. La Commissione europea valuterà la proposta entro sei settimane e il Piano dovrà infine essere approvato con raccomandazione dal Consiglio dell'Unione europea. Secondo le disposizioni transitorie, durante il periodo in cui è in vigore il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli interventi del PNRR possono essere presi in considerazione per l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro Inoltre, tale disciplina transitoria prevede che i progetti di spesa finanziati con i prestiti del PNRR, o con forme di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea negli anni 2025 e 2026, possano valere per modulare in modo più graduale la correzione di bilancio richiesta durante il percorso di aggiustamento. Nonostante il Piano rappresenti un documento di programmazione valido fino al 2029, il Governo italiano intende richiedere l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio a sette anni. Di conseguenza, il Piano espone la programmazione delle correzioni di bilancio richieste dalla nuova *governance* economica, in un orizzonte temporale che arriva al 2031 Il Piano strutturale di bilancio ha le finalità di: porre le basi di una programmazione pluriennale della politica di bilancio tendente alla sostenibilità delle finanze pubbliche e all'aumento della crescita potenziale supportata da riforme ed investimenti; affrontare le criticità strutturali del sistema economico e sociale dell'Italia, tra cui quelle riportate nelle raccomandazioni specifiche per Paese; per ultimo, contribuire al raggiungimento degli obiettivi connessi alle priorità comuni dell'Unione europea. Il livello dell'andamento della spesa netta prevista dal Governo tiene conto della necessità di ricondurre il rapporto tra indebitamento netto e PIL al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2026, in linea con le previsioni della NADEF 2023 e del Documento programmatico di bilancio del 2024. Si propone altresì di rispettare i criteri dell'analisi di sostenibilità del debito e le condizioni previste dalla normativa europea vigente. Il tasso di crescita della spesa netta indicata dal Governo risulta in linea con la correzione strutturale minima richiesta dalla procedura per disavanzi eccessivi.

della correzione di bilancio nei primi due anni, con l'obiettivo di correzione annuale del saldo primario strutturale, pari a circa lo 0,55 per cento del PIL nel 2025 e nel 2026, e obiettivi per una correzione lineare, pari a circa lo 0,52 per cento del PIL per gli anni dal 2027 al 2031. Secondo quanto esposto nel Piano elaborato dal Governo, i citati obiettivi di correzione annuale del saldo primario strutturale corrispondono al tasso medio di crescita annuale della spesa netta espressa a prezzi correnti, pari all'1,5 per cento fino al 2031, che la Commissione europea ha formulato nella traiettoria di riferimento trasmessa lo scorso giugno. In questo nuovo quadro europeo di *governance* economica, la sostenibilità del debito nel lungo periodo è assicurata tramite il raggiungimento di un obiettivo di miglioramento del saldo primario strutturale nel medio termine. Il raggiungimento dell'obiettivo del saldo primario strutturale è a sua volta assicurato dal rispetto di un profilo di crescita della spesa netta, che deve anche attenersi all'ulteriore indice di salvaguardia introdotto nel Patto di stabilità e crescita. Per quanto riguarda l'Italia, per la definizione del profilo di spesa rileva, oltre all'obiettivo del saldo primario strutturale, un indice di riferimento minimo che prevede per gli Stati membri che - come l'Italia - dal 2024 si trovano nella procedura per disavanzi eccessivi, un percorso di correzione di bilancio tale da assicurare un miglioramento minimo del saldo strutturale complessivo di almeno 0,5 punti percentuali di PIL all'anno. Le nuove regole prevedono una eccezione per gli anni 2025-2027 in relazione ai quali l'indice è applicato con riferimento non già al saldo strutturale complessivo, ma al saldo primario strutturale per tener conto dell'aumento atteso del rapporto tra spesa per interessi e PIL rispetto agli anni precedenti. Il profilo di spesa identifica i tetti massimi di crescita annuali della spesa netta che gli Stati membri si impegnano a non superare. Nel dettaglio l'aggregato della spesa netta sottoposto a sorveglianza fiscale è definito come spesa finale delle amministrazioni pubbliche al netto delle seguenti voci: spesa per interessi; spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziati da trasferimenti provenienti dall'Unione europea; spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; componente ciclica della spesa per disoccupazione; misure discrezionali dal lato delle entrate; misure *una tantum* e altre misure temporanee di bilancio. Il Governo adotta una metodologia differente da quella della Commissione europea per stimare l'andamento dei principali indicatori di bilancio. Nel Piano si fa presente come, introducendo il citato tasso medio di crescita annuale della spesa netta, il *deficit* possa migliorare più rapidamente di quanto previsto dalle stime della Commissione europea, pur considerando la previsione di crescita prudenziale. Ciò deriverebbe dal fatto che l'analisi della sostenibilità del debito della Commissione si fonda su una metodologia che considera parimenti comuni per tutti gli Stati membri e dati di partenza differenti rispetto a quelli usati dal Governo, per quanto riguarda sia il profilo annuale dell'aggiustamento, sia il valore dei dati di finanza pubblica considerati. Le metodologie impiegate dal Governo consentirebbero altresì un più elevato grado di titolarità nazionale delle scelte di programmazione economica. Infine, il Piano espone anche le variabili irrilevanti per la sostenibilità delle finanze pubbliche, i saldi di bilancio nominali e strutturali, gli investimenti pubblici con particolare enfasi sulla componente finanziata da risorse nazionali, gli interessi passivi e il rapporto debito PIL. Nel Piano strutturale di bilancio è espresso l'impegno a completare l'attuazione del PNRR e a estendere la portata negli anni futuri. Negli anni 2025-2026 l'Italia concentrerà i propri sforzi per conseguire la piena attuazione del Piano mentre negli anni successivi l'azione riformatrice sarà dedicata a consolidare e a sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti. Dopo il 2026 il Piano prevede ulteriori interventi strutturali volti a migliorare la qualità delle istituzioni e quella dell'ambiente imprenditoriale, con interventi in cinque ambiti: giustizia, amministrazione fiscale, gestione responsabile della spesa pubblica, supporto alle imprese e promozione della concorrenza pubblica amministrazione. La previsione di queste ultime misure tiene in considerazione anche gli altri programmi di intervento già avviati dall'Italia e finalizzati all'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio a sette anni. Il Piano descrive anche altre politiche di carattere settoriale per il perseguimento delle priorità strategiche nazionali ed europee che necessiteranno di forme di coordinamento con gli altri Stati membri dell'Unione europea: la resilienza sociale ed economica, l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, la transizione verde e quella digitale, lo sviluppo delle filiere produttive compatibili con il contrasto ai cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e il contrasto al degrado e all'illegalità. Il Piano include anche delle misure per il rafforzamento della capacità di difesa. Gli interventi delineati nel Piano offrono altresì una risposta ai rilievi emersi nell'ambito delle raccomandazioni specifiche del Consiglio dell'Unione europea indirizzate all'Italia dal 2019 ad oggi. Infine, il Piano nel suo insieme mira a sviluppare ulteriormente quanto intrapreso con il PNRR, in particolare con riguardo agli investimenti per migliorare le prospettive demografiche, l'istruzione e la ricerca, nonché l'allineamento delle competenze dei lavoratori a quelle richieste dal mercato del lavoro, oltre ad assicurare maggiori servizi di cura per la prima infanzia, il potenziamento delle politiche attive per il mercato del lavoro e la coesione economica e sociale, nonché ad accelerare le transizioni verde e digitale. Il Piano strutturale di bilancio espone anche la stima dell'impatto sul PIL reale delle riforme e degli investimenti del PNRR fino all'anno 2031, suddividendo tale impatto tra le riforme implementate e da implementare e tra gli investimenti implementati e da implementare. Sono inoltre analizzati gli impatti sul PIL delle nuove riforme valide per l'estensione del Piano strutturale di bilancio. La riforma prevista dal Piano relativa all'amministrazione fiscale è valutata nell'ambito del quadro macroeconomico programmatico del disegno di legge di bilancio 2025. Tuttavia, nel Piano si afferma che le misure in materia fiscale potrebbero avere un impatto positivo anche nel lungo periodo. Nel Piano si afferma pertanto che l'insieme delle riforme PNRR implementate produrrebbe un incremento del livello del PIL del 2,2 per cento al 2031; il completamento delle riforme da implementare produrrebbe al 2031 un ulteriore aumento di 1,7 punti percentuali; l'insieme degli investimenti PNRR implementati porterebbe ad un aumento del livello del PIL dello 0,7 per cento nel 2031, a cui si sommerebbe un ulteriore effetto positivo pari a 1,5 punti percentuali, realizzando anche gli ulteriori investimenti da implementare dopo il 2024. Per quanto riguarda le nuove misure valide per l'estensione del Piano, queste produrrebbe un aumento del livello del PIL al 2031 dello 0,5 per cento. Nel complesso, le misure valide per l'estensione del Piano, ovvero gli investimenti e le riforme da implementare del PNRR e le nuove riforme, potrebbero condurre ad un aumento del PIL del 3,8 per cento entro il 2031. Dopo l'approvazione con raccomandazione da parte del Consiglio dell'Unione europea del livello di variazione della spesa netta, il Piano sarà realizzato secondo le misure previste annualmente dalla legge di bilancio e dalle altre politiche pubbliche. Il monitoraggio è demandato alla relazione annuale sui progressi compiuti da trasmettere alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno. Dopo aver evidenziato la coerenza del percorso programmatico con il perseguimento di un obiettivo di saldo primario strutturale, sostanzialmente in linea con quello scaturito dalle condotte della Commissione, il Piano dimostra la conformità del medesimo percorso anche ai vincoli imposti sia dalla procedura sui disavanzi eccessivi, sia dalle clausole di salvaguardia quantitative individuate nel quadro della nuova *governance* economica europea. Queste ultime indicano una dimensione minima dell'aggiustamento fiscale annuo richiesto agli Stati membri, con riguardo al debito e al saldo complessivo di bilancio. Infine, la normativa europea prevede la clausola volta a evitare che la maggior parte dello sforzo di correzione del saldo primario strutturale sia differita agli anni finali del periodo di aggiustamento. In particolare per quanto attiene alla procedura dei disavanzi eccessivi, si ricorda che nel giugno scorso la Commissione ha pubblicato un rapporto, ai sensi dell'articolo 126, con il quale ha proposto l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo per sette Paesi, tra cui l'Italia, il cui *deficit* risultava superiore alla soglia del 3 per cento in ragione del PIL in tutti gli anni dell'orizzonte di previsione. La normativa in vigore non modificata sul punto rispetto alla precedente versione del Patto di stabilità e crescita, prevede che i Paesi soggetti a procedura sui disavanzi eccessivi operino una correzione annua del saldo di bilancio non inferiore a 0,5 punti percentuali del PIL in termini strutturali. Nel quadro programmatico delineato dal Piano, il *deficit* ritorna su valori inferiori al 3 per cento già dal 2026; la correzione annua del saldo primario strutturale risulta pari a 0,55 punti percentuali del PIL nel 2025-2026, mentre dal 2027 al 2031 assume carattere lineare, attestandosi sullo 0,52 per cento del PIL all'anno. Risulta quindi implicitamente soddisfatta la correzione richiesta dalla procedura

per verificare il rispetto della clausola occorre calcolare il valore medio della riduzione del rapporto debito-PIL, prevista per gli esercizi 2027-2029 compresi nel Piano.

restanti anni del periodo di aggiustamento, la riduzione ricavabile dalla tavola 2.1.4 del Piano si attesta sull'1 per cento nel 2030 e sull'1,4 nel 2031. Il Governo sostiene che l'avanzo primario strutturale conseguito alla fine del periodo settennale di aggiustamento, pari al 3,2 per cento del PIL, sarà sufficiente a garantire che, nei dieci anni successivi alla fine di tale periodo e in assenza di ulteriori misure di correzione fiscali, il rapporto debito-PIL sia posto su una traiettoria plausibilmente discendente. L'indebitamento netto continua a essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL. Sebbene la Commissione europea abbia richiesto esplicitamente di non considerare gli effetti sulle previsioni di crescita programmatica all'interno del piano delle riforme e degli investimenti non ancora attuati, nel Piano strutturale di bilancio il Governo mostra che l'impatto delle riforme del PNRR da attuare e delle riforme aggiuntive oggetto dell'estensione del periodo di aggiustamento del Piano strutturale di bilancio porterebbe il rapporto debito-PIL a ridursi fino al 102,5 per cento Anche con il metodo di analisi stocastico, l'ipotesi di riduzione del debito pubblico appare plausibile. In dettaglio, la probabilità che il rapporto debito-PIL si collochi nel 2036 un livello inferiore a quello del 2031 è pari al 74,5 per cento: quindi una probabilità superiore alla soglia minima del 70 per cento. L'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'audizione del 7 ottobre 2024, ha proceduto a validare le previsioni macroeconomiche programmatiche, dopo aver validato il quadro macroeconomico tendenziale sull'orizzonte temporale del Piano strutturale di bilancio. Infine, come ho detto in apertura, la Commissione programmazione economica, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento in discussione.

Ma, al di là di questo, segna un passo in avanti - secondo me - nella comprensione da parte della cultura politica e dell'opinione pubblica del valore non totemico ma sostanziale di una certa disciplina di bilancio e, infine, rappresenta la cartina di tornasole rispetto alla credibilità o mancanza di credibilità di diversi altri protagonisti della politica. Io vorrei dare atto al presidente Meloni e al ministro Giorgetti di avere tenuto la barra dritta, certamente aiutati da quei pur tanto deprecati vincoli europei, ma anche per l'emergere di una convinzione nuova in uno di loro due, non nuova nell'altro. Mi riferisco al fatto che il ministro Giorgetti, da molto tempo, pur appartenendo a un partito non sempre sulla stessa lunghezza d'onda con lui su queste tematiche, spesso su una lunghezza d'onda opposta, ha dato prova di capire il significato del bilancio pubblico e della sua disciplina. Ricordo spesso - l'ho fatto anche in quest'Aula il suo contributo, come Presidente della Commissione bilancio della Camera nel 2012, essendo il suo partito all'opposizione, all'approvazione della modifica costituzionale in ordine alla disciplina di bilancio. Ma molto più nuova e da salutare con sincerità è la ferma presa di posizione del Presidente del Consiglio che, nelle sue dichiarazioni in tutti questi mesi, ha detto cose di eminente buonsenso, tuttavia antitetiche a quelle che ella stessa usava dire - come molti esponenti delle opposizioni - nel corso degli anni precedenti. Queste modifiche di indirizzo io credo siano importanti da segnalare non per divertimento circa l'andamento grafico delle posizioni di una personalità nel tempo, ma perché danno il senso, nella cultura politica complessiva di un Paese anche di un Paese che non ha, nella sua tradizione, la comprensione che i soldi dello Stato sono i nostri soldi e i debiti dello Stato sono i nostri debiti - evoluzione è senz'altro positiva. Certo, nella sostanza è anche importante che questa presa d'atto di un miglioramento di fondo non offuschi quelle cautele, quelle preoccupazioni espresse in particolare dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio parlamentare di bilancio. In particolare, credo che occorreranno sforzi molto maggiori, per quanto riguarda il versante della spesa pubblica, in termini di revisione e in termini di contenimento. Personalmente, mantengo un dissenso piuttosto profondo sulla visione della distribuzione del prelievo fiscale che ha questo Governo. Per queste ragioni, mi riservo di leggere le mozioni, ma non credo che voterò a favore. Però, è importante - secondo me - molto più del mio singolo voto, che si constati questa evoluzione indubbiamente positiva. Infine, vale la pena che queste occasioni di verifica di avanzamento e di verifica di tappe nella storia politico economica di un Paese siano anche accompagnate da una valutazione delle conseguenze che tutto ciò potrà avere sulla stabilità e incidenza del Governo. Credo che come cartina di tornasole l'adesione della maggioranza alla linea Meloni e Giorgetti metta in luce in modo molto, ma molto evidente l'incoerenza in particolare di una personalità che ha perseguitato il dibattito politico italiano degli ultimi dodici anni, togliendo ad esso serietà inserendovi insulti e calunnie quando non, di fatto, incitazioni a compiere atti lesivi della libertà individuale. Mi riferisco al vice presidente del Consiglio Salvini. preoccupato se in lui prevalesse - come è ben possibile - il senso di una profonda dignità e di rispetto della coerenza, perché questo non potrebbe che condurlo alle dimissioni. Il presidente Salvini ha superficialmente, ma con consenso di pubblico e, a suo tempo, di applausi in molti luoghi da lui frequentati, demonizzato in particolare gli interventi che, in un momento drammatico per il nostro Paese,

che oggi non può dire di essersi preso a carico una parte di impopolarità per evitare il dissesto del bilancio dello Stato; tutti gli altri sì. Ha demonizzato tutto ciò che è stato fatto sulle pensioni e si è particolarmente accanito contro la seconda firmataria di quel provvedimento, il ministro Fornero, e il primo ero naturalmente io.

del sistema pensionistico e vi si leggono le premesse di ulteriori irrobustimenti necessari a tal fine. Il presidente Salvini, che per tanti altri aspetti trovo non solo di grande valore come uomo politico, ma anche figura interessante e simpatica, ha giurato - per quello che possono valere i giuramenti, in generale, e i suoi in particolare - di eliminare quella legge innominabile - lo seguo - non appena si sarebbe trovato in posizione di Governo. Si è trovato varie volte in posizioni di Governo e questa volta credo che finirà, con un decoroso silenzio, per accettare la posizione del Governo sulle pensioni. Presidente Salvini, non faccia prevalere la dignità. Capisco il suo intimo impulso a dimettersi in questo momento, ma non credo che, ora, questo farebbe il bene dell'Italia,

il Governo che deve stare lì a governare l'Italia. Speriamo quindi che il presidente Salvini sopporti, per il bene del Paese, qualche altro momento di intollerabile contraddizione intima, senza far prevalere il senso della dignità.

con il Piano strutturale di bilancio che arriva oggi in Senato si compie un'ulteriore tappa di avvicinamento molto importante alla manovra di bilancio dopo l'approvazione del Documento di economia e finanza. Mi verrebbe da definirla una *via crucis*, anche per i provvedimenti che sono stati approvati dal Governo. Con il Documento di economia e finanza è stato il tempo dei grandi annunci, coperti dal fatto che nel testo il Governo non aveva indicato alcun piano di programmazione, né in entrata, né in uscita. Con questo Piano strutturale si iniziano a vedere almeno i dati macroeconomici e le spese che si intendono fare - e non sono buone notizie per le cittadine e i cittadini italiani ma ancora mancano le strategie e il quadro programmatico, così com'erano mancati nel Documento di economia e finanza. Governare un Paese significa guardare alla costruzione di un futuro di crescita, occupazione e benessere. Questo Governo, invece, ha costruito un documento senza alcuna visione, il cui orizzonte è quello di questa legislatura: un piano economico che serve a salvare il presente per cacciare in avanti le responsabilità di far fronte alla crisi che vive il nostro Paese e, soprattutto, per rimandare alla prossima legislatura e al prossimo Governo l'onere di pagare tutto il debito. Non c'è traccia di un piano industriale, indispensabile per tornare a crescere. Le politiche industriali del Governo Meloni si riducono alla svendita degli *asset* nazionali e di qualche partecipazione; nessuna politica occupazionale e nessuna strategia per la pubblica amministrazione; politiche che vengono ampiamente citate, ma se andiamo a guardare gli interventi concreti, tutto è posticipato al 2027, che, se non sbaglio, a lume di naso, mi pare l'anno in cui si andrà a votare. Ancora, manca un serio piano delle riforme. Poggiate tutto sull'attuazione del Piano Come non ricordare, anche in quest'Aula, l'opposizione che Fratelli d'Italia fece a questo Piano nella scorsa legislatura? E non viene fatto alcun accenno alle riforme che serviranno al Paese per il futuro. Vi perdete per strada la transizione ecologica e digitale, così come la sfida per modernizzare il Paese. Le criticità di questo Piano strutturale di bilancio sono molte e sono emerse con forza durante le audizioni, sottolineate da enti che peraltro non hanno come compito quello di condurre l'opposizione a questo Governo, ma che sono chiamati ad ammonire rispetto alla strada che si intraprende. Ieri Bankitalia ha prima fatto luce sullo scenario programmatico, evidenziando che le previsioni del Governo sul PIL non coincidono con quelle di via Nazionale. Lo stesso è stato fatto notare dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Non si arriverà alla crescita dell'1 per cento del PIL nel 2024: lo hanno detto a chiare note e alla fine, anche ieri sera, il ministro Giorgetti lo ha confermato. L'audizione di Bankitalia ha soprattutto aperto gli occhi sul rischio reale in assenza di politiche per aumentare le entrate; ne cito una a caso: rafforzare la lotta all'evasione fiscale. Lo stesso taglio del cuneo fiscale può mettere a rischio il sistema previdenziale. Lo diceva poco fa il presidente Monti. Voi provate a nasconderlo, ma finanziate i vostri interventi - parlo del taglio del cuneo fiscale - con i soldi dei dipendenti e dei pensionati e intanto continuate ad aumentare il perimetro della *flat tax* e delle rottamazioni fiscali per chi evade le tasse. Vengo al cuore della questione che mi preme di più, a quel tema su cui questo Governo si è dimostrato essere campione di annunci e scarso nel raggiungere i risultati: la sanità. È su questo terreno che vengono a galla le contraddizioni della vostra azione di Governo: la spesa per la salute delle famiglie italiane, come ci ha ricordato, con dati precisi, proprio ieri la Fondazione GIMBE, è cresciuta del 10,3 per cento solo nel 2023 e sono più di 4,5 milioni le persone che hanno smesso di curarsi. Sono numeri preoccupanti che, uniti alle diseguaglianze regionali, alla migrazione sanitaria, alle liste d'attesa e alla carenza del personale sanitario, fotografano quella quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria emergenza per il Paese. Un quadro drammatico, che diventa ancor più critico se pensiamo che, in un'Italia ridotta in queste condizioni, voi volete attuare la legge sull'autonomia differenziata e divaricare così le diseguaglianze Sapete cosa significa questo? Che state facendo scivolare, piano, piano, senza dirlo, il nostro sistema sanitario nazionale verso il privato. Inizio a temere che, in fondo, una strategia ci sia e sia proprio questa: ridurre la presenza dello Stato, indebolire i servizi sanitari pubblici per favorire la sanità privata.

dell'orientamento di questo Governo. Questo è un punto decisivo e in questi mesi il Partito Democratico non si è limitato a criticare le scelte del Governo, ma ha cercato anche di proporre soluzioni per rafforzare la sanità pubblica, perché per noi questa è la condizione indispensabile per garantire a tutte e a tutti il diritto alle cure e l'unica strada possibile per non lasciare indietro i più fragili. Lo abbiamo fatto con la proposta di legge a prima firma Schlein per finanziare in tre anni il sistema sanitario nazionale e portarlo sulla media dei Paesi europei; e non ci siamo fermati. Solo ieri abbiamo proposto di invertire la rotta rispetto a una linea programmatica, quella che indicate voi con questo Piano strutturale, che rischia di portare al *default* la sanità pubblica: vi abbiamo chiesto - e lo proporremo anche nel disegno di legge di bilancio del primo anno di questo Piano - di destinare le entrate che avete previsto per la riduzione delle aliquote Irpef (4,3 miliardi di euro) alla sanità. Sarebbe il segnale concreto di un Paese che si assume la responsabilità di onorare l'articolo 32 della nostra Costituzione.

Sulla spesa sanitaria c'è anche un altro capitolo che rimane ancora senza risposta ed è quello dei fondi integrativi. Avete voluto un'indagine conoscitiva proprio in Senato, ma non si vedono risposte. Siamo preoccupati perché temiamo che, anche su questo terreno, alla fine prevarrà la logica privatistica. È per questo motivo - e mi accingo a concludere, Presidente - che oggi, in quest'Aula, non ci soffermiamo solo sul Piano strutturale di bilancio di medio termine in discussione, ma mettiamo le mani avanti, avanzando le nostre preoccupazioni in vista della manovra. Solo ad inizio estate erano state annunciate risorse per la sanità, ma con questo Piano strutturale di bilancio scopriamo che non c'è niente. Come possiamo essere ottimisti per la legge di bilancio? Siamo preoccupati perché, a giudicare dai dati e dalle previsioni che ci sono state presentate, scopriamo che le vostre politiche economiche colpiscono le fasce più fragili della nostra società. State costruendo un Paese nel quale chi è più forte ce la fa e chi è più debole rimane indietro, portandosi anche la colpa della propria condizione: essere poveri per questo Governo è una colpa. Ma un Paese senza crescita, senza occupazione di qualità e senza giustizia sociale è un Paese senza futuro. Se ne stanno accorgendo tutti.

il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, di cui oggi discutiamo, altro non è che quella che una volta chiamavamo NADEF, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, cioè quel documento che il Governo presentava in questo periodo dell'anno, tra settembre e ottobre, per indicare quali erano gli obiettivi del disegno di bilancio che avrebbe poi presentato di lì a pochi mesi. Come sappiamo,

In sostanza cioè per i prossimi anni queste saranno le linee di azione del Governo, quindi anche dello Stato italiano una volta approvato dal Parlamento, dalle quali non sarà consentito discostarsi,

che sarebbero ancora più difficili e imprevedibili rispetto alle stesse linee dettate dal Governo. Questa premessa, che potrebbe sembrare semplicemente didascalica, mi serve semplicemente per dire

che cosa intende intraprendere con i fondi del PNRR, con gli investimenti; quali azioni di intervento intende intraprendere nella sanità pubblica. Dove vogliamo andare con questa sanità? Sono due anni che continuiamo a tergiversare, senza varare misure che effettivamente intervengano per sanare il problema, per dare fondi ai cittadini per curarsi.

spesa quasi incontrollata, siamo stati chiamati a rendere conto, come degli studenti che un po' hanno dilapidato il patrimonio che gli era stato dato dai genitori: ne siamo consapevoli e tutti siamo responsabili. però gli strumenti adottati per ridurre il *deficit* e per uscire fuori da questa fase di *impasse* e di fermo della crescita che non ci convincono. Né in questo documento troviamo qualcosa che ci dica che il Governo ha capito che deve fare uno sforzo in avanti; che ci faccia intendere che finalmente ha trovato gli strumenti per una programmazione economica e che finalmente si è reso conto che è necessario un piano di rilancio industriale.

lo ammette: le cifre sono quelle che in questi documenti rendono evidente il discorso che le lettere magari possono lasciare ad interpretazioni fuorvianti; i numeri ci richiamano alla realtà. Quando lo stesso Governo disegna e ammette che c'è una curva discendente del PIL programmatico, che passa dall'ottimistico 1,2 per cento del 2025 allo 0,6 del 2029, questo altro non è che l'ammissione che le scelte economiche compiute dal Governo, nella previsione peraltro che lo stesso Governo fa di se stesso fino al 2029, sono al

ad arginare quella che è chiaramente, a questo punto, una tensione anche emotiva di fronte a un documento del genere, semplicemente basandoci su dichiarazioni programmatiche che poi, alla fine, vengono smentite dagli stessi numeri forniti dal Governo?

assumere in maniera leggera. E non se la possono assumere ancor di più perché, come sempre, anche questo documento interviene senza una previa, giusta e articolata consultazione con le parti sociali, ma solo e sempre con imposizioni fondate sui numeri della maggioranza. Signora Presidente, mi avvio alla conclusione, ma vorrei dire soltanto una cosa a proposito delle stime sulle pensioni e sulla riforma delle pensioni. Il presidente Monti è stato chiarissimo sul tema, ma c'è un dato che sconfessa le ambizioni della maggioranza, che, quando sedeva sugli scranni barricadieri dell'opposizione, la faceva

l'autorevole Istat, che richiama il Governo a un bagno di confronto con la realtà e forse anche a un bagno di umiltà, sulla base della previsione di crescita e di invecchiamento della popolazione italiana

signori del Governo, colleghi senatori, oggi discutiamo del Piano strutturale di bilancio di medio termine, un documento importante che, come sapete, ha due obiettivi generali: riportare

il Governo rientra nei ranghi della disciplina di bilancio europea. Rientra nei ranghi perché per anni l'attuale maggioranza ha criticato la stupidità del vecchio Patto di stabilità, contestando anche il nuovo, astenendosi nella votazione definitiva al Parlamento europeo e ravvisandovi le tracce della tanto odiata austerità Una posizione apparentemente simile a quella di Azione, che però aveva dichiarato ai tempi la propria al nuovo Patto per ragioni diametralmente opposte, come ricordai proprio nell'Aula del Senato il 24 aprile 2024, durante la discussione del DEF, sostenendo - cito testualmente che il nuovo Patto di stabilità è inadeguato rispetto a quella radicalità necessaria per aumentare la competitività, sostenere la spesa in materia di difesa comune e fare gli investimenti necessari per realizzare davvero la transizione ecologica e digitale. Mi perdonerete, so che è inelegante inelegante citarsi rispetto a un intervento. Lo faccio per una ragione molto semplice, vale a dire che quella previsione ha trovato conferma nel rapporto sulla competitività che il Presidente Draghi ha presentato alle Istituzioni europee nelle scorse settimane proponendo, lì sì, una vera e propria evoluzione economica istituzionale che va nella direzione opposta a quella che voi sostenete o che almeno una certa parte della maggioranza sostiene, cioè di una maggiore integrazione politica europea e del rafforzamento qualitativo e quantitativo del bilancio dell'Unione europea rispetto ai bilanci nazionali. E allora sì, questo documento vi fa rientrare nei ranghi della disciplina di bilancio europeo. Il problema è che voi non chiarite come lo farete e avete strutturato il vostro piano su delle previsioni di crescita e di maggiori entrate che, come minimo, si possono definire ottimistiche. Vi siete concentrati solo

è quantomeno "dopata" dal PNRR. Ieri è stato lo stesso ministro Giorgetti, al termine dell'esame del Piano in Commissione, ad ammettere che la stima di crescita per il 2024 è irrealistica. Ad oggi abbiamo speso 53,5 miliardi di euro su 194,4 miliardi totali del PNRR e nonostante questo, abbiamo un tasso di crescita basso. Ci rendiamo conto che questa stima di crescita non potrà far conto del fatto che i soldi del PNRR ci saranno sempre e che essi non vanno spesi, ma devono avere un effetto moltiplicatore sugli investimenti e sulla crescita che invece manca? È questo il vero fallimento del questo Governo sul tema. Noi abbiamo indicato le priorità sulla spesa sanitaria e sull'istruzione, e nella risoluzione che abbiamo depositato vi proponiamo una sfida riformatrice, volta ad inserire, a partire dalla legge di bilancio, il tema del nucleare di quarta generazione affinché alle parole seguano i fatti, altrimenti l'indipendenza energetica non sarà raggiungibile nel nostro Paese. Siete pronti a farlo o no? Questa è la sfida che vi chiediamo; non solo rientrare nei ranghi della disciplina di bilancio europea, ma indicarci in maniera seria e realistica come raggiungere questi obiettivi. Quello che questo documento purtroppo non contiene.

La CGIL ha detto che si tratta di austerità selettiva, scaricata su lavoratori e pensionati. La UIL dice che difficilmente il Piano porterà alla crescita di cui il Paese ha bisogno. La CISAL dice che è una cornice restrittiva. Confartigianato e Casartigiani hanno detto che è sbagliato tornare a politiche di *austerity*. Confesercenti ritiene che sia assente una spinta ai consumi. Confcommercio dice che i consumi delle famiglie languono. Potrei continuare all'infinito. Chiedo, se possibile, l'attenzione del Sottosegretario. Mi dispiace che non abbia ascoltato l'inizio di questo intervento *(Applausi)*, ma evidentemente è più comodo non ascoltare le audizioni, nemmeno quando esse vengono riprese in Aula. Il ministro Giorgetti ha detto chiaramente che la manovra di bilancio richiederà sacrifici. Le faccio allora un'altra domanda, caro Sottosegretario, sacrifici per chi? per chi? Non sembra che siete pronti a chiedere sacrifici alle banche, agli evasori fiscali, alle squadre di calcio a cui continuate a fare regali. I sacrifici, caro Sottosegretario, li state chiedendo ai pensionati a cui avete tagliato già nella scorsa legge di bilancio 60 miliardi di euro nei prossimi vent'anni; li state chiedendo ai malati, visto che siete siete tornati a tagliare risorse alla sanità, dove si investe meno di quello che si investiva prima della pandemia. Li chiedete poi all'industria, visto che non ci sono investimenti e la produzione industriale è infatti in calo da diciotto consecutivi. Li avete chiesti alla povera gente, a cui avete tolto anche il sussidio di sostegno alla povertà che li ha aiutati in questi anni. E allora, dobbiamo dirci chiaramente che siete tornati alla ricetta della vera e propria *austerity*, quindi l'avanzo primario, il precariato selvaggio, la privatizzazione degli *asset* strategici. Ma non era la stessa Presidente del Consiglio che, quando è entrata a Palazzo Chigi, in una delle prime interviste a «Il Sole 24 Ore», aveva detto che il debito si riduce con la crescita? Qui la crescita non c'è, caro Sottosegretario, perché Bankitalia e Ufficio parlamentare di bilancio hanno stimato la crescita al ribasso allo 0,8 per cento e di non ci avete detto quanto in realtà è legato al PNRR, perché l'Ufficio parlamentare di bilancio dice che il PNRR su questo 0,8 incide in una maniera significativa. Vede qual è la differenza tra noi e voi, Sottosegretario? Voi avete ereditato un Paese in crescita, un Paese con un PIL che era cresciuto in due anni di 20 punti, anzi è stato stimato al rialzo proprio in questi giorni; il rapporto debito-PIL era calato perché il Paese gli investimenti erano aumentati del 20 per cento nel 2021 e del 10 per cento nel 2022, i consumi delle famiglie erano in ripresa, così com'era in ripresa la produzione industriale e, soprattutto, c'era una rete sociale che proteggeva i più fragili, che è quello che si deve fare quando c'è una grande frammentazione sociale come quella che stiamo vivendo. Voi avete ereditato - e per fortuna, perché è l'unico strumento di crescita che c'è - il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il più grande piano di investimenti pubblici dal Dopoguerra ad oggi: 200 miliardi di euro che devono servire a modernizzare

totalmente sperperata, accettando, tra l'altro, un Patto di stabilità che ci costerà 13 miliardi di nuovi tagli e nuove tasse. Poiché è chiaro che non ci sono le coperture per la prossima manovra di bilancio e abbiamo capito che state cercando di capire dove tagliare per reperire risorse, vi faccio una proposta che in realtà è stata lanciata proprio qui in Senato la settimana scorsa dagli oncologi medici, dalla Fondazione Veronesi, dalla Fondazione AIRC, da tante fondazioni che si occupano di oncologia, partendo da una premessa: se non ve ne siete accorti, oggi siamo in una nuova pandemia, che si chiama pandemia oncologica, perché c'è un aumento della diagnosi dei tumori, soprattutto in fase avanzata, perché non sono stati fatti gli *screening*, perché oggi il tempo medio per una mammografia è di 700 giorni e fare una mammografia due anni dopo vuol dire scoprire un tumore che probabilmente non si può più curare, perché ci sono liste d'attesa per le prestazioni sanitarie che sono le più lunghe di sempre e non si può pensare di ridurre le liste d'attesa finanziando il privato. Poiché c'è questa pandemia oncologica, gli oncologi ci chiedono il coraggio

di cancro al polmone, che è la prima causa di morte per tumore: sa quanti sono i nuovi casi di cancro al polmone? Sono 44.000 ogni anno, di cui 29.000 sono legati al fumo. Spendiamo 2,5 miliardi all'anno per curare i tumori al polmone, 25 miliardi all'anno per curare in generale i tumori e qual è il modo più efficace per ridurre l'abitudine al fumo? Anche qui, non c'è bisogno di inventarci ricette che nessun altro Paese sta utilizzando, perché è già stato sperimentato negli Stati Uniti e in tutti i Paesi europei che hanno avuto il coraggio di fare questa scelta. Se si aumenta il prezzo delle sigarette, si riduce l'abitudine al fumo e questo vale soprattutto tra i giovani i giovani e tra le fasce più fragili della popolazione, quelle più economicamente svantaggiate, che poi sono anche quelle che fanno meno prevenzione. Si stima che, se raddoppiassimo il costo delle sigarette, se ne aumentassimo di cinque euro il costo per pacchetto, così come ha fatto la Francia,

signor Sottosegretario, vorrei che veramente dimostraste al Paese di essere patrioti così come avete detto in campagna elettorale. Un patriota difende il Paese e i suoi cittadini; pertanto, sposare progetti che non faranno altro che frammentare ancora di più il Paese, come l'autonomia differenziata, o inventarvi ricette che non esistono da nessun'altra parte del mondo (e un motivo ci sarà), come il premierato, concentriamoci su quello che possiamo fare. Rafforziamo la sanità pubblica, facciamo in modo che non si torni a tagliare e a indebolire il più grande e più importante pilastro che abbiamo, cioè il nostro Servizio sanitario nazionale, che deve restare pubblico,

il fatto che c'è una differenza nella spesa *pro capite* non solo tra l'Italia e gli altri Paesi europei di circa 900 euro, ma tra il Nord e il Sud del Paese di circa 800 euro. Ciò significa che noi stiamo

di metodo e una di merito. Quella di metodo non è semplicemente una critica a come è fatto il Documento: ieri in 5a Commissione si è visto che ci sono riferimenti a tabelle che non si trovano, note che non hanno riscontri, si vede che è un Documento fatto in fretta. Tuttavia, i limiti di metodo di questo Piano sono molto gravi per due ragioni: la prima è che siamo di fronte ad un cambiamento paradigmatico delle politiche di bilancio a livello europeo; la seconda è che questo tipo di documento, che riguarda cinque anni più due, se si fanno le riforme, quindi sette anni del futuro del nostro Paese a partire dal 2025, dovrebbe coinvolgere tutto il Parlamento, perché stiamo parlando di un orizzonte che va oltre questo Governo e che quindi richiederebbe un confronto autentico nel Parlamento e fuori dal Parlamento, con le parti sociali, con i cittadini, con la società civile, con i lavoratori e con le imprese. Niente di questo è stato fatto. Noi oggi siamo di fronte ad un esercizio econometrico sofisticato, molto lungo, come ieri in Commissione ci ha detto

ce lo dicono le istituzioni che noi abbiamo ascoltato in audizione. Io le vorrei citare, perché se parla un senatore dell'opposizione sembra che abbia un pregiudizio politico. Si segnalano alcune carenze di informazioni nel quadro tendenziale di finanza pubblica, che avrebbe potuto assorbire contenuti normalmente presenti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, la NADEF, come auspicato anche nel documento conclusivo del Parlamento sull'indagine conoscitiva: questo lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ancora, per l'Ufficio parlamentare di bilancio mancano spiegazioni delle dinamiche dello scenario a legislazione vigente. Manca un anno, vi siete persi un anno. Manca il 2028, per cui non sappiamo che cosa succede nel 2028. E per il biennio finale, dice l'UPB, mancano le voci che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche. Non sono presenti informazioni solitamente riportate nella NADEF. Si evidenzia la mancanza di informazioni circa la rimodulazione del profilo temporale e dell'impatto del PNRR sulla legislazione vigente. Mancano le informazioni sullo scenario a politiche invariate, nonostante la legge di contabilità

tutto sembra interessante, però serve capire quali sono i documenti e quali sono le informazioni. Allora questo non è solo un tema di metodo, ma un tema cogente di politica. Vi sono, però, alcuni elementi positivi in questo documento, cioè alcune affermazioni di verità. La prima: abbiamo scoperto che il Governo che ha fatto la storia, nel suo primo anno di attività ha invertito l'andamento crescente del PIL. Lo vogliamo dire questo agli italiani, visto che Fratelli d'Italia spende molte risorse anche in propaganda sui giornali, sui quotidiani e sulla stampa? Il PIL è cresciuto nel 2021, è cresciuto nel 2022 ed è decresciuto nel 2023. Quindi, io vorrei capire che tipo di storia questo Governo ha fatto nel 2023. Inoltre, come si è detto, i tendenziali del 2024 sono stati rivisti al ribasso da parte dell'Istat. Questo significa, come ha riconosciuto ieri il Ministro, che avremo grande difficoltà a rispettare questa modesta crescita anche nel 2024. Signor Presidente, colleghi, questo ci deve far capire che le misure di politica economica che questo Governo ha realizzato negli scorsi due anni, non solo non hanno prodotto la spinta che il Governo in qualche modo millanta, ma hanno portato dei passi indietro preoccupanti rispetto a quello che era un *trend* di uscita *post* pandemica. secondo punto riguarda le ore lavorate. L'UPB certifica che, sì, è vero che è cresciuta, partendo dal 2020, la curva degli occupati italiani, e di questo noi ci rallegriamo, ma che si lavora sempre di meno e si lavora con salari sempre più bassi. Questo è un elemento che, guarda caso, si ripercuote sulla caduta del potere d'acquisto e sulla riduzione della propensione al consumo, che pure l'UPB riconosce. Tanto è vero che proprio in quest'ultimo anno è cresciuta la propensione al risparmio da parte delle famiglie italiane, segno di una caduta della fiducia rispetto al futuro. Sono elementi rispetto ai quali noi non ci rallegriamo, ma evidenziamo piuttosto un andamento sbagliato nella politica economica di questo Governo.

d'Italia, l'UPB e anche la Corte dei conti. Questo Governo costruisce, sulla base del differenziale fra quello che era lo scenario previsto dal DEF e lo scenario attuale, un disavanzo dello 0,4 che deve servire a finanziare alcune misure nel 2024. Come dice giustamente la Corte dei Conti, vi è tutta una serie di misure che il Governo ha annunciato, ma quella dimensione lì, rispetto alla previsione del PIL, permette a stento di finanziare i dieci miliardi circa per il rinnovo strutturale del cuneo fiscale. Noi siamo contenti, ovviamente, di questa misura, ma ci chiediamo dove trovino un finanziamento tutte le altre misure. le altre misure. Ieri il Ministro ha detto: non attraverso nuova fiscalità, ma attraverso risparmi e tagli. Questo è un grosso problema, perché noi abbiamo, da una parte, il tema della riduzione della spesa netta, ma dall'altra parte abbiamo due questioni molto importanti: la questione della sanità e la questione degli enti locali, che ci sono state ribadite nelle audizioni dall'ANCI e da tutti gli altri soggetti. Sulla sanità il Ministro dice che noi stiamo impegnando risorse ad un tasso di crescita superiore a quello che è il tasso della spesa netta prevista.

Nello stesso tempo, c'è il grande tema della tenuta dei conti, evidenziato in particolare - in questo caso - dalla Corte dei conti per quanto riguarda la sostenibilità della spesa pensionistica e previdenziale. Nel complesso, questo è un documento

presenti in questo documento: non ci sono le politiche e stiamo commentando semplicemente dei numeri. Il problema è che quello che stiamo commentando vincolerà questo Paese per i prossimi sette anni. Se non riusciamo a fare politica e a parlare delle politiche qui, in questa sede, in Parlamento, per ciò che riguarda gli italiani e le italiane nei prossimi sette anni, mi spiegate cosa ci stiamo allora a fare? Perché perdiamo questo tempo? Perché stiamo discutendo di cose in merito alle quali non diamo al Parlamento la giusta centralità? Mi avvio

una frase di Keynes il cui senso avrebbe dovuto essere: le politiche di bilancio vanno valutate nel contesto. Qui il problema è un altro: noi non siamo in grado di valutare questo contesto, ma soprattutto, come ha detto la Banca d'Italia,

ipotesi non corrispondenti al vero. È un esercizio che può servire per mandare un documento alla Commissione europea, ma che non serve al Paese e soprattutto non rappresenta lo scopo e la finalità del nostro stare qui per gli interessi degli italiani e delle italiane.

provvedimento, che è molto importante. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine è previsto dalla riforma della *governance* economica europea quale strumento per la definizione del quadro programmatico di finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e e riforme ed è valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale. Il quadro di riferimento esposto nel Piano include un orizzonte temporale che si estende dal 2025 al 2029. Secondo le disposizioni transitorie, durante il periodo in cui è in vigore il dispositivo per per la ripresa e resilienza, gli interventi del PNRR possono essere presi in considerazione per l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni. Inoltre, si prevede che i progetti di spesa finanziati con prestiti del Piano di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea degli anni 2025-2026 possano valere per modulare in modo più graduale la correzione del bilancio richiesta durante il percorso di aggiustamento. Il Governo intende richiedere l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni. Nel Piano strutturale di bilancio, il Governo tiene conto della necessità di ricondurre il rapporto

Il tasso di crescita della spesa netta indicata dal Governo risulta in linea con la correzione strutturale minima richiesta dalla procedura per disavanzi eccessivi del luglio di quest'anno. Negli anni 2025-2026 gli sforzi saranno concentrati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal 2026 ci saranno interventi strutturali volti a migliorare la qualità delle istituzioni e dell'imprenditoria, intervenendo in cinque ambiti: giustizia; amministrazione fiscale; gestione responsabile della spesa pubblica; supporto alle imprese e promozione della concorrenza; pubblica amministrazione. Ringrazio il ministro Giorgetti, che non ha avuto sicuramente un compito facile, dopo la sospensione del Patto di stabilità nel 2020 e le spese e le politiche assistenzialistiche messe in campo dal Governo giallorosso, nel rimettere in carreggiata il Paese con politiche che vogliono invertire la tendenza assistenzialistica, per riportare l'Italia alle sue sacre origini di un popolo che lavora e produce. documento ambizioso, ma realistico», queste le parole che ha utilizzato il Ministro per definirlo e che facciamo nostre, guardando alla situazione reale di oggi, con una prospettiva futura ambiziosa: correggere in corsa con gli obiettivi ben saldi, ma soprattutto con i princìpi di centrodestra che caratterizzano le nostre azioni: rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale per sostenere le famiglie e i redditi deboli e accorpare le aliquote Irpef nei tre scaglioni per sostenere le imprese; misure a sostegno della natalità e delle famiglie numerose per contrastare la denatalità che inevitabilmente impoverisce sotto tutti gli aspetti, perché parliamo di 350.000 persone in meno

di risolvere questa cosa. Il primo intervento è stato appunto il decreto-legge sulle liste d'attesa e continueremo a immettere quelle risorse per portare la sanità verso i numeri che ci siamo prefissati, anche in linea europea. A pagare non saranno cittadini e imprese, ma i tagli saranno fatti anche sulla spesa pubblica. Qui si parla di dover rivedere anche le risorse all'interno dei Ministeri, utilizzando la utilizzando la digitalizzazione e cercando di avere un monitoraggio della spesa pubblica. Sentendo gli interventi qui in Aula, mi chiedo se si sia letto il Piano strutturale di bilancio, perché mi pare che al suo interno siano delineate ben chiare le azioni che nei prossimi anni si vogliono mettere in campo, analizzando le criticità che bloccano la crescita e frenano gli investimenti, partendo proprio dalla giustizia,

Sul miglioramento dell'ambiente imprenditoriale è prevista una legge quadro sulle piccole e medie imprese, per favorire l'aggregazione, la crescita dimensionale e il passaggio generazionale. famiglia e della natalità, per contrastare la tendenza demografica, facciamo riferimento a quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che mira a completare tutti gli investimenti per i servizi complementari, per la prima infanzia, per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e il bilanciamento degli incarichi di cura, nonché per migliori prospettive economiche ed occupazionali per le donne. Oggi ho sentito tirare in campo di nuovo la questione dell'autonomia differenziata,

questo grande divario si è formato proprio adesso che stiamo gestendo in maniera centralizzata tutti gli strumenti dello Stato; proprio questa gestione centralistica ha portato a tali divari.

vi fa più urlare davanti al popolo, vorrei utilizzare una frase che pronunciò Alcide De Gasperi nel momento in cui si parlava dell'autonomia trentina e che vorrei faceste vostra: faceste vostra: è «tutto un complesso di organismi e di criteri amministrativi che noi comprendiamo sotto la parola d'ordine "autonomia". Trovate forse meno esatta la parola? Può essere, ma noi l'abbiamo tolta bell'è fatta dal nostro vocabolario politico locale per significare: la migliore amministrazione possibile, fatta tutta per il popolo e più che possibile per mezzo del popolo stesso».

avvenga oggi, a soli due giorni dalla ricorrenza di quel maledetto 7 ottobre, quando persero la vita più di 1.400 persone e ne furono rapite 250,

che tutti riconoscano l'esistenza di Israele, per avviare un'effettiva possibilità di pace giusta e duratura. *(Applausi)*.

sul Piano strutturale di bilancio non scomoderei né De Gasperi né Keynes, che ho sentito evocare a vario titolo nel corso della discussione.

ancora sotto di 9 miliardi, una cifra che la dice lunga sulla nostra capacità di fare investimenti pubblici in questo Paese e su quello che ha fatto questo Governo. Ricordiamoci che quando il Governo si è insediato avevamo un PIL del più 3,3 per cento, con una crescita

la crescita del nostro Paese. Eppure la prima cosa che ha fatto questo Governo è stata congelare l'attuazione del PNRR per dieci mesi, per ridisegnare l'allocazione dei centri di potere, togliendoli al MEF per portarli alla Presidenza del Consiglio. Mi sembra che i risultati li stiamo vedendo anche anche nel PNRR salute, che sta andando particolarmente a rilento e il 2026 è domani. Non scomoderei neanche De Gasperi, come ha fatto la collega che mi ha preceduto, perché delle nuove generazioni non c'è proprio traccia gli statisti qui non ci sono e sinceramente non si ritrovano in questo Piano strutturale di bilancio. Non è che lo dico per fare l'opposizione; sinceramente avrei preferito stare in quest'Aula e nelle Commissioni a fare un grande patto sociale intorno intorno alla costruzione di una linea di remissione del debito nei prossimi sette anni e per affrontare le grandissime sfide che abbiamo. Ciò non è avvenuto, mentre è avvenuto tutt'altro, e i risultati sono quelli che abbiamo di fronte, ossia un Piano confuso:

della Camera, il CNEL o Confindustria). Lo stesso Ministro, per sua ammissione, parla di incertezza, cioè ci dice che questo quadro è delineato in una fase di incertezza perché il contesto è tale, non si sa bene quello che può accadere, quindi anche le misure che sono previste

per le cose che sono già state dette dai colleghi. Qualcuna di queste cose la vorrei riprendere. Abbiamo un'unica certezza in questo Piano strutturale di bilancio, e cioè che dobbiamo restituire 13 miliardi l'anno: questo è certo

e un taglio della spesa pubblica, questo a casa mia si chiama *austerity*. Pertanto, non ho capito alcuni toni trionfalistici su questo Piano. Mi sembra che stiamo tornando ad una fase passata, senza aver imparato la lezione. Non serviva

riforma, e senza le riforme dovremo restituire queste risorse non in sette anni, ma in cinque. Inoltre, mi chiedo: dopo la lettura del Piano, sulla spesa sociale, e cioè il nostro sistema di *welfare*, che cosa vogliamo fare? Nel Piano strutturale

la tenuta del sistema previdenziale è estremamente a rischio, oltre a condannare gli anziani di domani, che - lo voglio ricordare - saranno la maggioranza di questa popolazione, a situazioni di indigenza e di povertà. Dall'altro lato, sulla spesa sanitaria si fanno tante affermazioni continuando a pensare di eludere il problema con un aumento della spesa sanitaria in termini assoluti, quando in termini percentuali, come ci hanno ribadito tutti (compresa la Corte dei conti), stiamo scendendo a livelli inferiori a quelli che avevamo negli anni dei tagli, quando cioè abbiamo dovuto veramente ridurre la spesa sanitaria (dal sotto in termini percentuali; anche se continuate a dire che non è vero, questa cosa si scontra con la realtà dei fatti, cioè con le persone che abbandonano il mondo della salute, con la non attrattività delle professioni sanitarie e con più di 40 miliardi *out of pocket*, cioè pagati di tasca propria dai cittadini ogni anno perché non riescono ad avere accesso al Servizio sanitario nazionale. *(Applausi)*. errare è umano, ma perseverare è diabolico. Adesso ci siete voi: una proposta di riforma della tenuta del *welfare* per i prossimi venticinque anni la dovete fare e ce la dovete mettere sul tavolo; avreste dovuto farlo in questo Piano strutturale di bilancio, in cui invece non c'è nulla, nulla, neanche sulla demografia, che è il convitato di pietra in queste nostre assise, perché, con un andamento demografico come quello che abbiamo (nel 2050 avremo un lavoratore per pensionato), è evidente che non si tiene nulla. Abbiamo bisogno di una grande stagione di riforme

sono politiche universalistiche, sono politiche del lavoro femminile, dell'occupazione, sui salari, sulla casa, sui servizi. Se in questo Piano strutturale di bilancio si dice a un Comune in attivo, che ha fatto nuovi asili nido con il PNRR (badate bene), che per i prossimi anni non può assumere le maestre negli asili asili nido, è un piano della natalità questo? Ci stiamo prendendo in giro con l'insieme dei tagli che stanno avvenendo, e questo avverrà a Firenze e a Bologna, cioè nelle città che hanno i conti in ordine. Pensate a cosa accadrà nelle città che sono in dissesto: è l'abbandono dei servizi pubblici. Sull'immigrazione - mi avvio a concludere - l'INPS ci ha detto che l'attesa di lavoratori stranieri non riesce a coprire il *gap*, a causa delle persone in fuga dall'Italia: cioè l'esportazione netta positiva di quelli che se ne vanno è maggiore. Abbiamo un problema di attrattività di questo Paese sul capitale umano, di competitività delle nostre aziende e di investimento nella ricerca. E siamo ancora qui, con un Piano strutturale di bilancio che ci impegna per i prossimi sette anni e che non ha nessuna visione, se non quella meramente ragionieristica e certa di una restituzione di parte del nostro debito. Cosa giusta, per carità; ma non vorrei che poi, alla fine, l'operazione fosse perfettamente riuscita e il paziente morto.

strutturale di bilancio, sia la situazione del ceto medio, che, vedete, colleghi,

che aver immaginato aiuti anche per le categorie più in difficoltà della popolazione, che però vanno a discapito del ceto medio, debba necessariamente farci riflettere sulla lungimiranza di questo Governo.

l'assenza di politiche che il Governo sta portando avanti per contrastare il tema della diminuzione del potere d'acquisto. Considerate che una famiglia italiana, in una situazione di sostanziale equilibrio, oggi deve immaginare di pagare la sanità, come ha detto molto bene la senatrice Lorenzin prima di me, in una condizione di crollo sostanziale, che, secondo dati della

Vi sono quindi persone che in una condizione di normalità avrebbero tenuto botta, come si suol dire, perché

corriamo oggettivamente il rischio che queste stesse persone precipitino in una condizione di sostanziale povertà. Questo è un dato

il fatto che tutte le previsioni di crescita, anche sul 2024, sono state fortemente ridimensionate dall'Istat, è del tutto evidente che quello che raccontate

italiane, in termini concreti. Anche qui, parliamo di cose serie. Se il diesel aumenta, il costo del mezzo pubblico che porterà i bambini a scuola aumenterà la retta che dovranno pagare le famiglie nei Comuni. Se il costo di questi mezzi di trasporto pubblico aumenterà, ci sarà una ricaduta sui biglietti.

a proposito di Sottosegretari - che ci ricordava che avrebbe difeso la casa e le auto degli italiani?

a livello catastale le rendite degli immobili ristrutturati, perché potrebbe voler dire due cose, amici: che la revisione

che c'è una bella differenza: lo capite, amici di Forza Italia - voi che nel vostro percorso politico avete fatto della bandiera della casa una delle priorità assolute - che qui siamo di fronte al tentativo di tassarla, la casa, per gli italiani? Non solo le auto, non solo le accise. Capite, amici di Fratelli d'Italia, che prima la Meloni, andando in macchina, tirava giù il finestrino e diceva che

fare la spesa oppure rivolgersi al privato per una mammografia, perché le liste d'attesa non consentono di fare diversamente, è lì che si rompe in modo strutturale il rapporto fiduciario con le istituzioni e si mette in crisi l'asse portante del Sistema sanitario nazionale. Mi direte che i problemi ci sono, che nascono meno persone rispetto a quelle che muoiono, che le persone giustamente e auspicabilmente vivono anni, quindi costano di più alla spesa sanitaria. È tutto vero, ma quello di cui non mi capacito è il fatto che questo Governo, sul tema della riforma della sanità, non abbia ancora detto una parola in due anni. I problemi non si risolvono da soli, ma si risolvono se ci si mette la testa, se si ha un'idea di riforma strutturale, se si comincia a intervenire in maniera seria e non demagogica sulle liste d'attesa, se si mette in campo anche un rapporto proficuo tra privato e pubblico, ma sotto un'egida pubblica, se si comincia ad aguzzare un po' l'ingegno, perché il tracollo del sistema sanitario è vicino. C'è poi una

Avevate detto - ma anche qui stendiamo un velo pietoso, perché meglio del senatore Monti non potrei fare su questo tema: *ubi maior* - che la legge Fornero sarebbe stata messa in discussione e addirittura abolita. Ebbene, cittadini, amici e colleghi, sappiate che anche nelle previsioni di questo Piano la Fornero vive e lotta insieme a noi. *(Applausi)*. Questo perché non ce ne sono le condizioni; anzi, semmai in alcuni casi c'è un aggravamento delle condizioni che pone la Fornero e anche qui ricordare quelle cadute di stile, quelle azioni quasi persecutorie dell'attuale vice *premier* Salvini nei confronti di Elsa Fornero sarebbe quasi una banalità. banalità. In sostanza, questo è un piano che aggredisce, penalizza e mette fuori gioco il ceto medio italiano,

quindi un messaggio negativo di ulteriore tassazione per il Paese, senza dire però una sola parola sulla questione vera che vivono gli imprenditori italiani, che è vera e necessaria per produrre crescita. Mi al fatto di immaginare uno Stato con meno burocrazia e più semplificazioni e magari con qualche riforma della giustizia vera,

non si parla degli aggiustamenti del PNRR, della fuga di cervelli e delle misure di contrasto al fenomeno; non si parla di cultura, ma ovviamente dopo la vicenda Sangiuliano è anche abbastanza banale dirlo.

come Genova, dove si sono fatti interventi per la messa in sicurezza dei fiumi, la situazione ha retto, perché c'era il Piano nazionale Italiasicura e gli investimenti ci sono stati; in altri territori, invece, non si è potuto fare qualcosa di analogo, perché gli investimenti non ci sono più, a causa del fatto che Italiasicura è stata, sì, abolita dal primo Governo Conte, ma poi mai ripristinata neanche dal vostro Esecutivo. Io penso che

C'è stato un tempo in cui ci siamo indignati tutti perché gli studenti universitari di questo Paese protestavano fuori dalle università per la mancanza e il rincaro degli alloggi. Di questa battaglia sembra quasi essersi dimenticata ogni forza politica, ma non la nostra.

nel territorio italiano non hanno a disposizione alloggi o servizi e che, se hanno famiglie del ceto medio che non riescono ad aiutarli, spesso

Signora Presidente, è stato per me importante notare come questo dibattito sia stato aperto da una voce così autorevole come quella di Mario Monti, senatore a vita,

di attenzione che si riserva alla linea e al ruolo svolti in Europa dall'Italia dall'inizio di questa legislatura, grazie al presidente del Consiglio Meloni, al vice primo ministro Tajani

siamo, con questo piano, nella definizione di un insieme di riforme e di investimenti assolutamente concreto e pragmatico. in un momento storico caratterizzato da tendenze, da crisi altamente drammatiche, come vediamo in Ucraina e in Medio Oriente; in un momento di profonda incertezza. Il Governo del presidente Meloni, con questo documento programmatico, intende dare certezza e un termine di riferimento preciso. Ieri, il ministro Giorgetti in Parlamento sottolineava come la graduale e decisa riduzione del debito pubblico sia una necessità ineludibile e come dobbiamo tutti essere ben consapevoli del peso che hanno avuto sulle nostre finanze alcune politiche poco lungimiranti di diversi Governi che hanno preceduto quello attuale.

capacità di affrontare le criticità strutturali del Paese e di farlo in piena continuità e correlazione con gli adempimenti previsti dal PNRR, per consolidare tali adempimenti e questo percorso. Lo fa in perfetta linea con le raccomandazioni della Commissione europea, che chiedono all'Italia un allineamento agli obiettivi di crescita, di sostenibilità, di bilancio, di equità e di transizione verde, di forte capacità amministrativa, di politica industriale definita, che superi disuguaglianze territoriali e restrizioni alla concorrenza. Quindi è un piano strutturale, questo del Governo, che nasce da un'idea di economia sociale, di un mercato dinamico, aperto. Nasce dalla volontà di rendere la nostra Nazione un luogo più attraente per gli investimenti e più competitivo. Il in altre parole, quanto l'Unione europea sollecita da tempo e definisce, innanzitutto, linee di intervento che siano in grado di rafforzare le sinergie imprenditoriali nella nostra Nazione. Parlo di energie imprenditoriali, perché è qui che sta la crescita sta negli imprenditori, negli agricoltori, nei ricercatori, negli artigiani e in tutte le categorie che fanno la crescita del Prodotto nazionale lordo, auspicabilmente da aumentare, ma è un fatto reale, quali che siano le interpretazioni sui numeri decimali di cui si sta discutendo e si è discusso anche in quest'Aula. in quest'Aula. Desidero ricordare, perché è fondamentale, che il piano mette al centro il lavoro, presidia il sistema di ricerca e innovazione tecnologica, insiste sulla modernizzazione degli strumenti finanziari per gli investimenti, agisce sullo snellimento della burocrazia e accompagna l'evoluzione del mercato del lavoro. Tutto questo in una visione strategica di insieme della manovra di finanza pubblica a medio termine, ma anche a medio - lungo termine, se consideriamo come tali sette anni di orizzonte. Non c'è dubbio che, nel lungo termine, la sostenibilità del *welfare* dipenda, anche e soprattutto, dalla curva demografica. Il piano intende favorire risposte anche sotto questo profilo, per contrastare il terribile terribile declino che negli anni futuri ci vede oggetto di forte preoccupazione, non soltanto nostra, ma di altri Paesi occidentali, soprattutto in Europa. Il messaggio del Governo con questo piano è chiaro: non lasciare indietro nessuno. Il sistema Paese è vincente se è compatto, se lo si pensa come un lavoro di squadra. Mi soffermo su due punti che credo siano rilevanti oggi: il primo è quello di una *governance* efficace e pragmatica che è la grande sfida, non solo nostra, ma dell'intera Unione. Il rapporto Draghi lo evidenzia apertamente: sono necessari almeno 750-800 miliardi di euro in investimenti aggiuntivi annui per raggiungere gli obiettivi europei prefissati. Ci vuole un'Unione europea che sappia rispondere, perché, se vi è una criticità che frena gli investitori stranieri, questa è proprio il complesso quadro normativo dell'Unione europea, con oneri eccessivi legati alla reportistica nazionale, per esempio alla *due diligence*; questioni e adempimenti che sono, per la maggior parte delle imprese, un ostacolo agli investimenti. Proprio ieri ho avuto un interessante incontro e una possibilità di approfondimento con un'importante istituzione, la Camera di commercio statunitense in Europa, ho incontrato una delegazione di una quindicina di alti dirigenti di multinazionali che operano in Europa e in Italia. L'appello lanciato all'Italia - e la fiducia allo stesso tempo legata ad esso -

migliaia e migliaia di tonnellate di documenti per adempiere a queste norme che sono pensate in modo teorico, per un mondo perfetto. Ricordiamoci che il rapporto Draghi

ieri in Senato, nei settori critici per la nostra crescita: l'energia, la trasformazione verde, la sanità, i *device* (ossia l'aspetto non soltanto farmaceutico, ma anche delle macchine, delle strutture e delle cose di cui la sanità ha bisogno)

Non mi è stata illustrata l'altra faccia della medaglia e mi sono venuti dei dubbi perché potrebbe essere una cifra assolutamente ragionevole se il fatturato lo giustificasse. Sono però adempimenti e restrizioni al *business environment*, il clima degli investimenti, che fanno pensare. L'impegno del Governo Meloni sul piano interno ed europeo è questo, e se c'è coerenza nel Governo sono fiducioso che con la prossima Commissione e il Parlamento che si è insediato si procederà e si lavorerà con un'intesa che sia la più ampia possibile fra i Gruppi parlamentari. Se il fine è rilanciare la produttività, accelerare l'innovazione e aumentare le connessioni per l'Italia e l'Europa attraverso veri e propri *hub* digitali, logistici ed energetici, la transizione sta nelle nostre mani.

Fontana. Uno dei temi fondamentali del convegno era la capacità di creare degli spazi economicamente e geopoliticamente sempre più significativi e aggregati verso Occidente, con l'Europa,

come le alternative infrastrutturali alla via della seta e ad altre dimensioni, che possono favorire la spinta, attraverso l'Italia,

Questo vuol dire che la scelta che avete fatto - io non la condivido, però ce l'ha spiegata il ministro Giorgetti - di realismo e prudenza va contro questa impostazione. Però, se non si fa questa scelta che alcuni hanno indicato, non potete dire che questo piano

grazie al fatto che i lavoratori dipendenti e i pensionati pagano le tasse, perché questo avanzo di bilancio è frutto esclusivamente di tale dato, mentre abbiamo appena approvato un *omnibus* che prevede un condono tombale per coloro che invece non pagano le tasse. Ora noi abbiamo a disposizione queste risorse e dovremmo trovarne delle altre. Ieri abbiamo sentito dire che trovarne altre tutti devono fare sacrifici: è una falsità che tutti devono fare i sacrifici, perché se applichiamo quello che prevede la Costituzione, ognuno dovrebbe contribuire a seconda del proprio reddito e delle proprie condizioni. vuol dire, ad esempio, prevedere una progressività nella tassazione, che è esattamente il contrario della *flat tax* e, allo stesso tempo, chi più ha, più deve pagare. Però

opposte. Il problema è - come ho spiegato, o almeno ho cercato di dire - che se, ad esempio, i Comuni dicono che non sono più in grado di fare investimenti, anzi ritrovano con l'acqua alla gola da questo punto di vista, e noi pensiamo di scaricare sugli enti locali ad esempio una contrazione della loro capacità economica e quindi del ritorno delle risorse, come faranno a garantire i

Poi mi spiegate che bisogna valorizzare il capitale umano, perché così mi ha risposto il ministro Giorgetti. Il capitale umano si valorizza

non c'è alcuna proposta di intervento pubblico nell'economia. Voi sapete benissimo - e chi non lo sa, se è troppo giovane, basterebbe che guardasse a cosa è avvenuto in passato - che il nostro Paese si è sviluppato,

Signor Presidente, l'occasione della discussione sul piano strutturale di bilancio di medio termine e l'intervento di ieri alle Commissioni riunite del ministro Giorgetti, una discussione che noi consideriamo quasi unica, in realtà, sulla manovra economica che ci accingiamo ad affrontare nel Parlamento (peraltro quest'anno alla Camera, quindi con il Senato che sarà, ahimè, già lo sappiamo, in una funzione un po' ancillare, in questa sorta di monocameralismo di fatto che da diversi anni si è andato realizzando), sono momenti che io valuto in maniera unitaria. Noi ovviamente condividiamo gli obiettivi perseguiti. Il Gruppo Forza Italia è fautore di un europeismo operoso, non subalterno. subalterno. Alcuni criticano le nostre posizioni. Noi non siamo per un europeismo che accetti qualsiasi cosa (e citerò un episodio clamoroso di queste settimane), ma vogliamo un'Europa che sappia difendere se stessa. Ricordo ogni giorno a me stesso che ogni anno in India

irregolare o sleale, ci fanno una forte concorrenza e che crescono. In India, su un miliardo e mezzo di abitanti, i poveri sono sicuramente centinaia di milioni; tuttavia, il numero di ingegneri che si laurea in India supera quello dell'Europa. C'è quindi un mondo nel quale o l'Europa, con 500 milioni di persone, coesa, compete nella tecnologia, nella scienza, nell'industria, oppure non andiamo da nessuna parte. La Baviera, la Catalogna, il Veneto, la Sicilia o non so quale regione della Francia da sole non batteranno

Inoltre ho ammirato molto il piano che recentemente ha redatto il presidente Draghi, che conosco da epoche lontane e che stimo. Il presidente Draghi ha ideato un piano che costa 800 miliardi di euro l'anno.

Draghi ha fatto un piano da 800 miliardi l'anno ed io sarei in grado di farne uno da 900 miliardi di euro l'anno, perché ho la mia penna, ho dei pezzi di carta, mi metto a scrivere e faccio un piano che costa 900 miliardi. Si è detto che il Presidente Draghi ha sommato gli investimenti disponibili, quindi forse sono di più. il piano Draghi va benissimo, ma o l'Europa fa un'iniezione di risorse e crea un debito comune, ma poi bisogna spiegarlo ai Paesi virtuosi del Nord Europa (e lo dico guardando il presidente Monti, che di queste cose ha un'esperienza

Tutti hanno alleati strani, se vuole parliamo della commissaria spagnola designata alla concorrenza che porterebbe, da socialista, alla distruzione dell'industria europea *(Applausi)*, quindi spero non diventi commissaria per la transizione ecologica, perché con quelle ricette vedremmo la distruzione della Volkswagen, della Stellantis e di tutte le altre. Quindi pensate ai vostri alleati.

So che è difficile, ma questo Governo - e ho concluso davvero, signor Presidente - da gennaio ad agosto ha fatto crescere le entrate fiscali di 22 miliardi rispetto all'anno passato, senza aumentare le aliquote, senza aumentare le tasse, semmai diminuendole, perché è cresciuta la base produttiva, abbiamo superato i 24 milioni di occupati, sono scesi al 6,2 per cento i disoccupati. C'è una politica che fa crescere la base imponibile e per questo lo Stato incassa più tasse; non la politica dello sperpero e del reddito di cittadinanza, che aumentavano lo sperpero e faceva crescere la disoccupazione e la povertà, che non è stata abolita. *(Applausi)*. Con noi e con questo Governo cresce l'occupazione, diminuisce l'inflazione, diminuisce la disoccupazione e vogliamo che questo piano europeo ci aiuti. Quindi, oltre al piano Draghi - il mio piano di 900 miliardi, appena l'inchiostro si esaurisce, finisco di scriverlo - speriamo che l'Europa cresca. Quindi il nostro è un europeismo positivo e attivo, non quello dei socialisti spagnoli dell'auto elettrica domani mattina, che creerebbe tanti di quei disoccupati che il senatore Boccia impiegherebbe mesi interi per ascoltarli. *(Applausi)*.

mi consenta, per suo tramite, una battuta rivolta al collega Gasparri, che ha una fantasia smisurata, tale perfino da consentirgli di paragonare se stesso al presidente Draghi: complimenti. La fantasia non si ferma neanche quando si vuole autoattribuire i i meriti per 22 miliardi di maggiori entrate; se andiamo bene ad analizzare, vediamo che non sono certo dovute alla spinta e alla crescita di questo mirabolante Governo, che in realtà non ha fatto assolutamente nulla (tra poco argomenterò meglio). Andrei piuttosto a guardare quella stessa spinta che questa maggioranza ha ucciso, cioè il superbonus, che ha spinto la crescita del Paese (sì, quella misura) per anni di fila, facendo ridurre persino il debito di oltre 20 punti percentuali, cosa di cui oggi vi fregiate, senza però dire da dove arriva. *(Applausi)*. Non fate altro che parlare continuamente dei problemi che avreste ereditato da chi vi ha preceduto, ma non parlate mai dei meriti, che sono stati messi nero su bianco da Istat (la settimana scorsa o due settimane fa) e che vi consentono di fare alcune cosette di cui volete prendervi i meriti in questo piano strutturale di bilancio, senza però averne le capacità. Questo le capacità. Questo Governo sembra guidare a fari spenti nella notte, per vedere se poi è così difficile morire (per andare in scia alle citazioni di ieri del Ministro). Secondo me scopriremo solo se siete capaci di finire di distruggere il Paese oppure no. Lo dicono tutti gli auditi su questo piano strutturale di bilancio. Bankitalia e UPB hanno rivisto al ribasso

non avete imparato la lezione e quindi tagliate, tagliate e tagliate sulla spesa, andando in una direzione di *austerity* e mirando esclusivamente a ciò che ieri il Ministro ha definito il suo dovere morale, che quello dell'avanzo primario, questo dogma che aleggia sul nostro Ministero dell'economia e delle finanze e che l'Italia ha rispettato, negli ultimi trent'anni, per circa venticinque anni. L'Italia è stata prima in Unione europea per avanzo primario; peccato che questo dogma non sia assolutamente servito a far crescere il Paese, che infatti ha visto, in questi venticinque anni passati,

l'abbiamo abbandonato, nella legislatura passata; infatti l'Italia ha registrato crescite record, che non si sono viste in nessun altro Paese europeo. Sento dei borbottii, però lasciatemi dire che basta andare a guardare i dati dell'Istat, non è che me li sto inventando io. Smentitemi: una crescita dell'8,9

tutto l'impatto della bravura di questo Governo, siamo allo zero virgola. E allora si annuncia una manovra di sacrifici per tutti, una manovra lacrime e sangue: il ministro Giorgetti "mani di forbice" taglia su tutto. Cominciamo con la sacralità della casa, ribadita nottetempo dopo le improvvide parole di ieri del Ministro in audizione sulla revisione dei dati catastali, che hanno creato creato un po' di subbuglio; stamattina era subito lì a mettere la toppa al buco che aveva creato. Però voi fate dei tagli sulla casa, che quindi celano maggiori uscite per i cittadini. Non le volete chiamare tasse? Chiamatele come vi pare, però comunque mettete la mano nella tasca degli italiani, che tanto vi piace. Ve li ricordo brevemente: avete aumentato dall'8

e quindi gli altri li tagliate, perché dovete fare i vostri, non perché non ne volete fare nessuno. *(Applausi)*. Abbiamo poi lo *stop* alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte degli *under* 36 e alla detrazione dell'IVA al 50 per cento per l'acquisto di case con classi energetiche energetiche superiori perché la transizione ecologica proprio non vi piace e il futuro del pianeta non vi interessa. Pensate solo a oggi e ieri. Non Non parliamo poi dell'inaccettabile immobilismo che c'è stato da parte del Governo sul caro mutui per gli aumenti esagerati dei tassi di interesse, con profitti esagerati per le banche. Infatti, mentre sono stati subito pronti ad aumentare i tassi di interesse sui mutui, si sono dimenticati di aumentare i tassi di interesse sui

di 135. Il debito pubblico quindi in mano a voi purtroppo quest'anno sale al 135,8 per cento. Tornando sui tagli, mi sono dimenticata quelli alla sanità, che sono stati citati benissimo dai colleghi. Ieri il Ministro ha tenuto a precisare che la spesa in sanità non subirà la mannaia sotto l'1,5 per cento, come in altri comparti, ma viene preservata. però ben specificato di quanto. Siccome i documenti dicono che rimane comunque intorno al 6,2 per cento del PIL, vi rendete conto che ciò vuol dire che la spesa reale anche stavolta si riduce rispetto al passato. Capisco che a voi piace tanto parlare di numeri assoluti e il concetto di percentuale sul PIL, quando si parla di sanità,

la NATO, questo concetto lo capite benissimo, tanto che stiamo per spendere 2,8 miliardi per nuove armi da dare al nostro Esercito. 2,8 miliardi! Le voci dicono che invece sulla sanità quest'anno ci mettete qualcosa tipo 900 milioni: *wow*! 2,8 miliardi per le armi, 900 milioni per la sanità, che vi sta tanto a cuore. I numeri però dicono che non è vero, che la state definanziando e che volete tornare al passato. concludo con un piccolo passaggio. Brunetta durante le audizioni ci ha detto che far diminuire la spesa reale, cercando di ottenere la crescita, è una scommessa. Voi governate così: fate le scommesse sulla pelle dei cittadini italiani. Complimenti, noi invece siamo contro il gioco d'azzardo patologico e vi diciamo che sulla pelle dei cittadini italiani non si può scommettere, non vi dovete azzardare. L'ultima chicca: il Ministro ha detto che l'aumento del potere d'acquisto non spinge i consumi, ma spinge i risparmi. Mi verrebbe una citazione un po' meno aulica di quelle fatte dal Ministro ieri, quando ma è del mestiere questo? Sanno tutti che questo principio vale per le classi agiate del Paese, che non hanno problemi nel quotidiano e quindi, se hanno un soldino in più in tasca, lo mettono nelle banche amiche che magari a loro fanno dei tassi di interesse più alti, ma non vale per le classi meno agiate, per quelle che non hanno niente,

bui. Le classi più numerose di questo Paese, se hanno un soldino in più in tasca, lo spendono e l'abbiamo dimostrato sempre noi, quelli incompetenti che c'erano prima di voi, quando a chi era in difficoltà abbiamo dato il reddito di cittadinanza e quel reddito di cittadinanza ha fatto aumentare i consumi nel Paese. I dati dicono che anche su questo il Ministro ha sbagliato. Tornate a scuola.

colgo l'invito della collega Pirro e torno a scuola, cercando di tornare nel mio ruolo precedente

persone che sanno quello di cui si sta parlando - se il termine di paragone era il *lockdown*, è abbastanza probabile che nel momento stesso in cui uno esce di casa e ricomincia a lavorare il PIL cresca un po'.

prendersi il merito del fatto che si cresceva del 3 per cento o giù di lì. Invece, è molto più utile cercare di capire come sta andando la nostra economia in rapporto agli altri Paesi europei, perché sapete che c'è quella cosa che si chiama congiuntura, che significa che, indipendentemente da quanto bene o quanto male possiamo fare noi, c'è un'economia internazionale che per molti motivi - guerre, costi delle materie prime, inflazioni, decisioni di tassi da parte di banche centrali - a a un certo punto cala per tutti e, se tu stai facendo meglio degli altri, è probabile che sei bravo, se tu stai facendo peggio degli altri, devi cominciare a capire se è una questione esclusivamente tua, oppure se oggettivamente stai facendo degli errori. punto di vista - mi riaggancio a una osservazione che ha aperto questo dibattito - un esempio di scuola di un periodo in cui tutti crescevano e noi non crescevamo, anzi stavamo andando in recessione e quindi bisognava valutare se si stava sbagliando oppure se si stava facendo qualcosa di

tagliare eccessivamente le spese ha provocato dodici trimestri di recessione, mentre il resto del mondo cresceva. Probabilmente, quindi, le cose non andavano benissimo, non era una politica corretta da fare.

dopo la cura si è arrivati al 130, evidentemente la cura non ha esattamente funzionato. *(Applausi)*. Ciò significa che abbiamo inflitto delle sofferenze all'economia per far aumentare il rapporto debito-PIL. Basta, quindi, con queste lezioncine, è impossibile che ogni volta, quando uno ha i numeri che ormai sono

ma lo è perché è ridicolo sentir parlare di proiezioni a sette anni. L'Unione europea, per carità, ha le sue regole, si mettono tutti insieme in una stanza e decidono che il

è sciocco, cioè non risponde alle esigenze dell'economia italiana. Tuttavia, il compito che veniva assegnato in quel momento in quella stanza non era disegnare il Piano strutturale di bilancio ottimo per l'Italia,

del PIL che nel 2031 crescerà del 2,2 per cento. Spero sia piuttosto chiaro a tutti in questa Aula che nel 2031

ma chi lo sa? Adesso scoppia la pace nel mondo, la guerra nel mondo, si trova più petrolio, se ne trova di meno: non sappiamo cosa succederà l'anno prossimo, figurarsi se sapremo che cosa succede nel 2031. Il passato è costellato di sfondoni clamorosi fatti sulle proiezioni a tre anni

cui tutti quei conti fatti in passato subivano le famose revisioni progressive. È la stessa roba delle società di *rating,* delle banche e così via, quando il Fondo monetario internazionale fa le previsioni per l'anno dopo e così via, e poi fa le revisioni al ribasso o al rialzo. Che cosa significa? Significa che io vedo come sta andando e poi man mano, alla fine, coincide proprio con quello che ho detto, che ho revisionato un'ora fa.

così speranza, buoni propositi, ma una cosa è certa: in questo momento sta succedendo una cosa che non sempre succede e non è sempre successa in passato.

è usuale. In questo momento in Francia il nuovo Governo, che non sa neanche tanto bene dove vorrà andare e se troverà supporto per queste cose, punta ad avere un *deficit* del 6,1

ci arriverà. Succede che sono scarsi loro o siamo bravi noi? Probabilmente un po' tutte e due, mi verrebbe da dire, perché di solito, nei periodi di ordinaria amministrazione, dove non è possibile fare chissà quali cambiamenti o chissà quali eccessi di *deficit* o di tasse, o similari, la regola migliore è quella applicata tendenzialmente dai Governi di centrodestra; motivo per cui economicamente tendono a performare meglio di quelli del centrosinistra, vale a dire lasciare abbastanza in pace i cittadini. *(Applausi)*. se non si fanno dei cambiamenti epocali in termini di *deficit* e di debito, è meglio lasciare in pace i cittadini; ridurre al minimo gli incomodi alle imprese; cercare di sostituire delle tassazioni invasive con dei sistemi forfettari tali per cui uno non deve diventare matto, magari per per pagare la stessa cifra di tasse, facendo però una fatica incredibile con certi numeri e cifre. Quello che stiamo cercando di fare noi in questo momento è abbastanza chiaro e sembra che funzioni: a

per poter rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e la situazione un po' migliora. Sarebbe bello riuscire ad avere la possibilità di investire di più, perché potremmo permettercelo. In questo momento, come saldo commerciale, noi stiamo molto meglio rispetto alla Francia. Quindi, potremmo permetterci più più investimenti, che farebbero un gran bene alla nostra economia, e scenderebbe il rapporto debito-PIL. Purtroppo, le regole sono queste. Ripeto che noi facciamo buon viso a cattivo gioco, ma almeno partiamo con una bussola: non disturbare più di tanto i cittadini. D'altra parte, i risultati sembra ci stiano dando ragione.

il concetto semplice secondo il quale è inutile programmare a medio termine, anzi è perfino dannoso farlo. Io mi se un Governo rinuncia a una programmazione di medio termine, se una maggioranza non ha alcuna idea del futuro del Paese e continua a programmare in maniera trimestrale, esattamente come fanno gli *influencer* per vendere un prodotto, questo Paese finisce in recessione. Lo dico al collega Borghi: il Paese finisce in recessione, perché questo è l'esito naturale dell'assenza di una programmazione economica e sociale. Ecco perché consideriamo questo Piano strutturale di bilancio di medio termine un'occasione sprecata. È un'occasione sprecata proprio perché il fatto che, per un Paese in procedura di infrazione come l'Italia per *deficit* e debito eccessivo, sia aperta in attuazione del nuovo Patto di stabilità una componente correttiva di finanza pubblica non inferiore allo 0,5-0,6 del PIL, della durata del Piano, avrebbe richiesto un progetto, una strategia industriale ed economica, una capacità cioè di unire il Paese e non di dividerlo. Sono mancate tutte le forme di partecipazione e di coinvolgimento dei corpi intermedi. È mancato il coinvolgimento preliminare del Parlamento. Siete qui, questa mattina, addirittura a denunciare l'inutilità della programmazione a medio termine. Io mi chiedo come potete pensare di aiutare questo Paese ad uscire da una fase molto difficile. *(Applausi)*. Ho ascoltato anche le importanti e, come sempre, interessanti riflessioni del presidente Monti in materia di sostenibilità finanziaria e di politica economica europea.

quando questo Paese aveva ancora le misure restrittive per uscire dalla pandemia. Ora, solo con questi dati, visto che la produzione industriale dovrebbe rappresentare all'incirca un quinto del prodotto interno lordo, voi state sovrastimando la crescita. voi state sovrastimando la crescita. Lo avete fatto nel 2024, continuando a parlare, fino a poche ore fa, dell'1 per cento. Invece adesso ci dite, per ragioni di realismo e prudenza, pensate allo 0,8. Non dite quali sono gli elementi di correzione dei conti pubblici. Non indicate nessuna misura per incorporare una crescita inferiore all'1 per cento e continuate a sovrastimarla per il 2025-2026-2027, senza alcuna idea dello sviluppo economico e sociale di questo Paese. Continuo a pensare che voi non abbiate un piano ambizioso e realistico tra le mani, come ha detto il ministro Giorgetti. Voi avete il primo tradimento vero del programma di centrodestra e non avete alcuna soluzione per raccontarla agli italiani. Avete fallito sul terreno classico della destra: lo sviluppo economico. Ascoltate le audizioni e i corpi intermedi, prendete in esame la possibilità che gli stessi corpi intermedi comincino a immaginare che non bastino i condoni, i concordati e le *flat tax* per costruire nuovo sviluppo economico e garantire occupazione e crescita. Continuate invece a insistere in questo scambio. Pensate di mantenere il consenso delle piccole e medie imprese promettendo condoni e un fisco *à la carte*, quando sappiamo perfettamente che oggi il problema di fronte è più grande e alto e richiederebbe anzitutto - lo dico con grande chiarezza - la soluzione dei problemi interni alla maggioranza, che sono enormi. Voi denunciate quelli dell'opposizione, ma noi siamo all'opposizione, non al Governo, e ci sarà una ragione. Chi è al Governo dovrebbe almeno dire con grande chiarezza che oggi tutte le più importanti trasformazioni economiche in atto si affrontano con la dimensione europea. Ma qual è la vostra idea di Europa?

sui grandi profitti determinati dal *web*, dalle nuove tecnologie, ma sappiamo tutti perfettamente che servono un impegno e un investimento europei in questa direzione.

Questi problemi restano irrisolti perché sono al di fuori del dibattito politico. Voi presentate non un piano ambizioso e responsabile, ma un piano truffaldino che nasconde i problemi reali del Paese.

nell'intraprendere un'agenda delle riforme sbagliate, inversamente proporzionale a quella che servirebbe. In questa fase servirebbe forse un nuovo patto sociale e non una nuova autonomia differenziata. Probabilmente dovreste essere interessati più a come governare il Paese che non a come comandarlo per occupare il potere. *(Applausi)*. Voi avreste bisogno di un cambio radicale delle agende per le riforme in questo Paese. Voi le negate.

Nel Sistema sanitario italiano c'è bisogno di una riforma e potremmo trovare qui l'unanimità immediata, se volessimo veramente mettere al centro una riforma organica per garantire un diritto alla salute universale per tutti. Voi avete però un'altra idea e la state già praticando: nel non fare niente state spingendo i cittadini che ne hanno le possibilità economiche verso le assicurazioni e il pagarsi le prestazioni. Sono gli stessi a cui dite un po' meno tasse, senza però dir loro che stanno spendendo migliaia di euro per pagarsi un'assistenza sanitaria che la Costituzione prevede come diritto per tutti. Voi state anche demolendo il patto fiscale tra cittadino e Paese proprio perché, non facendo niente, state operando verso una privatizzazione che - ahimè - produce un effetto immediato. Non c'è bisogno dei numeri: chi non ha le possibilità economiche sta smettendo di curarsi, non ha più alcun accesso alla prevenzione e non ha un punto di e presa a carico del bisogno di salute nella dimensione territoriale. *(Applausi)*. Nei grandi ospedali e negli IRCCS ormai verticali c'è una grandissima specializzazione. Attenzione come ha scritto anche Mario Draghi nel suo documento, forse sarebbe giunto il momento di ripensare la sanità e l'istruzione, la formazione e la ricerca non come una spesa, ma come un investimento in questo Paese. *(Applausi)*. Questo richiederebbe una riclassificazione della spesa. Dovremmo chiedere ad Eurostat di ripensare l'investimento in salute, perché è un investimento. Pensate alle terapie avanzate, quando sarete costretti a dire

Voi state negando un principio fondamentale della nostra Costituzione, che sono i diritti di cittadinanza. Voi così rompete l'idea comunitaria e anche nel disegno perverso - ho finito, Presidente - che avete sugli enti locali - attenzione - voi state dicendo loro di fare da soli, di andare avanti: più autonomia è uguale a più responsabilità e più efficienza. No: voi sarete costretti ad un gigantesco taglio lineare sui servizi, perché state rinunciando a un patto tra i livelli di governo. Voi continuate ad evitare l'idea che si possa governare insieme senza conflitto e sarete costretti a tagliare i servizi, ma lì c'è la spesa del *welfare*, c'è la spesa utile alla dimensione della famiglia. Altro che genitorialità, se si rinuncia ai servizi sociali nei territori, perché mettete in campo tagli lineari. *(Applausi)*. Tutto mi porta a dire che, nel che, nel non fare niente, purtroppo, spingerete l'Italia in recessione e lascerete in eredità ai futuri Governi un peso enorme per la mancanza di idee, di serietà e di responsabilità che questo straordinario Paese meriterebbe.

e non costituisce certamente un percorso di austerità, ma, al contrario, si poggia su un programma di crescita e sostenibilità. Le riforme strutturali che il Governo Meloni sta portando avanti, apprezzate in Europa e anche a livello internazionale, consentiranno - ne siamo certi - a dare nuova linfa alla crescita economica del Paese, con un aumento del PIL che si presume possa arrivare al 3,8 per cento Come ha illustrato il ministro dell'economia Giorgetti, il Piano strutturale di bilancio adotta i dati aggiornati alla luce della revisione di contabilità nazionale rilasciati dall'Istat lo scorso 23 settembre e, dopo il confronto con le parti sociali, conferma la traiettoria della spesa primaria netta, che è il nuovo indicatore univoco previsto dalla Commissione, che avrà nei prossimi sette anni un tasso di crescita medio vicino all'1,5 per cento, compatibile con il profilo stimato dalla Commissione. Il dato positivo è che il *deficit* scenderà più rapidamente rispetto alle previsioni del DEF, consentendo alla nostra Nazione di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo già nel 2026, quando il *deficit* scenderà al 2,8, con buona pace dei gufi della sinistra - pochi secondi fa ne abbiamo sentito uno - e dei detrattori che ogni giorno remano contro il Governo Meloni. In tale ambito, il Piano si ispira a una linea seria, prudente e responsabile e coerente, con l'azione che il Governo porta avanti fin dall'inizio della legislatura, particolarmente apprezzata dai mercati internazionali e dagli investitori esteri, alla luce della prudente gestione dei conti pubblici, nonché del collocamento sui mercati dei titoli di Stato, se è vero, com'è vero, che il BTP valore è andato letteralmente a ruba. a ruba. Siamo certi che i mercati apprezzeranno l'impianto della prossima legge di bilancio, che a breve sarà all'esame delle Camere,

grazie anche alle maggiori entrate fiscali, agli acquisti di BTP che si intensificheranno, consolidando ulteriormente i *rating* che le agenzie internazionali daranno al nostro Paese. Come già rilevato dal DEF dello scorso aprile, l'andamento del rapporto tra debito e PIL nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, continuerà a essere fortemente condizionato dall'impatto del fabbisogno di cassa delle compensazioni d'imposta legate al superbonus e a tutti i *bonus* partiti dal 2020. Il rapporto debito-PIL, dunque, solo dal 2027 inizierà un percorso di discesa, in linea con le nuove regole che prevedono che si riduca in media di un punto di percentuale di PIL rispetto all'uscita dalle procedure per *deficit* eccessivi. Bene ha fatto il ministro Giorgetti a prevedere, fra gli obiettivi indicati dal Piano, quello di abbattere il rapporto tra debito e PIL, anche attraverso la cessione di partecipazioni di società pubbliche. pubbliche. Giudichiamo altrettanto audace e importante da parte del Governo mettere mano finalmente e riordinare tutto il sistema italiano delle *tax expenditure*, con particolare attenzione all'ambito dell'energia e della transizione *green*. Il riordino delle spese fiscali consentirà di definire un sistema di agevolazioni fiscali basato su princìpi di programmazione, selettività e monitoraggio *ex ante*, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Il Piano contiene inoltre un rilevante insieme di riforme e investimenti, alcuni in continuità con il PNRR, prestando particolare attenzione alla riduzione del cuneo fiscale per i dipendenti che percepiscono redditi fino a 35.000 euro, all'accorpamento di aliquote Irpef (già in vigore da maggio), e alle risorse necessarie per il rinnovo dei contratti pubblici, oltre al finanziamento di misure per favorire la natalità e il rifinanziamento di missioni di pace. Ciò conferma la determinazione del Governo Meloni a lavorare per il miglioramento della competitività dell'economia italiana, promuovendo una crescita sostenibile e il contrasto al declino demografico. Al contempo, si confermano il sostegno al potere d'acquisto delle retribuzioni e l'impegno all'attuazione della legge delega della riforma del fisco, compresa l'intensificazione dello sforzo di recupero del gettito fiscale (*record* in questi anni). Anche se l'approccio da parte della Commissione europea non si è dimostrato espansivo, non accogliendo le richieste italiane di considerare diversamente la spesa per gli investimenti, il ministro Giorgetti non si è perso d'animo: con il consueto dinamismo e l'assiduo spirito di abnegazione, che caratterizza lo spirito di questo Governo, ha assicurato che ci saranno più risorse per il Fondo sanitario nazionale, per non ridurre il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, salvaguardando il livello della spesa sanitaria e assicurando una crescita superiore a quella aggregata della spesa netta.

Nel contempo vi sarà uno stop definitivo alle spese nocive, improduttive e alla stagione dei *bonus*, che hanno buttato dalla finestra decine e decine di miliardi di euro creando disastri sul bilancio dello Stato compiuti dai Governi a 5 Stelle, che probabilmente è una caratteristica positiva solo nel comparto dell'*hôtellerie*. Sebbene la revisione dei conti Istat abbia abbassato il punto di partenza, con un rapporto che nel 2023 è al 134,8 per cento del PIL rispetto al 137,3 precedentemente stimato, il debito salirà nei prossimi anni fino al 138,3 per cento nel 2026. Queste sono le conseguenze del superbonus. Dopo due anni di legislatura è chiaro ed evidente che il modo di vedere le cose al fine di governare le politiche economiche di crescita in questa Nazione è molto diverso Ma la sfida più grande - come ha giustamente detto il Ministro - è rappresentata dall'elevato *stock* di debito pubblico e dai relativi oneri d'interesse. Gli spazi, sia pur limitati, per gli investimenti pubblici concessi nel piano 2027 e una politica di bilancio prudente e credibile saranno due elementi cruciali per aggredire il fardello del debito e della spesa per interessi, alleggerendolo in modo strutturale. Pur tuttavia, all'interno della prossima legge di bilancio per il 2025 non ci saranno nuove tasse, tanto care alla sinistra, né tantomeno si procederà con tagli indiscriminati. La traiettoria della spesa pubblica netta è in linea con le indicazioni della Commissione europea ad essere pienamente sostenibile per tutta la durata dell'impegno, fino al 2031. Al contrario, il Piano strutturale di bilancio non lascerà indietro nessuno. È tutto rivolto alla crescita e mette al centro il lavoro, concentrandosi sulla sostenibilità del sistema pensionistico e sulla qualità del sistema sanitario; una crescita sostenibile rivolta alle famiglie e alle imprese attraverso sgravi fiscali, nella consapevolezza che le risorse a disposizione certamente non sono molte, ma intendono sostenere quelle priorità che garantiscono un moltiplicatore migliore, ovvero le imprese che assumono, la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, la natalità e la salute dei cittadini. Questa è una direttrice dalla quale non ci siamo mai discostati, senatore Manca. E non abbiamo tradito nessuno dei cardini della nostra politica che ci hanno sempre contraddistinto. Il Piano strutturale di bilancio inviato da Palazzo Chigi alle Camere è un documento molto più corposo della vecchia NADEF e comprende una vasta sezione dedicata alle riforme e agli investimenti richiesti per estendere il periodo di aggiustamento da quattro rappresenterà il campo da gioco dei prossimi sette anni, con effetti che riguarderanno anche la prossima legislatura. Il Documento avrà 33 collegati, dalle pensioni alle famiglie numerose, al lavoro, alla povertà, fino all'ippica e alla caccia. Esso delinea - come più volte detto - la legge di bilancio per il 2025 e si inquadra coerentemente nel solco delle linee di politiche economiche e fiscali adottate dal Governo sin dall'inizio della legislatura, con un approccio prudente e realistico, ma nel contempo ambizioso e ottimista. L'attenzione ad avviare operazioni che facilitino il lavoro di donne, giovani e soggetti vulnerabili dimostra ampiamente come il Governo Meloni sappia coniugare perfettamente il sostegno alla famiglia e alla natalità con la crescita e lo sviluppo delle imprese, in particolare quelle di piccolissima, piccola e media dimensione. Questo, cari onorevoli colleghi, è il nostro linguaggio, che ci contraddistingue e ci connota positivamente. L'Italia che produce e dà lavoro merita la massima fiducia e il massimo sostegno. Questo è lo spirito che ci ha mossi finora nelle azioni intraprese, anche a livello parlamentare. Proseguiremo in questa direzione, convinti che, con il sostegno alle imprese, l'Italia rinascerà generando posti di lavoro, crescita e sviluppo dei territori e soprattutto una crescita della nostra comunità nazionale.

6. Esauriti gli adempimenti amministrativi, io ho provato diligentemente a prendere appunti. Devo dire che, riguardando tali appunti, esco da questa discussione con un desiderio e un senso un po' di spaesamento. Il desiderio è quello di essere invitato a cena dalla senatrice Paita: se infatti a casa della senatrice, sul comodino, ci sono la foto del senatore Salvini e Salvini e costantemente la professoressa Fornero, probabilmente ne uscirebbe una cena divertente. Quindi se la senatrice Paita vuole, io volentieri mi autoinvito a cena. *(Applausi.

troviamo. Il senso di spaesamento è dovuto al fatto che in alcuni momenti di questa discussione ho avuto l'impressione che parlassimo di un documento diverso da quello che io ho provato a leggere e studiare. di cui parliamo è sempre lo stesso, io credo che di tutto si possa accusare il Governo - in questo, solo in questo, solo in questo, sono d'accordo con il senatore Monti - tranne che di non aver inaugurato una stagione nuova per la politica economica di questo Paese e, aggiungo io, anche dell'Europa, posto che il Piano ha una sua cogenza a livello europeo e anche altri Paesi lo adottano in modo analogo. Mi riferisco cioè alla programmazione. Una delle accuse principali che ho sentito muovere al Piano è stata l'assenza di una programmazione. Eppure il Piano - intendendo con tale termine familiarmente tanto il piano quanto la traiettoria di riduzione del debito debito - è tutta e solo programmazione. Si può dire - e io dall'opposizione legittimamente questo mi attendo - di non condividere quella programmazione. Si può dire di voler proporre una programmazione alternativa rispetto a quella fatta dal Governo, e lì legittimamente l'opposizione farebbe il suo mestiere. Non si può dire però che questo Piano non ha programmazione. Ho annotato una serie di aggettivi, ma li risparmio.

passaggio - che il Piano - anzi, in questo caso la traiettoria, per essere corretti - scarichi sui Governi che verranno il peso del debito. A costo di essere noioso, a pagina 31, secondo capoverso,

i Governi che verranno si trovino alla fine della legislatura, o comunque a metà di quel settennato che durerà la traiettoria, a dover scontare della spesa maggiore. È fatto appositamente.

Questo è il Governo che lo scorso anno ha messo in legge di bilancio l'importo più alto che ci sia mai stato sul Fondo sanitario nazionale e che si è impegnato per la prima volta - primo Governo nella storia - a garantire un tasso di crescita della spesa sanitaria superiore superiore a quello fissato per l'obiettivo aggregato della spesa, che è qualcosa che in Italia non si era mai visto. *(Applausi)*. Nessun Governo si è mai impegnato, all'interno e all'estero, a garantire un tasso di crescita della spesa sanitaria superiore rispetto a quello - ora parliamo di obiettivo aggregato della spesa netta, perché questo è il parametro - ma comunque superiore al tasso di crescita che si programma. Non era mai successo. Ho sentito parlare di diseguaglianze rispetto alla fiscalità e allora mi fa specie dover ricordare - penso alla tassazione sul tabacco, che pure è stata evocata - che questo è stato il primo Governo

È l'unico Governo che lo ha fatto, eppure siamo accusati di non voler tassare il comparto del tabacco. Così pure ho sentito lunari dissertazioni rispetto a paventate fiscalità aggiuntive sulla casa. Eppure, sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro Giorgetti - se qualcuno fosse stato distratto, il testo dell'audizione è depositato -

per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa. La casa per il centrodestra - fatevene una ragione - è sacra e nessuno la tasserà. *(Applausi. Commenti)*. Commenti)*. Vi invito a rileggere il testo dell'audizione e a leggere quanto è scritto sul Piano: si tratta semplicemente di garantire l'interoperabilità di banche dati che mettono insieme l'aggiornamento catastale e il godimento di *bonus* edilizi. Nulla di più, nulla di meno. Anzi, quando è stato chiesto espressamente, in sede di redazione del Piano, di fare una modifica e un aggiornamento dei dati catastali, questo Governo, ritenendolo non essenziale e non necessario per lo sviluppo del Paese, ha detto di no e di questo nel Piano c'è traccia. Per rispondere poi a una delle obiezioni che personalmente mi addolorano di più, che è quella del senatore Manca, e cioè che in questo Piano manchino politiche, questo Piano è fatto di programmazione economica e di politiche degli investimenti. Si possono non condividere queste politiche, non chiedo e non pretendo che si condividano, perché altrimenti non ci sarebbe un'opposizione e non ci sarebbe una maggioranza, ma non si può dire che non ci siano. C'è una corposa parte del Piano, direi una buona metà, che declina quelle che saranno le riforme, dividendole in settori strategici e in settori meno strategici. Quelle sono politiche - non è politica - che

secondo noi, il Paese che vogliamo lasciare, il Paese che questo Piano di bilancio che, appunto, per la prima volta, ha una programmazione quinquennale e una durata di una traiettoria di decadimento della spesa di sette anni,

Signor Presidente, siamo in grande travaglio emotivo, nel senso che scopriamo un'Aula compatta su cose che oggettivamente non pensavamo, cioè c'è un momento di tripudio dei liberali, degli europeisti, persino dei montiani. Ci sentiamo in una grave difficoltà: come è accaduto che i sovranisti "no euro, abbattiamo l'Europa, traditori della Patria perché vi sottomettete al *Diktat* europeo franco-tedesco" abbiamo fatto prima un accordo per un rientro dell'indebitamento più severo e poi abbiano fissato dei numeri che effettivamente lo fanno? È straordinario, è una riscossa storica! Abbiamo il senatore Borghi Claudio che ci spiega perché dobbiamo essere adempienti con il tracciato europeo.

sottomessi, il popolo schiacciato dallo *spread* si ribellerà e a un certo punto vi porterà tutti a rispondere. Quante volte lo avete detto da lì? Io ero nei banchi del Governo e non facevate altro. altro. Si tratta del più grande processo di conversione che io abbia mai visto e lo fate come i convertiti: in modo entusiasta. Io plaudo a questa conversione, però forse dovete dire una parola dovete dire una parola di scuse per le balle che avete raccontato in questi anni all'opposizione di tutti i Governi. Forse dovete raccontare che le promesse di rivoluzione, dall'uscita dall'euro in poi, in questo Paese servono per non fare ciò che va fatto, cioè le riforme, illudere i cittadini che un video su Instagram determinerà il ribaltamento della Commissione europea, determinerà il fatto che noi saremo sovrani. sovrani. Parlate dell'andamento della Borsa, ma per uno che è stato vicino ai poteri forti è una soddisfazione straordinaria: vi interessate più all'andamento della Borsa che al potere d'acquisto. bisogna assicurarsi che lo *spread* sia sotto 100; Giorgetti era vicesegretario quando sul muro della Lega c'era scritto: basta euro. È un momento di giubilo, quindi intanto vorrei dirvi che ci avete fatto tutti immensamente felici. C'è un problema, altrimenti lo voterei: non spiegate mai il come rispetto a nulla. Ciò che fate è prendere ciò che la Commissione europea vi ha detto, metterlo su un foglio e dire che lo farete tagliando delle spese, ma non si sa quali. Poi occorrerà rivedere il prossimo anno, perché probabilmente non saremo in grado di tagliarle tutte, quindi stiamo già scrivendo una cosa che non funziona. Quello che manca è una visione di Paese. Ma siete andati al Governo dicendo che eravate quelli identitari. Occorre un po' di identità da qualche parte. Avete un Ministro della cultura - ovviamente non c'è una politica culturale - che ieri ha fatto un discorso incomprensibile per gli appassionati di filosofia;

ingenuità, ma voi siete molto più bravi di tutti perché siete patrioti e avete capito come si governa il Paese: il Governo del Paese si fa così, mettendo i numeri della Commissione europea, facendo i video Instagram in cui dite che avete cambiato l'Europa. Davvero, Sottosegretario, avete cambiato l'Europa? Avete messo esattamente i numeri che voleva la Commissione e non c'è uno straccio di visione di Paese su nulla. Persino una visione sbagliata: mettete una visione sbagliata, dite qualcosa su qualcosa. È una continua ripetizione degli stessi slogan senza un atto di verità, un secondo nei confronti del Paese in cui si dice qualcosa del tipo: no, noi non possiamo fare quello che vi abbiamo detto, perché il debito ci impone di tenere il Paese in sicurezza, altrimenti non pagheremo le pensioni. niente di tutto questo. Questa è la cosa che non si può accettare. Signor Sottosegretario, lei può citare le pagine nn. 131, 127 e 145, ma avete scritto delle banalità sconcertanti:

energetico potevate mettere il nucleare, cioè una misura su cui siamo d'accordo. Qual è il *mix* energetico? Andiamo a pedali? Cosa volete fare? Tutto questo non si sa, perché dicendolo scontentate qualcuno. Allora, siccome non volete scontentare nessuno, quello che vi serve è prendere i numeri della crescita economica, che io dico che sono buoni, e dire che è merito del Governo. Quando il prossimo anno andremo in recessione, e ci andremo, perché sta saltando il settore automotive, su cui non state facendo niente, voi, quando andremo in recessione, direte che è colpa di chi? Dei poteri forti, un'altra volta, dopo aver fatto questa manovra? Questo è il problema. Non sono i numeri che sono dentro ma il fatto che non c'è mai un'assunzione di responsabilità sulle cose che si chiedono al Paese, sulle balle che si sono raccontate al Paese. E se volete stare al Governo con dignità, questa è la prima cosa. Io, personalmente, mi sono profondamente stancato di votare i provvedimenti del Governo che ritengo giusti, ma di non avere mai, da questo Governo, l'ammissione di un fatto: che governare vuol dire prima di tutto saper raccontare la realtà agli italiani, spiegargliela e ammettere gli errori fatti.

la discussione è andata su livelli completamente diversi, che sono più di carattere politico che non un elencare di numeri e prospettive, che sono necessariamente nel Piano strutturale di bilancio. Piano che è una nuova forma di programmazione, che è stata condivisa

delle previsioni in economia lunghe così tanti anni. Però, è altrettanto vero che in questo documento - come è stato precedentemente detto anche dal Sottosegretario - c'è una programmazione e c'è una difficoltà nell'inseguire numeri o previsioni, da un punto di vista economico, che sono oggi prevedibili in un modo ma che domani, a seconda di quelli che saranno gli eventi

fondamentalmente, vi è programmazione di quello che è l'obiettivo. Noi abbiamo due visioni completamente diverse. Probabilmente, riusciremmo ad individuare una stessa patologia da curare, ma le cure che noi proponiamo, come le cure che propone l'opposizione, giustamente, vivaddio, sono completamente diverse. Noi scegliamo una traiettoria, voi ne avete sempre scelto un'altra ed oggi purtroppo paghiamo le conseguenze di un'economia, di una prospettiva e di una cura che avete individuato che non ha portato i risultati e che fa stare l'economia italiana in questa situazione. *(Applausi)*. Noi paghiamo le conseguenze di una visione di un'economia. Noi adesso abbiamo la responsabilità di guidare la prospettiva di sviluppo economico di questo Paese perché tale responsabilità ci è stata data dagli elettori e perché gli elettori ci hanno detto che fino ad ora, come stiamo operando, stiamo portando dei risultati che loro che loro reputano accettabili, tant'è che continuano a darci un sostegno da questo punto di vista. Ci muoviamo lungo quella strada. Tutti i parametri economici ci danno ragione da questo punto di vista, e ci indicano la strada intrapresa come la strada giusta. Quindi, continuiamo su questo tracciato. Ho sentito di tutto, ho sentito addirittura parlarci, giustamente, della difficoltà nella quale si trova il comparto sanitario in Italia, difficoltà enormi. È lì dove è mancata la programmazione anni a questa parte. Ci troviamo in questo stato di salute della sanità italiana, perché è mancata una programmazione rispetto a quelle che sono state le politiche portate avanti dai precedenti Governi. Quindi, adesso i cittadini danno fiducia a noi, grazie a Dio. Pensano magari che non stanno parlando con Dracula alla presidenza dell'AVIS e magari ci reputano più all'altezza, in questo momento, per per portare avanti queste economie. Ci limitiamo a poco. A me ieri è piaciuto il riferimento che faceva nella Sala del Mappamondo il Ministro. Egli ha chiuso l'intervento iniziale con Keynes ed ha chiuso la replica con Mogol e Battisti. Ed è stato bello, perché l'economia è varia. Si può citare Keynes, si possono citare Mogol e Battisti per chiudere un intervento sull'economia, ma è questo: noi ci accontentiamo di poco; ci accontentiamo di quei risultati che ci stanno dando ragione, di avere un avanzo

Continuiamo su questa linea, con tutti interventi mirati verso la crescita di questo Paese. Continuiamo in quest'opera di piccola crescita quotidiana,

ma per fortuna che è così perché c'è un dibattito che, se rimane sul piano politico e non scade sul personale, va benissimo, è il sale della politica. Noi continuiamo per la nostra strada pensando di averla di averla intrapresa nel verso giusto e convinti del sostegno da parte degli italiani.

l'attuale maggioranza ha il consenso degli italiani. Sono d'accordissimo, è vero, ma l'ha avuto nel momento in cui contava, ossia il 25 settembre 2022. Quello che succede ora non dovrebbe condizionare le scelte politiche. Oggi dovremmo fare l'interesse del Paese, a prescindere dal fatto che i sondaggi ci diano soddisfazione o no.

come è già stato rilevato prima di me dal senatore Calenda e dagli esperti auditi in Commissione. Fratelli d'Italia e Lega hanno costruito le loro fortune elettorali picchiando duro contro l'Europa dei burocrati di Bruxelles, coloro che decidono al posto nostro, ma poi nel Piano si pongono una serie di obiettivi in buona parte condivisibili, ma che fanno sì che il documento sembri uscito dagli uffici della Commissione europea. Una brava giornalista ha scritto che questo è il piano di "Ursula von Meloni". È un piano che ammaina per sempre alcune bandiere della destra che hanno fortemente contribuito ai suoi successi elettorali, prima fra tutte le accise sulla benzina. Non solo il Governo ha cancellato le mitigazioni introdotte dal Governo Draghi, ma nel Piano si parla di allineamento tra *diesel* e verde e, siccome lo stato dei conti pubblici è quello che è, questo allineamento sarà verso l'alto, con il *diesel* che arriverà a costare come la benzina verde. Gli automobilisti esultano.

Infine il caso più clamoroso è rappresentato dalle pensioni. Non solo non vi è traccia del superamento della cosiddetta riforma Fornero, grandissimo cavallo di battaglia della Lega, ma lo stesso Ministro leghista scrive nel documento che servono incentivi per allungare l'età lavorativa. In pratica, si passa dalla Fornero alla super Fornero, a partire dal pubblico impiego, con una nuova strozzatura nel ricambio generazionale e una perdita secca di nuove competenze da immettere nella pubblica amministrazione. Questo avviene in un contesto di assoluto disastro demografico, su cui non vi è un minimo accenno di proposta per affrontare questo che è uno dei grandi problemi dell'oggi. Se ciascuno di questi aspetti è preoccupante, lo è ancora di più il quadro generale. Il Piano strutturale di bilancio prevede che nei prossimi sette anni la spesa pubblica primaria, al netto dei cofinanziamenti europei, cresca ogni anno al massimo dell'1,5 per cento. negli ultimi sette anni, la spesa pubblica primaria è cresciuta ogni anno del 5,2 per cento, negli ultimi trent'anni del 5,7 per cento. L'Italia sta quindi assumendo un impegno stringente che non potrà essere modificato per il prossimo quinquennio, un impegno probabilmente mai visto da quando è esploso il problema del debito pubblico. In questa cornice mancano drammaticamente una politica per le riforme e la crescita economica. bilancio le riforme per la competitività vengono tutte rimandate al 2027, cioè alla prossima legislatura: geniale, ci penseranno i prossimi. Il Governo, insomma, si tiene ben lontano dal mettere mano a corporazioni e interessi consolidati; fa promesse, ma toccherà ad altri mantenerle e così rinuncia al potenziale di crescita che potrebbe venire da buone riforme sulle professioni, sulle ferrovie, sull'energia idroelettrica, sui servizi postali e quant'altro. Allo stesso tempo, non c'è una politica di stimolo ai consumi e alla domanda interna, laddove il mancato recupero del potere d'acquisto sta pesando sui servizi, essenziale per recuperare il PIL, mentre l'industria arranca. Non c'è neppure un quadro certo sulle coperture della spesa corrente, sui trasferimenti alle Regioni e ai Comuni, come hanno detto all'unisono gli amministratori locali, che sono quelli che danno i servizi ai cittadini e che, quindi, se i servizi non funzionano, saranno i primi che ci rimetteranno. La sanità è al collasso, com'è già stato detto, la spesa per la salute delle famiglie italiane è cresciuta del 10,3 per cento nel solo 2023 e sono più di 4,5 milioni le persone che hanno smesso di curarsi. Agli enti locali servono più risorse e non minacce di tagli. Ma l'aspetto più odioso è che mentre si predica austerità e si rinuncia a qualsiasi ambizione sull'innovazione e la competitività, in due anni sono stati fatti ben venti condoni. Le sanatorie e i condoni sono una particolare forma di perversione; si spera di fare cassa, ma più condoni fai, meno gli evasori sono propensi a regolarizzare le proprie situazioni, con l'unico effetto di punire i contribuenti onesti, cioè quelli che reggono l'intero sistema. Insomma, questo Governo istituisce nuovi reati come deterrente contro la delinquenza e istituisce condoni contro quelli che pagano le tasse, perché se poi andiamo a vedere le sanatorie non hanno riguardato il piccolo commerciante o il libero professionista in un momento di difficoltà. Parliamo di scudi fiscali per il calcio, parliamo di criptovalute, parliamo dell'ultimo ravvedimento speciale, che è una vera e propria offesa ai contribuenti onesti. Ma vi rendete conto di come si sente un libero professionista che per cinque anni ha pagato tutto regolarmente e poi scopre che un suo omologo se ne esce versando un misero obolo? In conclusione, signor Presidente, troppe cose non vanno. Il nuovo patto ha archiviato le regole che hanno contribuito a creare un sentimento di disaffezione verso l'Europa. Tuttavia, ne ha introdotto delle altre alquanto rigide per i Paesi ad alto debito, come l'Italia. Soprattutto, manca uno strumento di debito comune per finanziare gli investimenti per l'innovazione, la transizione ecologica e la crescita economica. Forse questo Governo, che rappresenta la terza potenza economica dell'Unione, poteva strappare condizioni migliori? È possibile che di più non si poteva fare, non saremo certo noi a soffiare sul pelo di un facile populismo, non è il nostro modo, ma se queste sono le regole scelte, se questo è il campo di gioco, bisogna dire la verità al Paese: sulla Fornero vi abbiamo mentito, sulle accise vi abbiamo mentito, sulla riduzione della pressione fiscale vi abbiamo mentito. E soprattutto, scusateci italiani, non abbiamo la forza culturale e politica per fare le riforme che abbiamo promesso e che servono al Paese per navigare in questo mare. Questo sì che sarebbe un atto di responsabilità da veri patrioti, perché, vedete, siamo tutti patrioti, ma alcuni tra noi che stanno seduti dall'altra parte rispetto al sottoscritto si sentano più patrioti degli altri. Gli altri però sono patrioti intellettualmente onesti e votano contro questo provvedimento. *(Applausi)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, penso che, sul passato, molti degli interventi che ci hanno preceduto abbiano chiarito che questo Governo è cintura nera di promesse non realizzate. Questo Governo, dalle accise alle pensioni, dalla NATO all'Europa, ha cambiato idea su tutto; il bello è che noi non possiamo nemmeno esserne così tanto tristi in alcuni settori. Quello però che manca - e lo dico con rispetto al sottosegretario Freni, che su questo ha espresso il proprio dolore fisico - è che manca proprio la direzione politica: se mi mettessi, come tutti gli altri, a parlare del passato, ripeterei un copione già scritto. Sottosegretario Freni, non c'è un'idea per il futuro. Ci aspettavamo un orizzonte, una visione, un sogno; ci avete dato un compitino fatto maluccio. Viene in mente - lo dico a lei che è un uomo di grande cultura la frase celebre e pluricitata del grande filosofo Kierkegaard, che diceva: la nave è ormai in preda al cuoco di bordo e ciò che trasmette al microfono del comandante non è più la direzione, ma è cosa mangeremo domani. Ci abbiamo messo un po' a leggere le centinaia di pagine. Ci aspettavamo di trovare una direzione, ma abbiamo trovato il menù; pensiamo anche - sia detto *en passant* - che alcuni degli ingredienti non siano presenti nella vostra cambusa. Ma fermiamoci solo su questo, sulla politica. Il mondo sta volando in una nuova era tecnologica; l'Italia affoga in una palude burocratica. Siamo d'accordo su questo? Bene. Il PSB elenca le riforme. Dove sono le vostre riforme, Sottosegretario? Avevate detto - e cito la Presidente del Consiglio la madre di tutte le riforme è l'elezione diretta del *Premier*. Avete portato una riforma, votata una volta in un ramo del Parlamento e che deve ancora andare

tale ruolo. Nell'unica riforma che doveva aumentare i poteri del Presidente del Consiglio, per la prima volta nella storia delle riforme italiane, non date al Presidente del Consiglio neanche il potere di revocare o nominare i Ministri. Metti caso che vi tocca un altro Sangiuliano, o si convince da sé o vi resta lì. Avete fatto l'autonomia. Alcuni dicono che con l'autonomia spezzate l'Italia. No, con l'autonomia avete unito l'Italia, perché siete riusciti nell'impresa di unire la CGIL, Confindustria e la CEI: sono tutti contro di voi. Avete unito il Sud della sanità e il Nord delle imprese. Avete unito - caso più unico che raro - solo in questo caso persino il centrosinistra. Avete unito proprio tutto. L'unica cosa che avete spezzato avete spezzato è l'unità del centrodestra, perché c'è un partito, la Lega, che prende i voti là dove l'autonomia va fatta, e c'è un partito, Forza Italia, che prende i voti dove l'autonomia non la vogliono. Avete parlato riforma energetica. Signor Sottosegretario, le voglio bene, ma per piacere non si adonti se qualcuno le dice che non avete dato una direzione politica. Io non entro Io non entro sul tema del nucleare (sono a favore); non entro sul tema dei termovalorizzatori (ce ne vogliono almeno cinque in questo Paese, a cominciare da Roma); non entro sul tema del gas e delle trivelle, rispetto al si è convertita sulla via di Damasco. Va bene tutto, ma sulle energie rinnovabili avete fatto un consesso, una riunione di cervelli tra Urso, Lollobrigida e Sangiuliano, che già detta così In questa riunione di cervelli avete partorito dei decreti, il FESR 2, e avete partorito l'agrofotovoltaico e le aree idonee. Grazie a questi decreti, in Italia le rinnovabili non si fanno più e il fotovoltaico diventa un miraggio costosissimo. Avete messo, anche con l'aiuto di altri, un blocco alle rinnovabili. Come fate a dire che vogliamo avere l'energia se per i *data center*, che vogliamo costruire con BlackRock o con altri, ci sarà bisogno almeno di dieci volte l'energia che c'è oggi? Dove la prendiamo l'energia, visto che siamo l'unico Paese

era 40 dieci anni fa, con noi. Certo, ha inciso la guerra, ovvio. Ha inciso il mercato dell'ETS, ma hanno inciso anche le misure del consesso di cervelli Lollobrigida, Sangiuliano, Urso. In Francia il costo è 40, in Germania è 70 e in Italia è 100. C'è qualcosa che non va, ne parliamo? Vogliamo avere una visione, un orizzonte su dove vogliamo portare il Paese? Sulla sanità, avete fatto un decreto sulle liste d'attesa, in piena campagna elettorale. Quando abbiamo convertito il decreto, avete visto che vi siete scordati anche i decreti attuativi. Nel frattempo, nelle stesse ore, il presidente degli Stati Uniti Biden riuniva a New York alcuni *leader* mondiali, ma non c'era la Meloni, così come non c'era all'incontro di Ramstein sull'Ucraina assieme agli inglesi, ai francesi e ai tedeschi, perché la Meloni c'è su Twitter, ma non c'è in questi convegni e in questi incontri internazionali. C'è il grande tavolo per lanciare il progetto di eliminare il cancro, che è la grande battaglia della comunità scientifica internazionale, mentre noi siamo a fare il decreto sulle liste d'attesa, che ci serve a prendere tre voti in più, ma che, paradossalmente, non riduce le liste d'attesa. E potrei continuare, ad esempio, sul tema della sicurezza. Piantedosi è venuto a dirci che nel 2023 i reati sono aumentati, è vero, ma nel 2024 va meglio. È come una partita che perdi tre a zero all'andata, ma al ritorno siamo uno pari alla fine del primo tempo. Mai hai perso tre a zero, hai aumentato i reati, hai creato più insicurezza. Non c'è una parola vera, non c'è una parola di verità sull'immigrazione. L'INPS senza gli immigrati non pagherà le pensioni, ma non avete il coraggio di dirlo, perché scalfisce la vostra prosopopea e la vostra arroganza. Chiamate Elon Musk ad Atreju, lo chiamate all'Atlantic Council, lo chiamate dappertutto, ma non lo chiamate nell'unico posto dove ci sarebbe bisogno: a Cassino, a Mirafiori, a Pomigliano. *(Applausi)*. Se siete tanto amici di Elon Musk, fatelo venire a investire in Italia e fategli portare i posti di lavoro in Italia. No, a voi servono i *tweet* e i *like*, non vi servono i posti di lavoro, perché state raccontando che, grazie a voi, tutto è migliorato. È falso. E le riforme purtroppo, signor Sottosegretario, non ci sono. Non ci sono sulla demografia, non ci sono sulla politica industriale,

per 100 milioni di euro. Gli 80 euro per 10 milioni di famiglie tutti i mesi erano una mancia; il bonus befana *una tantum* a qualche tipo di famiglia è invece una grande misura strutturale. Che poi agli altri porteranno il carbone, perché di sicuro non portano l'eolico e il fotovoltaico, visto che siete riusciti a bloccare anche quelli. *(Applausi)*. Mi fermo, perché la faccio troppo lunga nel merito. Mi limito a una considerazione politica: il mondo in questo momento sta vivendo una stagione incredibile, di problemi enormi. Pensate a quello che succede in Terrasanta, pensate a quello che succede in Africa e in Ucraina. Di fronte a questo quadro, io vorrei raccontarvi banalmente dove erano i nostri *leader* (perché sono anche nostri) la settimana scorsa, il Presidente del Consiglio e i due Vice Presidenti. Un Vice Un Vice Presidente del Consiglio, mentre tutto il mondo ricordava l'anniversario del 7 ottobre e parlava delle questioni internazionali sull'Ucraina, era a Marino,

a cercare la talpa delle *chat*. Voi siete gli aspiranti colpevoli. Chi è stato la talpa infame? Così è definita. Ora, in quest'Aula ha seduto Alessandro Manzoni, che ha scritto la «Storia della colonna infame». Siamo passati dalla «Storia della colonna infame» al futuro della talpa infame, un incrocio tra un *videogame* Signor sottosegretario, io l'ho apprezzata nel suo tentativo di fare la replica. Ma la verità è che la nave è davvero in mano al cuoco di bordo. C'è solo un punto fondamentale, e finisco. Il Parlamento servirebbe per fare le cose meglio: dovreste ascoltare e cercare di cambiare; voi venite e fate i passacarte di quello che vi dà il Governo (lo dico *in primis* ai colleghi della maggioranza). Questo approccio sul Parlamento sapete da cosa si vede? Da quello che avete fatto ieri sulla Corte costituzionale. Quando al Governo c'eravamo noi e litigavamo, ai 5 Stelle è stata data la possibilità, in un momento in cui erano opposizione durissima contro di noi, di esprimere un membro della Corte; alla destra è stata data analoga possibilità. La maggioranza ha scelto nel proprio seno,

le sorprese dicendo in *chat* di non dirlo a nessuno, «così non se ne accorgono e li freghiamo». *(Applausi)*. Imparate a rispettare il Parlamento, solo così rispetterete voi stessi!

in questa proposta che avete avanzato accettate supinamente l'impostazione dell'Unione europea che, a differenza degli anni scorsi,

che ci venderanno le auto a un prezzo accessibile. Sapete tutti, ad esempio, che la Cina è avanti anni luce nel settore e che gli industriali che sono andati lì con la presidente Meloni

e per fare questa cosa è necessario applicare la Costituzione, che dice che chi più ha più deve contribuire. Questa è la cosa che non funziona e rispetto alla

C'è una visione certamente diversa tra la destra e la sinistra su questo tema, fondamentalmente perché c'è una visione diversa sul fatto che

oggi ci sono dieci contratti all'interno della stessa azienda e molto spesso chi ha un rapporto di lavoro più debole magari non riesce a rinnovarlo, quel contratto.

ma questo è il punto fondamentale. È quindi possibile che ci siano 4 milioni di lavoratori che addirittura prendono meno di 9 euro lordi

di centrare maggiormente il tema in discussione in quest'Aula, cioè il Piano strutturale di bilancio di medio termine, che è uno strumento finanziario nuovo,

strutturali), va nella giusta direzione. Le principali finalità del Piano sono quelle di gettare le basi di una programmazione pluriennale della politica di bilancio

di bilancio ci sono scelte sicuramente difficili che il Paese deve fare, ma guardiamoci intorno, guardiamo alle circostanze avverse intorno a noi, agli andamenti dei costi, alle emergenze, alle sfide economiche e produttive, al contesto nazionale e internazionale, alla transizione demografica, all'impatto dei cambiamenti climatici, alla transizione energetica, nonché all'incertezza geopolitica. Mettiamoci tutto questo ed è sicuro che le scelte che il nostro Paese deve fare sono difficili.

dal primo giorno di questo Governo, di questa legislatura e di questa maggioranza di centrodestra, l'approccio è prudenziale rispetto alla finanza pubblica. Ciò però non significa che, proprio perché c'è prudenza, oggi non ci possa essere una spinta riformatrice, che c'è e che,

attuate nel nostro Paese: è un successo importante e una strada tracciata anche sulle riforme. È chiaro che, sul piano strutturale di bilancio, sia importante il controllo della spesa, quindi siamo impegnati su questo. La semplificazione amministrativa è un altro tema importante. Ne abbiamo parlato

è poi la riforma delle riforme, il cavallo di battaglia del nostro partito e del nostro Gruppo, Forza Italia, che è quella fiscale. Noi puntiamo alle tre aliquote, alla riduzione anche delle tasse per il ceto medio (questo è importante), oltre, come dicevo, alla crescita delle imprese.

Bisogna guardare la fotografia del Paese oggi e la realtà di quello che esso è in questo momento particolare. Quasi tutti i Gruppi di opposizione hanno parlato di sanità, che è un tema sicuramente importante e delicato. Questo Governo è impegnato sul fronte, ma ciò non significa che si scivoli verso il privato. Vorrei che qualcuno andasse ad ascoltare gli ultimi interventi fatti da *leader* dell'opposizione, anche dal Governatore pugliese, Michele Emiliano, che invece ha parlato proprio di sanità privata

una battaglia importante, che dovrebbe essere anche delle sinistre e del centrosinistra, invece è diventata nostra e noi renderemo strutturale, nella prossima manovra di bilancio, il cuneo fiscale. Questo significa più soldi nelle tasche dei cittadini e quindi più potere d'acquisto.

Si apre una nuova fase, forse: quella dell'indietro tutta. Ce l'ha ricordato il presidente Monti, richiamando la legge Fornero e facendo riferimento alle tante promesse delle destre,

il nuovo Piano strutturale di bilancio si presenterà come una mannaia nei confronti dei cittadini e delle imprese (lo ha detto chiaramente il ministro Giorgetti), aprendo, sì, una nuova fase, quella degli ultrasacrifici. A questo noi diciamo no, perché non vogliamo sacrifici per tutti. I cittadini e le imprese hanno già pagato in questi due anni di cattiva gestione del Governo Meloni. Noi vorremmo che i sacrifici li facessero gli amichetti di questo Governo: le banche, le aziende farmaceutiche, le industrie delle armi e le assicurazioni, chi ha speculato in questi anni di pandemia, crisi energetica e tassi elevati.

l'*austerity,* con la sottoscrizione del Patto di stabilità, che - lo ricordiamo tutti - era stato definito un buon compromesso, che però costerà agli italiani dai 13 ai 16 miliardi di euro.

Signori miei, l'avanzo primario significa, sì, far stare buoni i mercati alle spalle dei cittadini italiani, ma anche meno spesa pubblica, meno crescita

compressi i salari e la produttività delle imprese e lo Stato sociale ne ha subìto le conseguenze. In Europa serviva un cambio di paradigma e occorreva costruire un'economia europea eco-sociale di mercato al servizio dei cittadini, orientata alla crescita inclusiva e soprattutto alla piena occupazione. Avete invece preferito assecondare un'economia ancora schiava della finanza, dei grandi capitali, del mercato finanziario e della speculazione. È bene ricordare che l'*austerity* non tutela i cittadini e le imprese, ma garantisce solo i grandi capitali dall'inflazione. Attenzione, ormai la dottrina e gli studi scientifici dimostrano che per contrastare l'inflazione possiamo avere due strade: tagliare la domanda aggregata (sacrificando però i salari, la produttività e la crescita economica) oppure agire sull'offerta, così com'è stato fatto nel corso del Governo Conte II, quando abbiamo sostenuto gli investimenti, l'innovazione, la produttività, il lavoro e lo Stato sociale. Non ci può essere crescita economica senza sicurezza sociale. Oggi infliggete l'ennesima stangata agli italiani, di 13 e 16 miliardi, perché, oltre ai 9 miliardi derivanti dalla differenza tra *deficit* programmatico e tendenziale, il resto deriverà da tasse e tagli. In questo piano strutturale c'è un virus, un virus, quello del calo della spesa reale, perché c'è un vincolo che è un elemento agghiacciante: la spesa primaria netta, che non potrà aumentare in media oltre l'1,5 Questo produrrà una riduzione della spesa reale di 13 miliardi l'anno per i prossimi sette anni: questo dovete dire agli italiani.

Piano che rappresenta una vera e propria dieta. Forse in questo caso dobbiamo dare ascolto al ministro Giorgetti, che una cosa l'ha azzeccata, parlando di "sacrifici" *(Applausi)*, perché ci attendono anni di veri sacrifici.

a fronte adesso di uno zero virgola, addirittura rettificato recentemente anche dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

risorse che avete disponibili all'interno del PNRR. Siete riusciti a spenderne, sì e no, il 20 per cento. Oggi quella crescita dello zero virgola si basa non sulle vostre riforme, che hanno un impatto pari allo zero, ma semplicemente sul PNRR del presidente Conte *(Applausi)*, che abbiamo portato nel corso del Governo Conte II. Siamo fortemente preoccupati preoccupati per la situazione denunciata dagli enti locali, visto che, oltre al miliardo che avete già tagliato nella scorsa legge di bilancio, adesso annunciate altri tagli. Siamo preoccupati per la produzione industriale, in calo da oltre

e aumenta anche grazie alla precarietà che avete sostenuto, grazie ai salari poveri, perché non adeguate i salari e non introducete quello minimo.

Dicevo che siamo preoccupati anche per la pressione fiscale. La vostra bandiera l'avete ormai ammainata, perché la pressione fiscale - lo dice l'Istat

Vado alle conclusioni, signor Presidente. Avete introdotto un concordato preventivo biennale che negli auspici era anche condivisibile, quello di creare un nuovo rapporto collaborativo tra contribuenti e fisco. Vi sono state tre modifiche in meno di sei mesi,

la riduzione dei redditi reali del ceto medio e lo smantellamento dello Stato sociale. Altro che prudenza e responsabilità, qui stiamo andando verso il baratro (si parlava di rilancio). A questo punto forse, ritornando indietro (così come ho iniziato), la professoressa Elsa Fornero, di fronte al baratro di quegli anni, ha avuto almeno la decenza di chiedere scusa agli italiani e di piangere.

stupiti, facendo riferimento ad una citazione di Keynes: la difficoltà - diceva Keynes, citato da Giorgetti - non risiede nelle idee nuove, ma nello sfuggire a quelle vecchie. in queste ore mi sono chiesto: avanzo primario, tagli alla spesa pubblica, aumento delle tasse, l'idea di uno Stato minimo, per non parlare delle privatizzazioni, del lavoro povero, cosa c'è di nuovo in queste ricette delle destre contenute in questo Piano? Non c'è nulla. Rivolgo quindi un invito al ministro Giorgetti: forse dovrebbe sostituire i suoi occhiali, che guardano al passato, mentre avrebbe bisogno di un nuovo paio di occhiali, che guardano al futuro. Gramellini: le scelte bisogna farle con coraggio e non per paura. Ieri il ministro Giorgetti ci ha trasmesso paura. *(Applausi)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, inizio citando il ministro Giorgetti, che ha detto: questo Ministro fa il contrario di quello che fanno altri Ministri, che gonfiano la crescita per spendere risorse che non ci sono. È un approccio pragmatico e rivoluzionario, nella sua normalità. Spieghiamo perché è rivoluzionario nella sua normalità, facendo alcune riflessioni sulla spesa pubblica, sulle entrate e sugli interessi in relazione al Piano presentato.

considerando l'inflazione, sostanzialmente zero *budget*, tieni la spesa fissa. Il Piano recepisce la regola: la media della spesa nei prossimi sette anni è appunto l'uno e mezzo.

ovviamente ciò vuol dire che tutto il resto crescerà meno. Però su questo torniamo. Sulla sanità faccio due considerazioni che ci sembrano importanti, una di carattere politico e l'altra sui numeri. La prima, di carattere politico, è positiva: finalmente tutto il Parlamento, ma anche i *media*, hanno cambiato il *mood* sulla sanità. Il clima è cambiato, adesso sono tutti d'accordo sul fatto che bisogna investire in sanità. Ci ricordiamo bene gli anni dal 2012 in poi, quando la sanità era fonte di spreco, bisognava tagliare ed erano tutti d'accordo.

sono passati dal 6,9 al 6,2-6,3 del PIL. Quindi il grosso dei tagli alla sanità è stato fatto in quegli anni e in quel clima, dove a difendere la sanità c'eravamo noi, ma invece bisognava tagliarla e tutti erano d'accordo sul tagliarla. Guardiamo positivamente al fatto che c'è stato questo ravvedimento operoso e che adesso bisogna investire in sanità. della normale razionalità e rivoluzionario perché normale ha investito 5,2 miliardi in sanità; quindi solo l'anno scorso c'è stato un salto del 4

Dicevamo però che se alcune componenti crescono più dell'1,5 per cento, le altre necessariamente dovranno fare uno sforzo. È in questa ottica che vanno lette le dichiarazioni del ministro Giorgetti che afferma che le amministrazioni dovranno fare un sacrificio. È chiaro. Le amministrazioni in questo caso sono i Ministeri. È chiaro che se alcune componenti, in particolare la sanità, è attenzionata e cresce di più, gli altri dovranno fare un sacrificio. È però giusto così,

senza citare, per carità di patria, l'azienda ospedaliera. Un'azienda ospedaliera compra un robot di quelli per operare in maniera meccanica,

Ecco, questa non è proprio spesa di qualità. Quindi non solo quantità, ma qualità. È un tema che sarà sempre più necessario; proprio perché si va verso un periodo di zero *budget*, sarà sempre più necessario guardare alla qualità della spesa invece che alla quantità. Veniamo alle entrate.

per l'allargamento della base imponibile; mezzo milione di lavoratori in più dopo il taglio del reddito di cittadinanza *(Applausi)*, significa Irpef e contributi. È normale e rivoluzionario nella sua normalità, non ci voleva uno scienziato per capirlo. L'altro dato importante è la riduzione del *tax gap*, la

del *tax gap*, dell'evasione fiscale. In questa ottica il tanto criticato, secondo me totalmente ingiustamente, concordato preventivo è retroattivo, perché è un concordato che guarda sia avanti che indietro, e va esattamente e per definizione nell'ottica della riduzione del *tax gap*. Per aderire infatti sia al concordato retroattivo che preventivo devi semplicemente dichiarare un fatturato maggiore e quindi si riduce il *tax gap*. tal proposito la saggia prudenza del Governo prevede per questa misura zero euro di entrate. È giusto così: meglio spendere le entrate quando ci sono davvero, altrimenti succede quello che accade spesso. Andate a vedere le relazioni della Corte dei conti di Comuni in particolare stato di difficoltà, di dissesto o predissesto. Succede che si prevede 100 di entrate, entra 50, però la spesa viene prevista per 100; ma se è entrato solo 50 e fai spesa per 100, vai in dissesto. È così facile. Bene quindi essere prudenti anche nella stima delle entrate. Al riguardo faccio due esempi;

perché le barche stanno nel mare e, giustamente, nel mare ci si sposta e si sono spostate altrove. Attenzione alla patrimoniale, perché anche i capitali stanno nel mare della finanza e si spostano molto velocemente, anche più delle barche. il catasto, nessuna revisione delle rendite catastali: questo è quello che vuole la sinistra. Qui non c'è alcuna revisione delle rendite catastali, ma una normale e giusta manutenzione. Se un immobile non è accatastato, ma esiste (basta guardare su Google Maps), è giusto inserirlo nell'archivio. Se un immobile non è accatastato ma ha un'utenza della luce, del gas, magari anche di Dazn, è giusto inserirlo nell'elenco.

anche dello *spread*, perché adesso non è più l'Italia a essere il malato d'Europa, ma sono altri i malati d'Europa, vedi la Francia con il *deficit* commerciale, vedi la Germania con un modello industriale in difficoltà. è proprio la rivoluzionaria normalità del ministro Giorgetti e del Governo Meloni che garantisce questo *spread* basso, che garantisce, con credibilità, la tenuta sotto controllo dello *spread*, e poi la stabilità politica è un vantaggio competitivo del nostro sistema Paese. Buon lavoro, quindi, al Governo della rivoluzionaria normalità. Signora Presidente, in tanti, anche in quest'Aula, hanno ricordato quanto sia importante il Piano strutturale di bilancio nelle nuove regole europee noi, Sottosegretario, ci aspettavamo dal Governo un documento all'altezza di questa importanza, con una visione magari non condivisibile, ma con una prospettiva, impegni precisi sulle riforme e sugli investimenti da fare nei prossimi anni e magari anche un confronto con le parti sociali, con gli enti territoriali, un confronto meno frettoloso di quello che c'è stato. Siamo stati ingenui, ancora una volta, perché quello che abbiamo ricevuto dal Governo è molto diverso; è - lasciatemelo dire - un capolavoro all'incontrario, perché il Governo ci ha presentato un documento di 217 pagine assolutamente lacunoso e generico. Andate a vedere le audizioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Banca d'Italia e della Corte dei conti: mancano dati, mancano informazioni che noi chiediamo al Governo di integrare. Duecentodiciassette pagine che avete esaminato in una frettolosa riunione con le forze economiche e sociali, in una altrettanto frettolosa sessione di discussione parlamentare. Presidente, il ministro Giorgetti, ieri in audizione, ha definito questo Piano ambizioso e realistico. Mi dispiace per il Ministro, perché questo è un Piano che non è ambizioso e tantomeno è realistico, è un piano debole, e lo è innanzitutto sul versante delle riforme, perché è una fiera delle buone intenzioni per le riforme che servono. Dite che migliorerete l'efficienza della pubblica amministrazione e ridurrete i tempi della giustizia,

che, purtroppo, conferma le riforme sbagliate: conferma una riforma fiscale fallimentare, che non rilancerà la crescita e aggraverà le disuguaglianze in questo Paese, e conferma l'autonomia differenziata, che è una sciagura innanzitutto per le imprese. Andate a chiedere agli imprenditori se la loro vita migliora o peggiora con 21 leggi regionali sul commercio estero, 21 leggi regionali sulle grandi infrastrutture, 21 leggi regionali sulle reti energetiche o sulla Protezione civile. *(Applausi)*. Altro che semplificazioni! È un piano debole sugli investimenti. Mario Draghi - si può essere d'accordo o meno sulle sue proposte - ha pubblicato un rapporto che ha evidenziato in modo crudo i ritardi dell'Europa e dell'Italia e ha detto che, se l'Europa vuole fare davvero la transizione ecologica e digitale, deve investire ogni anno 800 miliardi di euro in più. L'Italia fa parte dell'Europa e quegli 800 miliardi vorrebbero dire per il nostro Paese 100 miliardi di euro in più tra investimenti pubblici e privati. Sfido il Sottosegretario, che è così pronto a citare le pagine del piano, a trovare un solo riferimento alle riflessioni europee, a come tradurle nel nostro Paese. Altro che investimenti pubblici e altro che investimenti privati. È un piano che non ha una strategia per la crescita e non ha una politica industriale, come infatti i numeri certificano. Signor Sottosegretario, se andiamo a vedere i vostri numeri e le vostre tabelle, vedremo che dal 2025 al 2029 le vostre previsioni sulla crescita italiana sono sempre sistematicamente inferiori a quelle del resto d'Europa. Questo piano certifica il declino del nostro Paese, non la crescita, la crescita, e porterà ad un aumento delle disuguaglianze! Il mio collega Garavaglia ha parlato tanto di sanità; signora Presidente, invito il collega Garavaglia a riguardarsi i dati: dal 2013 al 2022 la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL non è mai scesa al di sotto del 6,4

che tra il 2022 e il 2023 la spesa privata delle famiglie italiane, cioè i soldi che le famiglie devono mettere di tasca propria per pagarsi le visite e gli esami, è cresciuta di 3,8 miliardi. Questa cifra è equivalente alla grande riforma Irpef che ci avete tanto sbandierato. La vostra riforma Irpef se l'è mangiata la privatizzazione strisciante del sistema sanitario che voi state portando avanti con il sottofinanziamento. Signora Presidente, se vogliamo parlare di tasse, cari colleghi della destra,

senza mettere un euro in più sul trasporto pubblico! Voi farete costare di più gli spostamenti per le famiglie normali, senza potenziare il trasporto pubblico, senza rifinanziare il *bonus* trasporti, senza offrire un'alternativa alle famiglie normali. Siete andati avanti, perché avete parlato di tassazione in più delle imprese e confesso che nessuno di noi ci ha capito niente: se volete tassare i profitti, gli extraprofitti, i sottoprofitti; quello che è certo è che darete una stangata, proseguirete a stangare le imprese manifatturiere che producono, che esportano, che tengono su l'economia italiana, come avete fatto con la riforma fiscale. L'unica misura permanente in quella riforma è l'eliminazione dell'aiuto alla crescita economica (ACE) e tre miliardi di euro di tasse in più sulle imprese italiane. Andate avanti così, altro che politiche industriali e altro che politiche per la crescita. Signora Presidente, è un piano assolutamente fragile e scritto sulla sabbia per i presupposti su cui si basa. C'è un articolo interessante di Massimo Bordignon su «Lavoce.info» che vi invito a andare a leggere e che dice delle cose interessanti. Voi, in questo piano, volete mantenere stabile il livello degli investimenti pubblici, anche quando non arriveranno più i soldi dall'Europa, perché sarà finito il PNRR; sulla sanità, volete tenerla stabile in rapporto al PIL; dite di voler ridurre la pressione fiscale, il cuneo o l'Irpef. Non fate nulla contro l'evasione fiscale. Ho sentito il collega Dario Damiani: altro che condoni, parola arcaica. Avete fatto, pochi giorni fa, l'ennesima sanatoria sul concordato preventivo biennale: uno schiaffo, non solo ai dipendenti e ai pensionati, ma agli autonomi che fanno il loro dovere nei confronti del fisco. *(Applausi)*. Questo è il vostro concordato e il vostro ennesimo condono. Non lottate contro l'evasione. Vi viene l'orticaria anche quando il vostro Ministro parla di rendite catastali o di sacrifici. Ma allora da dove vengono fuori i soldi che servono per finanziare questo piano? Alcune cose state iniziando a dirle: le tasse. Vedremo quante nuove tasse arriveranno nei prossimi giorni. L'altra cosa non detta la spesa sociale, perché voi sulla sanità avete detto qualcosa, ma non avete detto assolutamente nulla sulla spesa previdenziale, sulla spesa per il *welfare*, sui soldi che servirebbero per finanziare la riforma dell'assistenza agli anziani. Su tutto questo si prospettano tagli e li vedremo a partire dalla prossima legge di bilancio. C'è un ultimo punto che incrina la credibilità di questo Piano ed è il PNRR. Voi incorporate l'ipotesi che sia completamente attuato entro il 2026. l'Ufficio parlamentare di bilancio ha dato dei numeri terribili: voi avete speso nove miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno, sui quarantaquattro che avevate programmato. Ho fatto i conti: con questo ritmo, il Piano lo completerete nel 2036, non nel 2026. *(Applausi)*. È chiaro che, con questi presupposti, il Piano è scritto sulla sabbia e che le scarse previsioni di crescita rischiano di condurci verso la stagnazione. Doveva essere un nuovo PNRR, questa era l'ambizione che ci aspettavamo dal Governo; invece, abbiamo avuto una lettera di Natale con tante promesse sulle riforme: faremo, forse; finanzieremo, chissà quando; nessun progetto concreto per fare ripartire il Paese, quando il PNRR, che noi abbiamo ottenuto in Europa, non ci sarà più e sarà vostra responsabilità indicare una prospettiva di crescita, di coesione sociale e di sostenibilità ambientale, che è totalmente assente da questo documento. Il vostro Piano è un'occasione persa, non è quello che serve all'Italia ed è la conferma dell'inadeguatezza di questo Governo. noi stiamo per votare il primo piano strutturale di bilancio di medio termine, alla luce di quelle che sono le regole date dalla nuova *governance* economica europea. europea. Questo dibattito, onorevoli senatori, è un po' surreale. e vi spiego perché. Sembra quasi che non ci foste anche voi, insieme a noi, a portare avanti quel negoziato complicato, difficile,

Forse lo ricorderete anche voi, come il nostro Ministro, alla luce di quelle che sono state le risoluzioni, approvate peraltro all'unanimità dai senatori nella Commissione bilancio, per cercare di ottenere maggiori spazi di manovra di bilancio. Ebbene, quel negoziato è andato come è andato. Voi sapete bene che l'Italia e molte altre nazioni non hanno votato favorevolmente. Ma tant'è: queste sono le regole che ci sono state imposte. Noi cercheremo quindi di portarle avanti nel miglior modo possibile per il benessere dell'Italia e del popolo italiano.

Solo in Italia noi abbiamo 700.000 pensionati a fronte di 379.000 nati. Pertanto, mi chiedo e vi chiedo: non sarebbe utile scomputare le spese per rilanciare il tasso di natalità e la demografia in Italia e in Europa? Assolutamente sì. In questo scenario, in cui abbiamo intenzione di continuare la nostra azione pervicace e consistente nei riguardi dell'Unione europea, andiamo comunque a varare un piano con una previsione del *deficit* tendenziale in rapporto al PIL, pari al 3,8 per cento l'anno, in netta riduzione rispetto al dato consuntivo del 2023.

Il *deficit* è stimato in riduzione e il tasso di crescita medio è stimato all'1,5 per cento nel periodo di aggiustamento tra il 2025 e e il 2031. Gli obiettivi di *deficit*, coerentemente con la traiettoria programmatica di spesa netta, corrisponderanno a un andamento migliorativo del saldo primario. Questi dati sono certificati da tutti gli organismi, tra cui l'UPB.

innanzitutto sulla famiglia, perché è assolutamente fondamentale sostenerla, sull'impresa, visto che peraltro ha un calo produttivo, assolutamente sì,

Io parlo quando stanno zitti gli altri, perché è un fatto di educazione.

sono i dati. Continueremo con le nostre politiche, per esempio, per implementare il piano Mattei e sostenere i rapporti con un'Africa che ci sta dando risultati straordinari, anche in termini di flussi migratori, così come sulle geopolitiche, geopolitiche, appunto, per quanto concerne la piattaforma italiana che è nel Mediterraneo, che stiamo cercando di ottimizzare in ogni modo e che sta portando a trasformare l'Italia in un grandissimo *hub* energetico, utile per l'Italia, ma direi utile per l'Europa tutta. quindi che questo Piano va a fotografare una situazione sicuramente non semplice. La sfida che ci si è presentata è complessa, perché ci impone e impone a tutti di riuscire a conciliare ciò che sembra difficilmente conciliabile. La sfida è quella di conciliare una prudente gestione della finanza pubblica con la crescita economica. Io credo, signori, che le sfide vadano accettate. Comunico che sulla proposta di risoluzione n. 6, accettata dal Governo, sono stati presentati alcuni emendamenti, i cui testi sono in distribuzione,

dal senatore Misiani in dichiarazione di voto, la risoluzione n. 6 è tecnicamente inemendabile, altrimenti con i Gruppi di opposizione avremmo provato a lavorare per un insieme di emendamenti che avrebbero potuto migliorare il testo. Però, signora Presidente, ci tenevamo a sottoporre all'attenzione delle colleghe e dei colleghi di maggioranza due emendamenti alla risoluzione n. 6: il primo riprende l'ultimo passaggio della dichiarazione di voto finale del senatore Misiani sulla sanità, perché vi invitiamo a sostenere la spesa sanitaria, incrementando il livello della spesa stessa, arrivando in un quinquennio ad una percentuale sul PIL non inferiore al 7,5, allineandola, signora Presidente, alla media europea. È evidente il nostro obiettivo: l'aumento degli stipendi per le diverse categorie; i finanziamenti dei servizi di prossimità, case e ospedali di comunità, centrali operative territoriali, completamente dimenticati dal Piano strutturale di bilancio e un'indicazione chiara nello stesso Piano degli investimenti in prevenzione, a partire dai consultori salute mentale e il benessere psicologico. Tutto questo, signora Presidente, perché nel Piano strutturale di bilancio, presidente Zaffini, è successo anche questo (immagino che nella foga di approvare il parere, la maggioranza non se ne sia accorta): avete dimenticato i divari territoriali legati proprio alla vostra politica sanitaria, che resta bloccata sul 6,3 di PIL, che è il livello più basso degli ultimi dodici anni.

le seguenti:* "con esclusione, nell'ambito del riordino delle spese fiscali, dell'allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina, al fine di neutralizzare» - e sottolineo «neutralizzare» - «l'impatto degli aumenti sull'autotrasporto, sul trasporto pubblico locale, sui lavori pubblici e sul comparto agricolo». Colleghe e colleghi della maggioranza, diteci

il noto messaggio che l'attuale Presidente del Consiglio, all'epoca *leader* di Fratelli d'Italia, affidò ai *social* nel 2019, quando la benzina costava un 1,576 euro e il gasolio 1,471 euro, e aveva promesso di intervenire sulle accise.

la Presidente del Consiglio, quando si è insediata a Palazzo Chigi, aveva la benzina che costava 1,678 euro.

benzina a settembre 2024: 1,755 euro; il gasolio: 1,632 euro. Chiediamo, signora Presidente, che l'allineamento, l'allineamento, che è a pagina 116, non produca un impatto sulle accise e che quell'impatto venga neutralizzato. Altrimenti sarà inevitabile per noi definirla, in questa legge di bilancio, una tassa aggiuntiva Meloni. *(Applausi)*.

e che ha imposto non solo all'Italia, ma a tutti i Paesi, di togliere le agevolazioni sul diesel. Sì, è proprio così, collega Boccia: chiedete ai vostri amici a Bruxelles di togliere questo allineamento.

voi avete presentato un piano strutturale di bilancio che non contiene delle cose chiare sul tema della sanità. E, quindi, noi vi proponiamo nell'emendamento una cosa semplice: riaprire il tema del del MES, perché, se volete investire sulla questione del MES, avete l'opportunità di dare un contributo sul tema delle liste d'attesa e della sanità. Nel vostro Piano non compare la parola «giovani». Giovani significa residenze per gli universitari e rientro dei cervelli.

chiaro e solenne a non aumentare la pressione fiscale in questo Paese. Siete disponibili a votarlo oppure continuate a immaginare che possa esserci un aumento delle tasse, soprattutto sulla casa, come ieri il ministro Giorgetti ha fatto intendere a tutti noi? Questi sono i fatti, la polemica sta a zero. Se volete prendervi un impegno, qui ci sono le opportunità per farlo. Altrimenti fate come sempre: con una mano provate a raccontare agli italiani dei complotti e con l'altra invece li tassate.

renziana che abbiamo imparato a conoscere, hanno messo cose condivisibili, come il finanziamento del Sistema sanitario nazionale, insieme al divieto di tassare gli extraprofitti dei colossi e

il DEF approvato nell'aprile 2022 prevedeva, per l'anno corrente e per l'anno prossimo, un totale di 11 miliardi in meno di quanto l'attuale Governo ha già approvato in legge di bilancio.

Senatrice Malpezzi, la prego di lasciar concludere il senatore Malan. Potrà intervenire in dichiarazione di voto, se vuole. MALAN Capisco che disturba sentire ricordare questo. *(Applausi)*.Ricordo che chi faceva parte di quella coalizione oggi ha votato un aumento di 11 miliardi.

ricordo che, sempre negli anni precedenti, la benzina aveva già superato il prezzo medio, non il prezzo fotografato nella stazione di montagna, in situazioni disperate e disagiate… *(Commenti)*. PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, la prego. Mentre oggi, come ha detto il presidente Boccia, il prezzo medio è 1,75, 1,65, il prezzo aveva già superato i 2 euro e ci sono stati due anni di inflazione, sia pure moderata. chi fa il maestro forse ha meno titoli dei presunti allievi, che saremmo noi. Noi stiamo facendo le cose che sono possibili alla luce anche del fatto che, con 20 miliardi all'anno di peso del superbonus indubbiamente si hanno meno risorse di quelle che ci si sarebbe augurati, che si potrebbero mettere nella riduzione delle accise o nell'aumento delle risorse per la sanità. Nonostante questo, sono aumentate le risorse per la sanità, la benzina è a prezzi molto più bassi di quanto lo sia stata anche solo nel 2022 e noi siamo certi di

bilancio, distinguono in modo molto chiaro i livelli dalle percentuali. Non è un caso che nell'intervento che ho appena sentito si insiste su 11 miliardi. Nella pagina che la Corte dei conti dedica alla sanità si dice che, secondo questo Piano, alla fine del periodo ci saranno 10 miliardi in meno per la sanità. L'UPB calcola che, per avere lo stesso livello di sanità in rapporto al PIL del 2019, ci vogliono almeno sette miliardi in più.

ma alla fine questi sono i risultati: ci sono meno risorse e una minore percentuale - probabilmente la più bassa - a livello europeo. Sul petrolio la Banca d'Italia e l'UPB fanno notare come le previsioni, che sono contenute a livello del prezzo al barile, in questo Piano fanno riferimento ad un'aspettativa che arriva addirittura a 69 dollari per barile, quando nell'ultimo anno sono stati tra i 90 e i 100 dollari. La Banca d'Italia dice che dal loro punto di vista è un po' ottimistico, senza considerare tra l'altro le spinte inflattive. Sulla questione del prezzo medio vi ha risposto l'Antitrust, affermando che le misure che avete fatto non sono significative. Detto questo, la questione principale riguarda il fatto che tutti gli enti indipendenti che abbiamo ascoltato ci hanno ripetuto una storia diversa, compresa quella sottolineata dalla senatrice Mennuni sull'incremento del lavoro che esiste effettivamente e parte dal 2020, ma che è dall'altra parte è dall'altra parte controbilanciato da una riduzione sostanziale documentata dall'UPB delle ore lavorate e da una riduzione dei salari che sono pure incrementati, ma che a livello medio restano significativamente inferiori alla media europea.

visto al battesimo di questo nuovo Governo, alla prima legge di bilancio dove, con il favore delle tenebre, ha tolto lo sconto sulle accise, permettendo a tali idrocarburi di

che è stato classificato uno dei più gravi disastri ambientali della storia provocati dall'uomo. Erano le ore 22,39 di quel giorno a Longarone e nei paesi limitrofi dormivano, guardavano la TV, la partita di calcio o cose simili - quando un'enorme frana si staccò dal monte Toc, precipitando nel bacino alpino formato dalla diga. Nel cadere nell'invaso, quella frana sollevò un'onda che scavalcò la diga, finendo poi nel fondovalle. In pochi minuti interi paesi vennero spazzati via. In pochi minuti sparì un intero territorio. Persero la vita troppe persone: quasi 2.000. Fu una tragedia immane, che non abbiamo mai dimenticato e che è corretto ricordare. Certo, questa tragedia avvenne anche e soprattutto per gravi responsabilità umane. Assicurare una cornice di sicurezza ai cittadini significa saper apprendere la lezione che la natura ha voluto anche in quella occasione insegnarci. Assicurare una cornice di sicurezza ai cittadini significa saper fare passi avanti. Oggi, a distanza di tanti anni, con il dolore che si rinnova, chiedo a quest'Aula qualche attimo di silenzio in memoria della tragedia del Vajont.

come lei ben ricordava all'inizio di questa seduta, è una tragedia immane che non possiamo dimenticare. La sera del 9 ottobre di sessantuno una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia si staccò dal monte Toc e precipitò nel bacino artificiale della diga del Vajont, tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, provocando un'onda di distruzione e morte che spazzò

Un disastro, una tragedia, che ci ricorda che il dolore non sbiadisce, anche a distanza di tanti anni. Questo ci ricorda - ed è importante farlo in quest'Aula - quanto sia essenziale proteggere il nostro territorio e agire con responsabilità per permettere che tragedie simili non accadano mai più. Una tragedia annunciata, che forse, appunto, poteva essere evitata, ma che oggi è giusto ricordare. E io lo vorrei fare anche attraverso alcune

cascano nel lago dietro alla diga e sollevano un'onda di 50 milioni di metri cubi. Solo la metà scavalca di là della diga, solo 25 milioni di metri cubi d'acqua Ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra cinque paesi: Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, Faè».

sopravvissuti. Voglio dire, anche qui in quest'Aula, un grazie a questo straordinario scrittore, interprete e attore, perché ha portato al grande pubblico, ha fatto conoscere al grande pubblico la tragedia immane di quel popolo, di quegli abitanti, in quelle terre che sono state così toccate, ma che poi è una tragedia nazionale.

«Non esiste più niente della vita di un tempo. Tutte le civiltà scomparse sono state cancellate in qualche anno. La nostra in due minuti. Ci siamo ritrovati il giorno dopo a partire da zero, in altri luoghi, in altri modi, con altri tempi, usando cose che non conoscevamo. È stato come nascere un'altra volta. Nascere vecchi è come vivere morti. Non ci si adatta a ciò che non si conosce.». E soprattutto vorrei esprimere, anche a nome del mio Gruppo Italia Viva, vicinanza e solidarietà a quelle popolazioni, alla mia Regione, il Veneto, e anche all'Emilia-Romagna e alle tante altre Regioni che anche in questi giorni, come nelle settimane scorse, sono state colpite, ancora una volta, da alluvioni e hanno vissuto momenti difficili a causa del maltempo. Concludo ricordando a questo Governo, grazie alla presenza del Vice Ministro, che forse rimettere in piedi una struttura come Italia Sicura potrebbe essere un aiuto importante per andare nella direzione della prevenzione del nostro territorio. Signor Presidente, come lei ha ricordato, sono passati sessantun'anni da quella terribile sera del 1963. Impossibile dimenticare quello che accadde alle ore 22,43 del 9 ottobre. Dal monte Toc, dietro la diga del Vajont (la diga a doppia curvatura più alta del mondo), si staccano, tutti insieme, 260 milioni di metri cubi di roccia che cadono nel lago artificiale e sollevano un'onda gigantesca che, precipitando a valle, spazza via il paese di Longarone e devasta Castellavazzo, Erto e Casso, facendo 2.000 vittime (1.913, dicono le cifre ufficiali): un disastro gigantesco, ma non certo una fatalità, piuttosto una tragica conseguenza di precise responsabilità umane e della devastazione di un territorio stravolto nel suo assetto naturale e sociale. Eppure da tre anni la montagna mandava segnali e gli abitanti, conoscendo bene i luoghi, avevano manifestato preoccupazione. Gli esperti avevano fatto sopralluoghi e indagini e lanciato allarmi. Come sapete, una giornalista coraggiosa come Tina Merlin aveva denunciato i pericoli che si nascondevano dietro il progetto della SADE. Tutti sapevano, nessuno si mosse: questo scrisse subito dopo la tragedia. Nessuno si mosse perché gli interessi industriali e finanziari ebbero la meglio. Anche lo Stato abdicò alle sue funzioni di controllo e salvaguardia del territorio e delle popolazioni. Tina Merlin - come sapete - venne addirittura denunciata per aver turbato l'ordine pubblico. Solo undici anni fa, in occasione del cinquantesimo anniversario, le più alte cariche delle nostre istituzioni si sono scusate e inchinate per quello che accadde, per le omissioni, i silenzi e le responsabilità. Nel 2008 le Nazioni Unite hanno considerato il Vajont come il primo tra i più grandi disastri

riflettere sul fatto che, se vogliamo dare un senso attuale e non retorico alla memoria, e se vogliamo davvero rispettare quelle vittime e il dolore immane dei sopravvissuti, dobbiamo fare della tutela del territorio, della messa in sicurezza della montagna, della difesa del suolo e della sicurezza idrogeologica una vera e propria priorità nazionale, perché oggi non è purtroppo ancora così. Troppo spesso l'azione dell'uomo, invece di preservare il territorio, lo sottomette a logiche e interessi particolari, con conseguenze pesanti in termini ambientali e anche produttivi. La nuova recente alluvione in Emilia-Romagna, così come un'altra tragedia che il Veneto non dimentica, quella della Marmolada, sono lì a ribadire quanto la tutela del territorio, la difesa del suolo e la sicurezza idrogeologica siano una vera e propria emergenza La prevenzione è la sfida principale. Abbiamo bisogno di una grande opera di riassetto del territorio, di infrastrutture ambientali che lo mettano in sicurezza e di interventi di prevenzione legata ai rischi naturali. Troppe volte, anche in Italia, è successo che si siano commessi errori già compiuti in passato. Davvero non deve più accadere. Abbiamo il dovere di ricordare e in questo senso è stata giusta la scelta di riportare a Belluno la sede dell'archivio processuale. In conclusione, signor Presidente, faccio tesoro ancora una volta delle parole pronunciate dal presidente Mattarella proprio l'anno scorso in quei luoghi, quando disse che «occuparsi dell'ambiente, rispettarlo, è garanzia di vita». Presidente, colleghi, oggi si ricorda purtroppo una tragedia, quella del Vajont, di cui ricorre il 61° anniversario. Ognuno di noi ha il dovere di ricordare e di raccontare quel 9 ottobre del 1963 per onorare le vittime e far sì che una catastrofe, come quella avvenuta a causa del crollo della diga del Vajont, non si ripeta più. Da quel giorno, dal 9 ottobre, tanti territori portano una profonda e insanabile ferita, da Longarone a Rivalta, da Pirago a Villanova, Faè, Erto, Casso e Castellavazzo: intere comunità scosse dalla tragedia, a cui esprimiamo ancora una volta la nostra totale e piena vicinanza. Il nostro pensiero oggi è rivolto alle 1.910 vittime, che devono essere ricordate con profondo rispetto e in maniera solenne: vite strappate via dalle proprie famiglie, dai propri amici e dalle proprie comunità; tra loro 487 bambini e giovani vite che si erano appena affacciate al mondo; la più piccola, Claudia Martinelli, aveva soltanto ventuno giorni. Dobbiamo riflettere tutti sul ruolo della memoria. Ricordare significa portare rispetto, tenere vivo il ricordo di chi oggi non c'è più, ma anche rievocare le gesta di chi, fin dai primi momenti successivi alla tragedia, si è recato a prestare soccorso alle popolazioni colpite. Un commosso pensiero è rivolto anche a tutti i loro. L'attenzione verso il prossimo e la forte solidarietà che è stata dimostrata in quella circostanza sono stati uno degli insegnamenti della tragedia del Vajont. Quella terra ha spesso saputo rialzare la testa, grazie al valore della solidarietà, e ha saputo reagire con forza di fronte alle difficoltà. La memoria esigente deve esserlo. Non possiamo limitarci a ricordare con le parole. Ricordare, quindi, significa impegnarsi per la continua ricerca della verità e impegnarsi per saper ricostruire il Vajont, tragedia determinata dalla cattiva coscienza dell'uomo e diventato un punto fermo da cui ripartire; un impegno per le istituzioni a portare avanti la difesa dell'ambiente, una giustizia efficace e un'adeguata formazione per le prossime generazioni. Il Vajont ci ha insegnato cosa vuol dire essere comunità, un valore da portare avanti giorno per giorno, ricordando il passato e il sacrificio di chi non c'è più e allo stesso tempo guardando con fiducia al domani, con la consapevolezza di quanto gli errori umani commessi nel passato debbano spronarci a realizzare una società nuova, ancor più solidale e giusta, in cui la sostenibilità ambientale prevalga sulle logiche del profitto. Sarà questo il vero orizzonte al quale guardare per le prossime generazioni.

Signor Presidente, lei per primo e poi gli altri che sono intervenuti prima di me hanno già abbondantemente descritto gli eventi di quel 9 ottobre 1963, per cui non mi ripeterò. Il senatore De Poli poco fa ha affermato giustamente che bisogna fare tesoro delle esperienze del passato e allora cerchiamo di capire cosa è successo allora con gli occhi di chi visita adesso quei luoghi. Provate ad andare a Longarone e a risalire la la chiusa del Vajont sotto quella diga imponente che è ancora lì e che è veramente impressionante vista da sotto. Poi, arrivati a livello della diga, dove dovrebbe esserci il lago vedete una serie di colline colline boscate, perché nel frattempo è cresciuto il bosco, però si vedono ancora tutt'intorno i confini di quello che doveva essere l'alveo. Poi si va avanti lungo la strada che porta a Erto, fino al passo Sant'Osvaldo, la vecchia strada che collegava valli tra le più povere delle Alpi, ossia la valle del Vajont, la val Cimoliana, le cui popolazioni per secoli hanno combattuto per sopravvivere nei modi che allora erano consentiti dall'agricoltura di sussistenza. nell'immediato Dopoguerra succede quello che è successo un po' in tutte le Alpi, cioè accade che ci sono persone e imprenditori con una certa visione che, in assenza di regole, trovano i quattrini necessari e decidono di fare grossi investimenti sul territorio; lo hanno fatto per i comprensori sciistici, realizzando degli impianti di risalita e spianando delle piste, e lo hanno fatto con gli impianti di produzione idroelettrica: venivano scelti dei luoghi dove c'erano delle valli chiuse, si faceva la diga e si faceva il lago. Ebbene, tutto questo avveniva, come detto, in una situazione di regole molto relative, quindi c'era il rischio, come si è verificato in questo caso, che le cose andassero storte. Finché andava storta la costruzione di uno skilift, lo si smantellava e la cosa era risolta; mentre è diverso se va storta la costruzione di una diga. Credetemi, bisogna andare a vedere a vedere per capire cosa è successo al monte Toc, che aveva - lo si vedeva prima che crollasse - la sua stratificazione rivolta verso il basso in direzione del lago. Era ovvio, con il senno del poi, capire che sarebbe venuto giù, però allora c'era questo slancio, tipico del *boom* economico, di fare. Anche oggi noi ci troviamo in un momento in cui vogliamo fare: vogliamo realizzare il benessere della nostra gente usando la montagna, in maniera corretta, per produrre ricchezza. Ecco, quello che oggi non dobbiamo fare è come si fece allora, e cioè dobbiamo studiare prima che cosa potrebbe accadere. Oggi abbiamo le leggi, abbiamo la VIA, abbiamo la VAS: sono tutte cose che fanno burocrazia, e la burocrazia, come sappiamo, è la nostra peggiore nemica, la peggiore nemica del del fare. Però questa burocrazia è necessaria, poiché bisogna essere attenti a seguire quello che ci dice il territorio attraverso gli occhi di chi lo conosce e di chi lo sa studiare. Credo che questo sia l'insegnamento più grosso che ci dà quella tragedia. Il ricordo commosso va agli oltre 1.900 morti, alle loro famiglie e a quello che ha dovuto patire la valle del Piave per ricostruirsi. Se voi andate lì adesso, vedete che non c'è più traccia di quell'immane tragedia, perché quella della valle è una popolazione laboriosa che si è costruita un futuro. Ebbene, questo messaggio deve rimanere, ma soprattutto dobbiamo prevenire, come diceva prima di me il senatore Martella, il rischio che queste cose succedano ancora. Ne approfitto, senatore Spagnolli, per ricordare che, su sua iniziativa, oggi alle ore 20 in Sala Nassiriya viene proiettato il docufilm "Pericolosamente vicini" - io ci metterei un punto di domanda - sugli orsi. Le ho fatto pubblicità.

nel bacino del lago artificiale della diga del Vajont, alta 250 metri. Un'onda di 50 milioni di metri cubi, di cui soltanto la metà scavalca la diga, ma è sufficiente per correre nella gola che conduce a Longarone e in pochi minuti spazza via interi paesi. 1918 vittime, di cui molti bambini e molti adolescenti, diversi dei quali mai più ritrovati. La sera - è stato detto e lo ricordiamo oggi del 9 ottobre 1963 passerà alla storia come una delle pagine più tragiche e drammatiche dell'intera vicenda civile del nostro Paese. Ma quella del Vajont - ha molta ragione, a mio avviso, il senatore Martella che l'ha ricordato - non fu una questione di natura crudele, quanto piuttosto una tragedia annunciata, che oggi ci fa dire come non sia soltanto necessario piangere le vittime e tramandare il ricordo, ma soprattutto imparare qualcosa. Come ha detto Renato Migotti, che all'epoca aveva sedici anni ed è stato per molti anni presidente dell'Associazione dei superstiti, sessant'anni dopo il peggiore disastro che potremmo commettere è dimenticare e ripetere gli stessi errori. Sì, perché quella del Vajont non fu una fatalità, ma una catastrofe causata dall'uomo e dalla logica del profitto a tutti i costi. Ricordare il Vajont vuol dire anche ricordare la la voce che aveva cercato di mettere in guardia l'attenzione pubblica sui rischi di quel progetto, presentato all'epoca come un prodigio dell'ingegneria, candidato a diventare un impianto idroelettrico da primato mondiale. Quella voce era - è stato anche questo giustamente ricordato - quella di Tina Merlin - la voglio citare anch'io in quest'Aula - una coraggiosa giornalista dell'Unità, partigiana prima ancora, che invano aveva scritto dei pericoli della diga e che, per tutta risposta, non solo non venne coinvolta sufficientemente, anzi venne ignorata dalle istituzioni e fu finanche processata, sebbene poi fortunatamente assolta. Soltanto vent'anni dopo, nel 1983, riuscì a trovare un editore per pubblicare il suo libro "Sulla pelle viva", la drammatica testimonianza di quello che era accaduto. Non fu sufficiente denunciare, prima di quel tragico 9 ottobre 1963, gli affari della società elettrica che aveva progettato la diga, la SADE; non fu sufficiente raccontare dei terreni argillosi, dei boati, delle frane, dei sismi. Non fu sufficiente dare voce alle paure degli abitanti di Erto, di Casso, di Longarone, di queste piccole comunità montane della valle, che pensavano e temevano come quel luogo scelto per il progetto non fosse quello giusto. La gente protestò, ma la società di elettricità non volle ascoltare. Aveva dalla sua parte la politica, o almeno larga parte di essa, le concessioni governative, i mezzi di informazione, che anche dopo il disastro si limitarono a parlare in larghissima parte di tragica e crudele fatalità naturale. Dinanzi alle proteste si intervenne con la forza e, nonostante la montagna desse segni di cedimento, si decise di andare avanti lo stesso, di falsificare i documenti, di cancellare i rapporti inviati alle autorità. Come si legge proprio nel libro di Tina Merlin, resterà un monumento a vergogna perenne della scienza e della politica, un connubio che legava quasi tutti gli accademici illustri del potere economico: in questo caso il monopolio elettrico della SADE, che a sua volta si serviva del potere politico per realizzare grandi imprese dalle quali ricavare grandi profitti. La regola era all'epoca, ma purtroppo ancora oggi, quella dello scambio. Da questo coro si sottrasse - anche lui penso che vada richiamato in quest'Aula oggi - un ingegnere geologo, era stato anche lui un giovanissimo partigiano della Brigata Garibaldi. Si chiamava Floriano Calvino ed era il fratello minore di Italo Calvino, docente universitario, unico esponente del mondo cattolico che accettò di produrre una consulenza tecnica senza pregiudizi, rendendo giustizia agli alluvionati. Ebbene, penso che il coraggio suo e della Merlin valgano oggi come un gran… Ed è per questo, Presidente, anche per questo, che io penso oggi sia doveroso ricordare il Vajont, per stringerci attorno a quelle popolazioni, ma anche per non ritrovarci in futuro a piangere altre vittime innocenti. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia si vuole associare al ricordo della tragedia del Vajont. Sono passati esattamente sessantun'anni da quel 9 ottobre 1963 in cui crollò una gigantesca frana nel lago a monte della diga del Vajont, facendo tracimare un'onda di acqua che travolse i paesi che erano lungo la sua strada, sia a riva che a valle. In pochi minuti furono spazzati via case, oggetti e uomini, registrando ben 1.910 vittime, la maggior di queste a Longarone, ma anche a Codissago, a Castellavazzo, a Erto e a Casso. L'onda fu però talmente grande che, scendendo lungo la valle del Piave, colpì anche i Comuni di Soverzene, Ponte nelle Alpi, Borgo Piave nella città di Belluno, e Vas. Mentre l'infrastruttura della diga tenne, si puntò il dito sulla fragilità del territorio, su quel grande bacino idroelettrico, su cui era stato progettato e costruito. Quindi la negligenza, o meglio l'errore dell'uomo, concorsero ad amplificare un evento naturale come quello di una frana disastrosa. Per assurdo, quella che era stata una grande opera di ingegneria, iniziata nel 1957 e finita nel 1959, si rivelò un colossale errore progettuale e dopo molti anni vennero condannati gli ingegneri che avevano progettato l'impianto. Quello che però ha lasciato il segno nella memoria collettiva fu la reazione a quella tragedia e la voglia di ricostruire quanto era stato distrutto, anche se in modo differente. Le vite perse di tutte le vittime di quella tragedia, purtroppo, furono un doloroso tributo a quegli errori e a quelle colpe. Oggi la diga rimane un luogo della memoria di quella tragedia ed è oggetto di visite assieme ai borghi di Erto e Casso a monito duraturo di quanto successo e che non dovrà succedere più. I disastri cui abbiamo assistito nelle ultime settimane e negli ultimi tempi, a causa delle bombe d'acqua, delle alluvioni, del cambiamento climatico che hanno devastato interi territori, ci devono spronare a interventi sul territorio, che tengano sotto controllo il dissesto idrogeologico. Opere fatte bene possono eludere il ripetersi di enormi danni materiali e, soprattutto, evitare quel tributo di vite umane che portò con sé la tragedia del Vajont. Questo è il monito che traiamo oggi per l'attualità da quella grande tragedia. *(Applausi)*.

Ricordo che la prima volta che ho sentito parlare del Vajont risale a circa venti anni fa, in tardissima età. Questo perché è una tragedia che, per quanto annunciata, non è mai stata

È sulle spalle di chi è rimasto tutto il segno di quella tragedia. Sabato ho partecipato con il sindaco di Longarone a un convegno di circa quattro ore, in cui associazioni familiari vittime del Vajont ed altre associazioni ci chiedevano, oltre la memoria e la commemorazione, di fare qualcosa di concreto. Noi abbiamo depositato con altre forze politiche un disegno di legge costituzionale che modifica l'articolo 111 della Costituzione per inserire tutte le vittime di reato Non c'è l'accordo di tutti i Gruppi. Credo però che sia nostro dovere provare a superare tutte le divergenze che ci sono per fare in modo che queste tragedie non solo insegnino, ma portino poi degli atti concreti per superare quelli che sono gli effetti nefasti su Io credo che sia un dovere di tutti noi che siamo in quest'Aula e uno sforzo che mi auguro sia condiviso da tutte le forze politiche per realizzare questa modifica costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, come senatore del Friuli-Venezia Giulia, non senza commozione intervengo oggi per ricordare una delle tragedie più dolorose della nostra storia, il disastro del Vajont. Voglio anche inquadrare storicamente il momento in cui sono avvenuti questi fatti: siamo negli anni Cinquanta, quando l'Italia, un Paese in fortissimo e veloce sviluppo, ha bisogno di energia elettrica. In questo piano viene progettata anche la diga del Vajont, che andrà a creare un bacino artificiale lì in quella gola, che è formata tra il torrente Vajont in provincia di Pordenone nel Comune di Erto, uno dei paesi colpiti. I lavori termineranno nel 1960, si trattava allora della diga più alta al mondo e addirittura oggi è tra le sette dighe più alte a livello globale. Lì, però, dietro quella diga, si muoveva - era evidente, si sapeva il monte Toc, il cui nome non a caso in lingua friulana significa "pezzo", proprio a significare la sua fragilità. I movimenti del monte, una volta riempito il bacino, aumentarono in maniera considerevole, mettendo tra l'altro in allerta - e qui è il nostro rammarico - i gestori della diga. Nell'ottobre del 1960 i movimenti del pendio arrivarono alla velocità, documentata proprio dagli atti di quel periodo, di tre centimetri al giorno. La ditta SADE, che si occupava di quella costruzione, se ne accorse, ovviamente, ma era evidente, erano state fatte delle perizie commissionate al famoso geologo austriaco Leopold Müller, che diagnosticò che lì c'era una frana di due chilometri, profonda centinaia di metri, ignorata da tutti. Le soluzioni, però, non c'erano e se furono introdotte erano ormai tardive. Così, come è stato detto dai miei colleghi, nella sera del 9 ottobre 1963 si staccò dal monte Toc quella frana lunga più di due chilometri, composta da oltre 270 milioni di metri cubi fatti di terra e di rocce. L'impatto della frana con quel bacino creò tre gigantesche onde, due colpirono gli abitati di Erto e di Casso distruggendoli, la terza poi si riversò su Longarone. Si calcola poi che la forza d'urto proprio di quest'ultima onda d'acqua, soprattutto fatta da rocce e detriti, che finì poi per abbattersi sull'abitato meridionale di Longarone, portò a uno spostamento d'aria del tutto simile a quello provocato dalla bomba atomica di Hiroshima. Il 9 ottobre 1963 quasi 2.000 vite, tra cui - lo abbiamo ripetuto e ci teniamo a sottolinearlo - 487 bambini innocenti a cui fu evidentemente negato un futuro, furono strappate via in pochi terribili minuti, distruggendo intere comunità e lasciando una ferita profonda e ancora aperta nel cuore della nostra terra. È nostro dovere ricordarli perché il loro sacrificio non sia stato vano.

che auspico venga ratificata al più presto anche dalla Camera dei deputati. Si tratta della modifica della denominazione della Giornata in memoria delle vittime dei disastri ambientali causati dall'incuria dell'uomo, dove tutti assieme abbiamo deciso di togliere quel termine "incuria" in quanto questi disastri sono stati causati dall'uomo. *(Applausi)*. una piccola differenza, ma di grande importanza: le tragedie come quella del Vajont non sono il frutto di un caso o di una negligenza temporanea, ma di scelte consapevoli, di errori di valutazione e, purtroppo, anche di interessi economici anteposti alla sicurezza delle persone. Non possiamo, dunque, più parlare di incuria, dobbiamo riconoscere la responsabilità umana in tutta la sua gravità e forse questo contribuirà anche ad una La tragedia del Vajont deve rimanere un monito per tutti noi, dobbiamo imparare dagli errori del passato e costruire un futuro più giusto, un futuro più sicuro e, soprattutto, più rispettoso per tutti. Solo così potremo onorare davvero la memoria delle vittime e garantire che nulla di simile possa più accadere.

del processo rimanessero a Belluno, dove con tanta cura e tanta maestria li abbiamo conservati dopo il terremoto dell'Aquila, perché per noi bellunesi non sono solo 5.205 fogli di carta, ma sono qualcosa di Nell'intervenire faccio mie le parole di un altro bellunese, Dino Buzzati, che, quando scrisse di Vajont, disse: è come chiedere a un uomo di fare il necrologio alla morte del proprio fratello. È con la stessa commozione e con lo stesso coinvolgimento che oggi anch'io intervengo in Aula per ricordare le 1.910 vittime, quasi 500 delle quali bambini, come è stato ricordato, che la che la tragedia del Vajont vide morire dopo che l'onda d'acqua e l'aria distrussero gli abitati dei Comuni di Longarone, dell'allora comune di Castellavazzo (oggi Comune di Longarone) e dei Comuni di Erto e Casso. Tale tragedia ha sconvolto profondamente non solo l'Italia intera, ma

accanto a lei ci sono un giovane Giampaolo Pansa, Indro Montanelli ed altri, come lo stesso Buzzati, che hanno raccontato magistralmente quella catastrofica quella catastrofica valanga d'acqua che si è abbattuta sulla terra e sulla nostra gente nel pieno del sonno, quasi fosse qualcosa di ancor più vigliacco, che colpisce la gente nel momento in cui era più debole e indifesa. Difficilmente ciò potrà essere dimenticato, perché ancora oggi quella è la valle della sciagura. Fango, silenzio, paura e dolore, nient'altro era rimasto; un disastro talmente grande che oggi non si definisce il disastro del Vajont, è comunemente chiamato il Vajont e a tutti richiama già quel terribile disastro. Non una speranza si percepisce nei racconti di chi è sopravvissuto, se non attraverso i volti degli alpini della Cadore, delle altre Forze armate, dei Vigili del fuoco, dei tanti soccorritori che in quelle ore di agonia, con fiducia e determinazione, hanno cercato, scavato e camminato in un letto di terra e di detriti. Uno scenario apocalittico di guerra si era battuto su una valle ormai stravolta e che solo le luci dell'alba hanno consentito di vedere nella sua drammatica interezza. Emblematica è una foto, quella della scuola da campo che gli alpini allestirono

più bella della speranza di un popolo che si è rialzato dopo pochissimi giorni e che abbiamo visto agire nelle stesse condizioni nel 1976, quando Gemona fu colpita dal terremoto. Si tratta di una voglia straordinaria, di una forza straordinaria di un popolo del Nord-Est, che mai si è arreso neanche davanti a tragedie come queste. Il Vajont, però, rappresenta per la nostra Nazione il simbolo dell'errore che diventa orrore, signor Presidente. Errare per profitto, per egoismo, per superbia, sottovalutare la natura e i suoi limiti, forzare il rischio fino al punto massimo di tenuta, questa è la storia del monte Toc e della valle del Vajont; un racconto ammonitore,

dell'umanità. Si tratta di una dolorosissima lezione da cui non smettere mai di imparare e sulla quale continuare a fare opera instancabile di prevenzione. Affrontare le grandi sfide epocali nel pieno rispetto della natura che ci ospita è la vera risposta ad una delle pagine più buie che l'Italia ricordi. Avere il coraggio di ascoltare i territori, la sua gente, le sue sentinelle; avere la lungimiranza e l'intelligenza di fare la differenza sul rischio idrogeologico, con azioni ed interventi determinanti. Rispettare le montagne, averne cura, a partire dalla gente che le abita, veri e propri custodi di un patrimonio che il mondo ci invidia, è un impegno che la politica deve prendere sul serio, senza tentennamenti e senza passi falsi; a maggior ragione in una terra come il bellunese, dove una diga non è solo un'opera ingegneristica, ma il simbolo di una ferita ancora aperta. Lo dobbiamo a chi, vittime sopravvissute di quella notte del 9 ottobre 1963, non conosce pace. Ringrazio tutti voi per questo doveroso ricordo ammonitorio, come è stato detto.

Il provvedimento, di iniziativa del senatore Zanettin, nella sua originaria formulazione si componeva di tre articoli. L'articolo 1 apportava delle modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale, rafforzando il divieto del sequestro e del controllo delle comunicazioni, comunque riconoscibili come intercorrenti tra L'articolo 2 modificava l'articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di proroghe delle operazioni captative successive alla prima, se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione non fossero emersi elementi utili alle indagini. Nel corso dell'esame in Commissione, sono state espunte dalla proposta di legge le disposizioni in tema di comunicazioni tra imputato e proprio difensore, in quanto la materia è stata oggetto di intervento da parte dell'articolo 2 della legge n. 114 del 2024. Il disegno di legge, quindi, oggi consta di un solo articolo. Il comma 1 aggiunge un ulteriore periodo all'attuale articolo 267 del codice di procedura penale, introducendo un limite di durata complessiva per operazioni captative non superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione. Ricordo che l'attuale vigente articolo 267 del codice di procedura disciplina i presupposti e le forme del decreto di autorizzazione delle operazioni captative. Oltre ai presupposti in presenza dei quali può essere disposta l'intercettazione, le condizioni che legittimano la richiesta sono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura, la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 267, il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione deve indicare le modalità e la durata delle operazioni. La durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di quindici giorni, sempre che permangano i presupposti del provvedimento. A questo comma, pertanto, è stato aggiunto un nuovo comma, come risulta dal presente disegno di legge. Ricordo che nel disegno di legge c'è il comma 2 dell'articolo che interviene sull'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, che è stato convertito nella legge 203

per i quali si applica la disciplina dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152. È opportuno ricordare all'Aula che l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 reca una deroga alla disciplina contenuta dall'articolo 267 del codice di procedura penale sopradescritto,

sufficienti indizi di reato, anziché gravi indizi, e quando è necessaria per lo svolgimento delle indagini, anziché assolutamente indispensabile. Nelle stesse ipotesi, le intercettazioni ambientali sono consentite nel domicilio o altro luogo di privata dimora, anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

il provvedimento che l'Assemblea si accinge a esaminare rappresenta perfettamente lo stato confusionale in cui versa l'attuale maggioranza di Governo relativamente al settore giustizia. Originariamente il disegno di legge aveva ad oggetto le modifiche della disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché di proroga delle operazioni. L'ormai, direi leggendario, disegno di legge Nordio, volto ad assurgere a manifesto delle politiche di centrodestra in materia di giustizia, ne assorbiva, ahimè, parzialmente, il contenuto, andando a normare il divieto di intercettazione tra l'indagato e il proprio difensore, riducendo conseguentemente il dibattito in ragione della mole di mostruosità giuridiche contenute nel *mare magnum* di quel provvedimento. si stava discutendo, esaminando e approfondendo l'argomento in Commissione, con un'attività emendativa *ad hoc,* e invece, con un altro provvedimento (il disegno di legge Nordio, giustappunto) si è deciso di intervenire sul punto, cessando, cassando e annullando tutto il lavoro fatto. Inoltre, dopo la prima scadenza emendativa, ne sono seguite altre due: la prima relativa alla presentazione di un emendamento della relatrice e la seconda alla riformulazione dello stesso. Quest'ultima scadenza, che, in buona sostanza, rivoluzionava il disegno di legge, è stata prevista per il giorno successivo rispetto a quando veniva proposto. In buona sostanza, per emendare il presente disegno di legge, la Commissione

(data in cui è stata presentata la riformulazione dell'emendamento)? Che il pubblico ministero non può intercettare per più di

mani nei capelli. Attualmente il gip, nel valutare la richiesta del pm, deve innanzitutto prendere in considerazione la propria competenza territoriale e funzionale; successivamente, i limiti di ammissibilità sanciti dall'articolo 266, cioè i limiti di pena previsti, ovvero la rispondenza al catalogo dei delitti ivi indicati; infine, i presupposti di merito di cui all'articolo 267, quindi i gravi indizi di reato e, successivamente, l'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini. L'assenza anche di una delle citate condizioni comporta l'inammissibilità della domanda del pm. L'assenza anche di una delle citate condizioni comporta anche l'impossibilità di poter ottenere una proroga delle intercettazioni che, ricordo a me stessa, allo stato attuale possono essere disposte per tutta la durata delle indagini preliminari. Non sono una penalista, ma, leggendo la norma, così come è stata formulata, sembrerebbe che quarantacinque giorni di intercettazione siano sufficienti gli attuali presupposti, mentre a decorrere dal quarantaseiesimo, per essere autorizzato il successivo periodo di ascolto, serva un *quid pluris* ulteriore, ovvero l'emergere di ulteriori elementi specifici e concreti tali da giustificare l'assoluta indispensabilità delle operazioni. Quindi, anche qualora siano sussistenti tutti gli elementi che attualmente occorrono per disporre le intercettazioni, tali non risulterebbero sufficienti per la proroga, poiché manchevoli del requisito degli ulteriori elementi emersi nel corso dei rischia cioè di avere un impatto fortissimo sull'efficacia delle indagini, senza che la scelta di questo termine abbia una specifica ragione nella prassi giudiziaria. Si tratta, in sostanza, Presidente, dell'ennesimo ideologico salto nel buio, che non ha alcuna attinenza con la realtà. Va infatti sottolineato come sia difficile l'acquisizione di elementi specifici e concreti nei primi giorni delle intercettazioni, che spesso hanno un carattere ambiguo, in quanto gli indagati usano sovente linguaggi cifrati che diventano più chiari soltanto quando tra interlocutori si abbassa la guardia. Proprio in queste occasioni possono emergere quegli elementi specifici e concreti che la norma richiede. Ciò accade raramente nei quarantacinque giorni: mi sembra un rischio più che eccessivo. Non ravvedo un equo contemperamento tra i valori costituzionali previsti dagli articoli 15 e 27 della Costituzione. Un ulteriore elemento, signor Presidente, su cui vorrei rendere edotta l'Assemblea: la norma è scritta *sic et simpliciter*, senza eccezioni. Le uniche sono quelle previste del doppio binario mafia e terrorismo; nient'altro, Presidente. Noi, tra Noi, tra gli altri, proponiamo anche di estendere una normativa derogatoria - chiedo grande attenzione sul punto - anche nei confronti delle donne vittime di violenza. Non c'è ragione per dire di no agli emendamenti che abbiamo presentato sul punto. Infatti, la riduzione temporale della possibilità di intercettare appare molto rischiosa, in quanto espone noi donne ai delitti che attentano alla nostra sicurezza, anche solo percepita, in ragione della riduzione degli strumenti volti al contrasto. Le intercettazioni sono assolutamente necessarie per provare la violenza, in particolare quando c'è reticenza da parte della persona offesa nel farla emergere. Un ulteriore elemento di criticità è dato dal fatto che, qualora la violenza fosse perpetrata in un periodo antecedente rispetto all'autorizzazione delle intercettazioni e nei successivi quarantacinque giorni non emergano elementi ulteriori, specifici e concreti rispetto a quelle che hanno giustificato l'utilizzo delle intercettazioni, non sarà più possibile proseguire all'ascolto. Vi rendete conto della gravità? Tema simile potrebbe anche essere quello del regime derogatorio per i delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, molto spesso le intercettazioni rappresentano l'unico - e ripeto l'unico - strumento adeguato al fine di rompere il rapporto sinallagmatico tra corrotto e corruttore. Mi auguro - e concludo Presidente - che nel corso dell'esame la maggioranza torni sui propri passi e valuti positivamente il lavoro delle opposizioni. Potrebbe essere il provvedimento giusto per iniziare la redenzione in materia di giustizia. *(Applausi)*.

con questo provvedimento si intende mettere un tetto alla durata delle intercettazioni per tutti i reati, a parte qualcuno di cui poi dirò, tetto che è stato fissato in

basata su dati, su una durata media di intercettazioni oggi nel nostro Paese, per cui si può ritenere che quella sia la durata media e quindi il termine massimo da utilizzare? Questo numero, quarantacinque giorni, è stato scelto a caso

è stato indicato in totale assenza di qualunque istruttoria. Su questo provvedimento di legge così delicato, che riguarda la durata massima delle intercettazioni, noi in Commissione non abbiamo fatto alcuna istruttoria, perché si è detto - lo ha detto la Presidente, in modo secondo noi del tutto irragionevole - che, siccome avevamo fatto l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, non c'era bisogno di fare un'indagine puntuale su un provvedimento così delicato che riguarda la durata massima delle intercettazioni. È stato quindi messo questo numero, che non si sa bene da dove salti fuori. La cosa grave è che questo numero di quarantacinque giorni, che è il tetto massimo di durata delle intercettazioni, si applica a tutti i reati, salvo quelli che riguardano la criminalità organizzata e il terrorismo. Lo ripeto: tutti i reati. Colleghi, questo significa che per tutti i reati, tranne criminalità organizzata e terrorismo, ci sarà un tetto massimo di durata delle intercettazioni di quarantacinque giorni, a meno che

un giudice delle indagini preliminari abbia dato la possibilità di fare intercettazioni perché ci sono gravi indizi di colpevolezza a carico di una persona

giorni, se non ci sono elementi specifici e concreti che giustifichino la richiesta di proroga, si spegne l'interruttore.

per avere un'ulteriore proroga, altrimenti questa non può esserci. Colleghi, si sta mettendo una tagliola clamorosa alla possibilità di fare indagini, nelle quali intercettazioni sono indispensabili, su reati anche molto gravi. Non è così che si legifera, è pericoloso questo modo di legiferare. Possibile che non ci si renda conto dei rischi che si stanno correndo? Noi eravamo disponibili a discutere sull'opportunità di mettere un tetto alla durata massima delle intercettazioni; è giusto ragionare di questo, ma non si fa così, non in questo modo, poiché è rischioso. Pensate che all'inizio questo testo di legge non prevedeva alcuna eccezione. Nella proposta di legge della maggioranza era cioè previsto che questo tetto di fosse applicabile anche ai delitti di mafia e di terrorismo, per i quali non bastano a volte dieci mesi per avere un quadro chiaro delle responsabilità. È solo grazie alla nostra presenza che vi siete resi conto degli errori clamorosi in cui stavate incorrendo e che si è fatta una modifica in fase istruttoria in Commissione. Questo non basta, perché rimangono fuori troppi reati gravi per i quali le intercettazioni sono indispensabili. L'invito che vi facciamo è di ripensarci: affrontate la fase emendativa in quest'Aula e poi alla Camera per ripensare a una norma e a una riforma che rischia di mettere a repentaglio la possibilità di accertare reati molto gravi. Questo è il rischio che stiamo correndo per una proposta di legge che è stata fatta male ed è superficiale e sbagliata: fermatevi. Signor Presidente, ogni volta che affrontiamo un provvedimento che ha a che fare con la giustizia, riceviamo commenti negativissimi; Come giustamente qualcuno ha sottolineato, sono dovuti a un convincimento ideologico, cioè che il Governo e il centrodestra in generale non siano capaci di mettere in atto provvedimenti che possano contemperare le esigenze di indagine con quelle della libertà dei cittadini. cittadini. Noi troviamo strano che ci sia chi continui ad affermare che i cittadini possano essere ascoltati e intercettati per più tempo, senza che, con lo scorrere del tempo, ma con l'assenza di elementi ulteriori, ci sia la possibilità di fermare l'intercettazione e quindi

con decreto motivato (perché naturalmente il pubblico ministero deve dire il motivo per cui vuole intercettare un libero cittadino), dall'indagine (e non solo dalle intercettazioni che sono state predisposte) debba emergere che quello che

a essere intercettato, senza che l'indagine stia portando a nulla. Se invece l'indagine porta a qualcosa di concreto, come tutti ci auguriamo, quando un'indagine viene iniziata e il pubblico ministero ritiene che sia necessario intrudere nella vita del cittadino attraverso le intercettazioni, e ci sono nuovi elementi, questi possono portare a scatti ulteriori di quindici giorni, senza limite. Quindi in teoria, se

corretto e che non ci sia niente di ideologico nel porre un limite nei confronti di colui che, attraverso l'indagine

intercettare un libero cittadino. Penso che questo sia parte di quella filosofia di trasformazione della giustizia che è alla base dei provvedimenti che stiamo portando in essere e che ha proprio il fine di assicurare la giustizia e contemperarla con la libertà dei cittadini. Ho sentito dire che nei primi giorni di intercettazione uno sta più attento. Se uno è intercettato, normalmente non lo dovrebbe sapere e quindi si continua a comportare come si comportava prima. Non è che dopo dieci giorni, come nel "Grande fratello", si dimentica di essere intercettati e quindi iniziano quegli atteggiamenti per cui molti guardano in televisione

Io penso che, se è in corso un'indagine in cui si pensa che si stia vendendo della droga e la persona coinvolta non fa il verduriere e dice di vendere un chilo di mele, sia facile dirlo già dal primo giorno che quel chilo di mele corrisponde a un chilo di droga.

si è derogato a questa nuova normativa per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Continuiamo a dire che, sebbene siano scomparsi due articoli per quello che è stato detto per le misure del Governo,

non c'è nulla di ideologico: il provvedimento va nel solco della riforma della giustizia che noi abbiamo iniziato due anni fa da quando siamo arrivati al Governo.

Presidente, questo provvedimento arriva in Aula con una grave anomalia. La Commissione giustizia, per prassi, sente gli esperti prima di emanare provvedimenti legislativi; in questo caso, la Commissione giustizia non ha ritenuto necessario sentire gli esperti, cioè quelli che operano sul campo, ossia i magistrati o i poliziotti che ogni giorno utilizzano le intercettazioni. Arriviamo qui senza un minimo di corredo informativo su che cosa stiamo facendo. Non si sa che differenza vi sia tra le intercettazioni ambientali e quelle telefoniche, né conosciamo quale sia il periodo medio

cioè quello entro il quale, sulla base dell'esperienza, sono state captate intercettazioni con elementi significativi da un punto di vista probatorio. Una statistica non ce l'abbiamo non sappiamo se questo periodo cambi a seconda dei tipi di reati, a seconda dei tipi d'autore. Non si sa come funzionino le intercettazioni telefoniche. cui abbiamo a che fare è una criminalità altamente professionalizzata, che quindi, quando comunica, usa un linguaggio cifrato e criptico. In base alla mia esperienza, nei processi di mafia a volte abbiamo impiegato quattro mesi per capire cosa dicevano gli indagati. Vi faccio un esempio concreto: si parlava, in un processo di mafia e appalti, dell'uomo con la S; noi e i carabinieri non l'abbiamo capito, abbiamo preso un'altra pista e dopo cinque mesi abbiamo capito che la persona non era Angelo Siino, ma era un altro. Non è così facile come sembra: non c'è cattiva volontà, è proprio una difficoltà di carattere oggettivo. Non si sa neanche che le intercettazioni telefoniche vengono usate come intercettazioni staffetta,

Quando hai acquisito queste informazioni di base e quindi sai dove si riuniscono e dove parlano in chiaro, senza linguaggio criptato, a quel punto sai dove mettere l'intercettazione ambientale e quindi ascolti chiaramente quello che dicono. giorni sono stati bruciati, utilizzati per capire dove effettuare l'intercettazione ambientale, hai chiuso prima ancora di cominciare. Ecco perché - poi ritornerò sugli altri emendamenti abbiamo fatto una prima distinzione di carattere basico: cominciamo a distinguere la durata delle intercettazioni telefoniche dalla durata dell'intercettazione ambientale e cerchiamo di mettere un periodo che sia parametrato rispetto all'esperienza sul campo, che non è di quarantacinque giorni, perché non stiamo parlando di improvvisatori del crimine, ma di un Paese in cui ormai l'attività criminale si è dematerializzata, come avviene per quella normale. Oggi solo un cretino fa un furto in mezzo alla strada, perché si possono fare un furto, una rapina o un'estorsione con l'informatica si tratta di persone che hanno una capacità criminale che richiede un tempo di investigazione. Ecco perché, con questo primo emendamento, distinguiamo la durata delle intercettazioni ambientali, per le quali riteniamo che ci vogliano almeno centoventi

il senatore Berrino ha detto che questa riforma non è problematica perché stabilisce che le intercettazioni possono, sì, durare

le persone che sono sotto intercettazione hanno un periodo di stasi criminale (uno ha un incidente, oppure l'*iter* di una pratica va avanti) e quindi non si captano

a questo grave *vulnus,* stabilendo che gli elementi specifici e concreti non sono soltanto quelli che si captano di quindici giorni in quindici giorni, perché è evidente a tutti che possono esserci quindici giorni in cui i criminali non fanno comunicazioni rilevanti, ma possono essere anche elementi che si traggono da altre fonti di prova: documenti, dichiarazioni testimoniali o collaboratori. Se sopravvengono queste altre fonti di prova, anche se nei quindici giorni non ci sono elementi specifici, si possono prorogare le intercettazioni.

insieme alla mafia, la forma più grave di criminalità organizzata siano le cosiddette associazioni a delinquere finalizzate alla corruzione, quelle che la stampa chiama comitati d'affari, Si tratta di un esercito sterminato di termiti che, da Bolzano a Palermo, stanno succhiando il sangue vivo della Nazione. Esse hanno la stessa finalità delle mafie: non vogliono commettere soltanto alcuni reati, hanno lo scopo di acquisire il controllo di interi settori della pubblica amministrazione e di diventare monopolisti e oligopolisti nell'assegnazione degli appalti e delle concessioni pubbliche. Proprio per questo motivo, per questa particolare pericolosità, noi abbiamo proposto un emendamento con cui, per questi reati associativi di particolare gravità, il termine delle intercettazioni venga esteso a centottanta

non prevedere una deroga in caso di violenza sulle donne sia una grandissima responsabilità che vi state assumendo nei confronti delle donne che subiscono determinate condotte. Le stiamo lasciando al loro destino, al loro incubo. Io questa cosa non l'accetto e non accetto che l'Assemblea non si esprima in maniera favorevole a questo emendamento.

renderci conto però che stiamo discutendo di una violazione del diritto costituzionale alla *privacy* e alla riservatezza. Ora, se il reato è complesso e richiede che la magistratura intercetti per molto tempo, data la complessità del reato, è giusto che l'intercettazione sia prorogata, ma se si tratta di un fatto di violenza singolo, mi chiedo cosa possa esserci da intercettare per più di quarantacinque giorni. Se si tratta cioè di un singolo atto di violenza, anche grave, credo che in quarantacinque giorni di tempo una magistratura mediamente efficiente riesca a chiarire il caso. Non dobbiamo dire che, siccome il reato è grave, si può violare l'articolo 15 della Costituzione per molto tempo. Dobbiamo dire che il reato è complesso e complicato. È quello che dice il senatore Scarpinato: nei reati di mafia abbiamo bisogno di moltissimo tempo, perché dobbiamo comprendere come si svolge la dinamica delle conversazioni,

lo voglio sottolineare certe volte - siamo a favore della violenza contro le donne, ma perché riteniamo che non sia questo il caso. Va allungato il tempo per l'intercettazione quando la reiterazione

massimo alle intercettazioni per evitare che la continua reiterazione delle proroghe determini un tempo infinito, quindi va benissimo; tuttavia, non si fa così, non con questi termini draconiani non giustificati da nulla: il punto è questo. La previsione

dei quali, se non emerge alcun elemento ulteriore, si spegne e non si ha più la possibilità di utilizzare intercettazioni per accertare l'omicidio di una persona. Ma vi pare possibile? Vi pare sensato? Ha ragione il senatore Scarpinato: bisogna distinguere almeno per fasce di reati. Bisognerebbe avere contezza di quanto dura in media un'intercettazione per accertare un delitto. Non si può scegliere un termine draconiano privo di

Signori, è il caso di intervenire. Non possiamo permetterci di intervenire con l'accetta su un tema così delicato e importante come le intercettazioni.

rimango veramente esterrefatto. Stiamo chiedendo garanzie per evitare che da un buco, come quello del bambino che salvò la diga mettendoci un dito, si apra una voragine, ma nessuno ha detto che ciò sia indulgente verso il cosiddetto carnefice, verso la persona che delinque. Ci mancherebbe. Io divenni

dissi chiaramente: esistono rischi molto forti che "un chilo di bambino" diventi un chilo di eroina prezioso per i singoli delinquenti o associati. Ci mancherebbe altro che ci fosse un minimo d'indulgenza col rischio di far passare inosservate inosservate queste persone, ma non si può aprire per sempre il diritto all'intercettazione. Sono molto d'accordo con il senatore Scalfarotto: ma che ne facciamo della salute e della garanzia istituzionale? Possiamo aprire a vita,

la maggioranza si sia resa conto che contrarre soltanto a quarantacinque giorni il termine massimo delle intercettazioni è un ritiro unilaterale dello Stato nei confronti della criminalità *(Applausi)*, tant'è che ha dovuto stabilire che almeno per mafia e terrorismo quarantacinque giorni non sono sufficienti. Noi chiediamo però alla maggioranza: la strage, l'omicidio,

È veramente un atto di irresponsabilità nei confronti del Paese. Il nostro emendamento prevede invece che sia previsto un termine superiore,

Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, questo è un dibattito molto più serio di quello che pensiamo di liquidare tra opposti schieramenti. Il tema delle intercettazioni, cui viene posto un limite temporale che si può estendere sulla base di un provvedimento motivato del giudice, non è - lo dico con rispetto, ma anche con molta determinazione al senatore Scarpinato - la resa dello Stato rispetto alla criminalità. Se infatti passa questo concetto, affermiamo l'idea che chi intercetta ha sempre ragione mentre gli intercettati sono dei cittadini potenzialmente criminali *(Applausi)* e non dei cittadini sottoposti a una tutela costituzionale.

nella giurisprudenza di questi anni è che un provvedimento di intercettazione privo dei requisiti previsti dall'ordinamento sulla base dei valori costituzionali è

ma non posso accettare che nel dibattito, nella più alta sede democratica del Paese, il Senato della Repubblica assieme alla Camera, si faccia passare il messaggio che chi accetta l'idea di mettere dei limiti sulla base dei valori costituzionali e di un articolo della Costituzione e di provvedimenti della Corte di cassazione,

che abdica di fronte alla criminalità. Non è criminale dire che ci vogliono dei limiti nel tempo dell'infosfera dei diritti, come dice qualcuno. Il tema del rispetto dei diritti e della *privacy* è un tema di diritti umani. Dopodiché si possono avere le opinioni di tutto il mondo sul provvedimento di legge, ma si abbia il rispetto di dire qui, in questa sede, che chi chiede di mettere dei limiti alle intercettazioni non sta facendo un regalo alla criminalità, ma sta difendendo la Costituzione della Repubblica italiana.

Signora Presidente, anch'io devo segnalare un certo disagio per come si è svolto il dibattito. terrei, signora Presidente, a ricordare a tutti noi che, nel momento in cui andiamo a legiferare sul processo penale e nel processo penale, ci muoviamo sempre dentro un terreno estremamente delicato, dove si confrontano due esigenze diverse. C'è un'esigenza dello Stato di reprimere il crimine, di punirlo e anche di prevenirlo. Dall'altra parte - e io temo, signora Presidente, che noi ce ne dimentichiamo spesso spesso - c'è un cittadino o ci sono più cittadini che sono oggetto dell'azione penale. Questi cittadini, fino a prova contraria e fino a sentenza definitiva, sono innocenti. Sta sulle spalle dello Stato l'onere di provare la loro colpevolezza e non viceversa; fintanto che non giunga la sentenza definitiva, questi cittadini devono godere di tutti i diritti costituzionali. Questo significa che l'onere di organizzarsi per reprimere il crimine in modo efficace è dello Stato. Noi non possiamo stabilire di comprimere il diritto del cittadino

Il problema di capire se quell'imputato è colpevole o innocente non è dell'imputato, ma è dello Stato. Allora, se riteniamo di aver bisogno di più mezzi diritto in un tempo minore e arrivare alla verità, che sia lo Stato a dare strumenti alla magistratura e alla Polizia giudiziaria, che trovi i mezzi tecnologici per le intercettazioni meglio funzionanti e così via. legislatori abbiamo il dovere, signora Presidente, di legiferare in maniera generale ed astratta e di ricordare sempre che dobbiamo contemperare questi due valori costituzionali e questi due obblighi che sono davanti a noi. Mi permetta di utilizzare un'immagine paradossale. uno Stato di polizia perfetto, un Paese qualsiasi (non faccio nomi) dove a ogni angolo di strada c'è una telecamera che ti fotografa e controlla ogni tuo spostamento, dove tutti i tuoi mezzi informatici sono controllati dallo Stato, si immagini un Paese così (ce n'è qualcuno). In quel Paese la criminalità sarà zero, signora Presidente, perché per eliminare completamente la criminalità basta eliminare completamente la libertà. Se posso utilizzare un'immagine, la criminalità è l'uso scorretto, sbagliato e perverso della libertà. Tu hai una libertà da parte dello Stato, te ne approfitti e vai contro gli interessi della collettività, facendo del male, perché hai abusato della libertà che ti è stata data. Ora, signora Presidente, io non credo che noi possiamo radicalmente negare quella libertà solo perseguendo l'unico interesse della repressione del crimine, perché purtroppo, anzi per fortuna, siamo uno Stato democratico e dunque dobbiamo ammettere che ci sia qualcuno che utilizza quella libertà in modo scorretto e dobbiamo attrezzarci per fare in modo che chi lo fa sia punito e sia evidentemente repressa l'attitudine di altre persone ad andare in quella direzione. È per questo che noi riteniamo che mettere un tetto

perché non è tanto quello il tema. Devo riconoscere che il collega Bazoli stesso ha detto che c'è bisogno di un limite, perché indosseremo degli occhiali potenti e saremmo molto miopi se non ci rendessimo conto del fatto che spesso lo strumento delle intercettazioni è stato utilizzato abusando anche di quelle che sono le regole. E allora sta a noi legislatori riportare il bilanciamento tra quei due interessi e dire che c'è un tempo massimo che ovviamente non può essere assoluto e inderogabile. È infatti evidente che se nel comprimere quel diritto alla riservatezza si scoprissero fatti che meritano degli approfondimenti, nulla vieterebbe alla pubblica accusa di chiedere al giudice terzo di allungare quel termine. Deve però essere successo qualcosa,

più i primi quindici. C'è scritto «dall'emergere» e non quando. Quindi nel momento in cui il gip si rendesse conto che è indispensabile procedere ancora, bene, lo si faccia, però in mente che siamo in una situazione eccezionale. La situazione nella quale lo Stato è legittimato a entrare nella nostra corrispondenza, nelle nostre vite private, nei nostri *device* elettronici, non è la norma, ma l'eccezione e in quanto tale, essa richiede di essere specificata e regolamentata. Il mio timore è che noi si sia perso un po'

infatti gli interventi di alcuni illustri colleghi, come il senatore Scarpinato, di fatto, sembra che la situazione ideale sarebbe quella di avere l'intercettazione permanente di

che considero me stesso un profondo liberale e sono attaccatissimo ai valori costituzionali, credo che sia proprio indispensabile che noi non indossiamo le casacche delle guardie o dei ladri, men che mai accusando qualcuno di tifare per i ladri perché si stanno difendendo i valori della Costituzione. Gli equilibri di cui

È un appello che parla direttamente alla pancia del Paese. Se però partiamo da questo presupposto, il principio della presunzione di innocenza non esiste più. Dipingiamo altresì un'immagine di un Paese nella quale io sinceramente non mi riconosco.

quindi fare in modo che gli strumenti che mi servono per reprimere il crimine siano commisurati alle mie necessità. Voglio dire, in conclusione, di fare attenzione anche alla vicenda dei reati spia che dobbiamo allargare il novero di tali reati, correndo il rischio di fare la lista della spesa. Ci sono reati spia sui quali dobbiamo agire. Se reato spia vuol dire che una volta ogni 10 o una volta ogni 50 un certo reato ne indica un altro,

diciamocelo, perché a quel punto significa abbandonare le nostre libertà, abbandonarci a uno Stato di polizia, però le dico la verità, signora Presidente: io, in uno Stato di polizia, non mi riconoscerei e non riconoscerei la Costituzione della Repubblica che ho giurato di servire.

provvedimento, che è stato sostanzialmente svuotato nel corso dell'esame in Commissione attraverso la trasposizione delle disposizioni più rilevanti dell'Atto Senato n. 808, che poi, passato alla Camera, è stato definitivamente approvato ad agosto ed oggi è legge. Questo ha sostanzialmente impedito un'analisi completa e organica di tutta la disciplina delle intercettazioni e soprattutto, considerato che il testo oggi all'esame dell'Aula è profondamente cambiato rispetto a quello iniziale, ci troviamo a votarlo senza aver avuto il modo di sottoporre quest'ultimo testo agli operatori del settore. Il testo posto in votazione, infatti, è il risultato di un emendamento, nel suo testo 2, presentato in Commissione in prossimità della fine dei lavori, senza che siano state autorizzate audizioni. Di conseguenza, è pressoché impossibile valutarne gli effetti concreti in rapporto alle attività investigative. Dispiace il voto contrario, perché la questione che il provvedimento vuole affrontare è di certo di interesse anche della mia parte politica. È infatti indiscutibile la necessità di assicurare alla difesa le garanzie stabilite dai principi costituzionali nel bilanciamento degli interessi in gioco, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità, ed è altresì indiscutibile che la Corte costituzionale più volte si sia espressa indicando la necessità di ben delimitare le intercettazioni. Ma è chiaro che le modalità con cui si è giunti in Aula non sono condivisibili e che il rischio di immettere nell'ordinamento un provvedimento che nei fatti limiti l'attività delle procure e ostacoli la funzione giudiziaria è troppo grave per poter essere corso. Diverso sarebbe stato se fosse stata autorizzata un'istruttoria approfondita sul punto, attraverso l'audizione di esperti, istruttoria che la maggioranza non ha consentito. In questo modo si è esautorato il lavoro della Commissione e si è impedito di convergere su un testo più condiviso. Il nostro voto sarà quindi contrario, dato che non è stato possibile accertare che i limiti posti alle intercettazioni - limiti molto ridotti, come è stato detto il testo ammette appena quarantacinque giorni, salvo proroghe in casi specifici non si trasformino in ostacoli alla possibilità di accertare la commissione di reati gravi e di grande allarme sociale, come quelli, per esempio, connessi alla violenza contro le donne. Sarebbe stato davvero importante portare a termine un'istruttoria completa ed eventualmente apportate altre modifiche per evitare complicazioni nello svolgimento dell'attività di indagine. Così però non è stato e di conseguenza concludo annunciando il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

che è uno dei punti programmatici più significativi in tema di giustizia del centrodestra di Governo e del ministro Nordio. Tutto parte dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva che la Commissione giustizia, sotto la preziosa presidenza della senatrice Giulia Bongiorno, ha svolto nei primi mesi di questa legislatura. Ricapitoliamo. La prima *tranche* della riforma ha riguardato il divieto di intercettazione dei colloqui tra difensore e cliente ed è stata approvata all'interno del disegno di legge Nordio, quindi è già legge. La seconda *tranche* riguarda il sequestro degli *smartphone* e dei supporti informatici, la cosiddetta scatola nera della vita di ciascuno di noi; quell'importante disegno di legge è stato già approvato qui in Senato ed è ora all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Viene ora in discussione, appunto, la terza *tranche*, forse la più controversa, come ha dimostrato il dibattito che si è svolto poc'anzi, che riguarda i limiti delle proroghe delle intercettazioni. Nei giorni scorsi questo disegno di legge, a mia prima firma, è stato pesantemente criticato, in particolare dal dottor Di Matteo dalle pagine di un noto quotidiano. Sostiene il dottor Di Matteo che la novella renderebbe più difficoltose le indagini di mafia, perché alcuni dei reati interessati da questa riforma consentirebbero anche di smascherare i mafiosi, quindi limitando le investigazioni si limiterebbero anche le possibilità dei magistrati di colpire la mafia. Dobbiamo intenderci bene, il dottor Di Matteo dice che sostanzialmente ogni reato è mafia, perché perseguendo quel reato si può individuare un mafioso. È la teoria dei cosiddetti reati spia, categoria peraltro metagiuridica, di carattere meramente sociologico, che non trova ingresso in nessun trattato di diritto. È quanto ripete spesso in queste Aule anche il collega Scarpinato, quindi nessun doppio binario è giustificabile: perseguendo anche il responsabile di un semplice divieto di sosta, in effetti, si può incappare in un pericoloso mafioso. A monte di questo ragionamento, però, va risolto un dilemma che definirei quasi filosofico. È del tutto evidente che con gli strumenti tecnologici sempre più sofisticati e in continua evoluzione che la tecnologia ci offre, come *trojan,* telecamere nei luoghi pubblici e privati, intercettazioni telefoniche ed ambientali, riconoscimento facciale di massa di massa (è quanto peraltro sta già accadendo in Cina, in particolare nella provincia del Xinjiang, per la repressione della minoranza uigura), il potere oggi è probabilmente in grado di assicurare alla giustizia praticamente tutti i criminali; anzi, forse è anche addirittura in grado di prevenire i reati con arresti e condanne preventive, mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale predittiva, partendo magari dall'analisi della mimica facciale dei cittadini, dalle frasi pronunciate, dai movimenti del corpo, dalla famiglia di provenienza, dal livello scolastico dell'autore. Ma questo grande fratello è davvero ciò che vogliamo? Personalmente, da liberale, mi ribello a una tale prospettiva. Voglio rimanere un libero cittadino e non diventare un suddito. La questione filosofica ed etica su cui richiamo l'attenzione dell'Assemblea si pone nel corretto rapporto di equilibrio da individuare tra i diversi valori contrapposti: da una parte ci sono le esigenze investigative per reprimere i reati (certamente un valore costituzionale primario), ma dall'altra c'è anche il rispetto della *privacy* e della sfera più intima del cittadino, che pure è un valore costituzionale di altissimo rango, che non può essere violentata e vivisezionata in ogni suo dettaglio, per mesi e anni, alla ricerca del reato che altrimenti non si trova. Il bilanciamento tra i diversi interessi in conflitto vale, colleghi, per tutte le grandi questioni che si pongono all'esame di questo Parlamento. Pensiamo ad esempio al fine vita, di cui, tra l'altro, sono relatore. Anche in questo caso si contrappongono il principio dell'autodeterminazione individuale, da una parte, e, dall'altra, il rispetto della vita sacra e inviolabile; entrambi i valori sono per certi versi inconciliabili e la politica è chiamata a trovare la sintesi più opportuna. È questo il tema di fondo del disegno di legge oggi in discussione: trovare il punto di equilibrio. Per i reati di minore gravità è lecito disporre intercettazioni senza limiti temporali? La mia risposta è un secco no, non ne vale la pena, anche se in qualche caso dalla loro investigazione si incappa in un mafioso. Sfatiamo innanzitutto una mistificazione mediatica: i limiti delle intercettazioni che proponiamo non riguardano i reati più gravi di mafia e terrorismo e le fattispecie più gravi. Terrorismo e mafia sono reati gravissimi e certamente Forza Italia non ha mai avuto nessuna intenzione di restringere gli strumenti a disposizione dei magistrati per combatterli. legge che oggi discutiamo riguarda, invece, i reati che non sono né mafia né terrorismo. Dopo i quarantacinque giorni, la proroga delle intercettazioni è comunque consentita, ma deve essere specificatamente motivata sulla base di quello che è stato acquisito nelle varie investigazioni

Noi chiediamo invece che le proroghe siano giustificate dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. Signora Presidente, io sono rimasto assai sorpreso dalla intervista rilasciata oggi dal procuratore di Genova, dal procuratore di Genova, in cui dichiara che la sua inchiesta sul presidente Toti non si sarebbe potuta concludere se fossero state in vigore le norme che oggi proponiamo, dal che trarrebbe la conclusione che queste norme non vanno bene. È un argomento che mi sarei aspettato dal titolare di una inchiesta esemplare, che ha portato risultati eclatanti di cui andare particolarmente fieri. Non mi pare proprio il caso dell'inchiesta di Genova. Vogliamo fare un bilancio di questa inchiesta? Tre anni di intercettazioni, venti *terabyte* di dati digitali acquisiti al fascicolo processuale. E cosa hanno portato? A 1.500 ore di lavori socialmente utili. Ripeto: 1.500 ore di lavori socialmente utili. È un risultato di cui una procura deve andare particolarmente orgogliosa? Sono davvero sicuri che quella sia un'indagine da portare ad esempio? Ne valeva davvero la pena? A meno che l'obiettivo della procura non fosse la condanna penale, esito normale di un procedimento giudiziario, ma piuttosto il ricambio ai vertici della Regione. In quel caso, però, Presidente, la procura avrebbe commesso un evidente abuso di diritto, un classico *détournement de pouvoir,* per dirlo alla francese, di cui dovrebbe semmai vergognarsi.

Per tutte queste ragioni il Gruppo Forza Italia voterà convintamente a favore del testo in esame. A conclusione, credo sia assolutamente doveroso rivolgere un particolare ringraziamento al vice ministro Sisto, che ci ha seguito in tutto l'*iter*

questo disegno di legge va molto al di là dei suoi fini apparenti. Non è affatto, come lo si vorrebbe far apparire, solo una diversa disciplina tecnica del regime delle autorizzazioni e delle intercettazioni, ma è un atto politico destinato a indebolire gravemente la capacità dello Stato di garantire un efficace contrasto alla criminalità, con gravi ricadute sulla qualità della nostra convivenza civile. un atto di irresponsabilità nei confronti del Paese, che si iscrive in un lucido disegno politico che questa maggioranza governativa persegue sin dall'inizio della legislatura: il disegno di approfittare dei rapporti di forza contingenti, per smantellare selettivamente, uno dietro l'altro, tutti gli anticorpi, tutti i presidi dello Stato contro il dilagare della criminalità dei potenti. Politici e pubblici amministratori, che piegano il potere pubblico al perseguimento di interessi di grandi e piccole *lobby*, affaristi spregiudicati, dediti alla predazione sistematica delle risorse pubbliche, riciclatori di capitali sporchi di ogni genere. È un variegato un variegato mondo di colletti bianchi, sempre più spesso legato da segreti matrimoni di interessi con le mafie. Mafie che hanno capito benissimo che oggi, per arricchirsi a costo zero, bisogna delinquere negli stessi modi in cui delinquono i colletti bianchi, godendo così dei loro medesimi privilegi di impunità di classe. Questa maggioranza ha inaugurato la legislatura premiando l'omertà dei condannati definitivi per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. È quello che la stampa definisce cricche e comitati di affari, che infestano il Paese da Bolzano a Palermo. Infatti, sono cambiate le norme della legge anticorruzione del 2019, in modo che i condannati per questo reato possono uscire dal carcere ottenendo i benefici penitenziari anche se tengono la bocca chiusa sui complici non identificati e sul bottino occultato. La maggioranza ha proseguito cancellando il reato di abuso d'ufficio, ridimensionando il reato di traffico di influenza e quello di peculato per distrazione, facendo così divenire l'Italia un caso unico in Europa, un Paese sempre più simile alle Repubbliche sudamericane. Avete approvato una serie di riforme con le quali avete già limitato il potere di intercettazione per i reati dei colletti bianchi. Dopo aver ridimensionato il controllo di legalità della magistratura penale, vi apprestate a proseguire l'opera castrando anche il potere di controllo della Corte dei conti. E tuttavia, non è ancora sufficiente perché, nonostante tutto questo, le cronache giudiziarie dimostrano come, pur perdendo colpi, la magistratura riesca ancora a portare alla luce una sequenza impressionante di casi di corruzione e malaffare di cui sono protagonisti personaggi dell'*establishment*. la necessità di intervenire in modo ancora più incisivo e radicale. Alla Camera avete così accelerato la riforma della Costituzione per separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri e rendere l'azione penale discrezionale, sottoponendo l'attività giudiziaria al controllo della politica. Ma poiché questa soluzione radicale e definitiva richiede tempi lunghi, era urgente intanto mettere in campo un rimedio di emergenza, rapido, per limitare i danni, cioè per limitare la capacità di investigazione della magistratura inquirente. Ecco, dunque, il colpo d'ingegno di compromettere gravemente l'efficacia delle indagini della magistratura contraendo a soli quarantacinque giorni, prorogabili solo in casi di difficile e incerta realizzazione, l'utilizzazione delle intercettazioni, l'unico mezzo di prova in grado di perforare lo scudo di omertà blindata e complicità trasversale che avvolge l'attività illegale dei ceti superiori. Un mondo, quello dei colletti bianchi, nel quale i reati non si commettono in strada sotto gli occhi del pubblico, ma all'ombra discreta dei corridoi di palazzo. La riforma prevede che dopo quarantacinque giorni non sono più sufficienti i requisiti dei gravi indizi e dell'assoluta indispensabilità dell'operazione, ma occorre anche che dalle intercettazioni disposte nei primi quarantacinque giorni siano emersi elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione. Pertanto, se questi elementi specifici e concreti non sono emersi, cessano le intercettazioni, anche se permangono i gravi indizi di reato e l'indispensabilità delle operazioni, cioè l'impossibilità di acquisire prove con mezzi diversi. Quindi, con questa riforma la maggioranza sta statuendo che per reati gravissimi (come stragi, omicidi plurimi, femminicidi, rapina, estorsione aggravata, reati da codice rosso, tratta di persone, traffico di organi, acquisto e alienazione di schiavi e tanti altri reati previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale) la magistratura può indagare per due anni perché sono reati gravi e tuttavia, quarantacinque giorni, se non ha la sorte di acquisire in tale manciata di giorni elementi specifici concreti, deve staccare la spina delle intercettazioni e proseguire le indagini per altri ventidue mesi solo con gli stessi mezzi che si utilizzavano prima dell'età tecnologica (pedinamento, osservazione a distanza). *(Applausi)*. Siamo, dunque, dinanzi a un vero e proprio favoreggiamento del crimine e a un disarmo unilaterale dello Stato. *(Applausi)*. un prezzo enorme che si fa pagare a tutto il Paese pur di raggiungere il risultato dell'impunità di casta. Ho iniziato questa dichiarazione di voto definendo questa riforma un grave atto di irresponsabilità nei confronti del Paese, del Paese, non solo per i devastanti effetti finali che appare destinato a produrre, ma anche per le palesi anomalie che hanno caratterizzato l'*iter* della sua approvazione in Commissione giustizia del Senato. È gravemente irresponsabile approvare una riforma che riduce a quarantacinque giorni la durata delle intercettazioni, sconvolgendo così, di punto in bianco, i protocolli operativi delle Forze di polizia e della magistratura collaudati nel corso di decenni, senza avere prima sentito la necessità di acquisire il parere degli esperti, di coloro che nella quotidianità operano sul campo del contrasto al crimine. Una mancata audizione degli esperti è anomala perché in palese deroga alla prassi costantemente seguita dalla Commissione giustizia del Senato. Non è stato così possibile acquisire una statistica che indichi quali siano stati, in centinaia di migliaia di indagini, i tempi medi nei quali sono stati acquisiti elementi di prova utili nel corso di intercettazioni. La media è stata di quarantacinque giorni, oppure di sessanta, centoventi, centottanta o di altri ancora? Non è stato accertato se questo periodo utile di captazione sia diverso a seconda che si tratti di intercettazioni telefoniche, ambientali o telematiche e a seconda della tipologia dei reati e degli indagati. Una riforma varata in fretta e furia, senza un corredo di informazioni minimali, indispensabili per non far fare al Paese un salto nel buio, per non causare un ritiro unilaterale dello Stato nel contrasto ai criminali, lasciando i cittadini indifesi. Una grave mancanza di responsabilità che si è manifestata anche nel non aver voluto prendere in considerazione alcuno degli emendamenti dell'opposizione che non avevano intenti ostruzionistici, ma miravano soltanto a modulare la riforma in modo da trovare un bilanciamento ragionevole: dalla tutela del diritto costituzionale alla riservatezza delle comunicazioni alla tutela dei diritti costituzionali dei cittadini alla salvaguardia della propria vita, della propria incolumità fisica e morale, dei propri beni, che possono essere compromessi dal crimine, se la capacità di risposta dello Stato viene depotenziata oltre misura. Sono stati bocciati tutti gli emendamenti proposti proprio al fine di garantire un bilanciamento ragionevole: quello diretto a differenziare la durata massima delle intercettazioni, distinguendo le telefoniche da quelle ambientali;

Viene da chiedersi come vi giustificherete domani, quando di fronte a gravi omicidi, a stragi, a femminicidi, a violenze di gruppo, a rapine a mano armata, la magistratura dovrà deporre le armi e dichiarare *forfait*, perché dopo quarantacinque giorni ha dovuto staccare la spina delle intercettazioni, non essendo stata così fortunata ad acquisire le prove in quel breve periodo. Cosa direte alle vittime e ai loro parenti? Cosa direte alla pubblica opinione per questa denegata giustizia, per questa resa unilaterale dello Stato dinanzi al dilagare del crimine e delle impunità? Sappiamo già che per eludere le vostre gravi irresponsabilità addosserete la colpa all'inettitudine della magistratura e della polizia. Speriamo che quando questo accadrà gli italiani ricordino i volti e le parole di tutti coloro che, oggi, per interessi di casta, hanno contribuito a rendere peggiore la vita di tutti noi. Per questi motivi dichiariamo il nostro voto decisamente contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

devo iniziare questo mio intervento rappresentando lo stupore per i toni ed anche la direzione che ha assunto la discussione in corso, con una tendenza ad un allarmismo veramente fuori fuori luogo, direi certamente motivato dalla capacità del tema di essere facilmente oggetto di uno sfruttamento mediatico che alcune testate - lo si ricordava poc'anzi sono capaci di fare sui temi della giustizia e su quelle che si ritengono essere delle aggressioni a un sistema di indagine, forse tipico di alcuni magistrati nella loro carriera. Poc'anzi un collega ha rappresentato alcune delle tendenze e dei *desiderata* di una parte della magistratura che - lo comprendiamo - è cresciuta in un mondo antico, quel piccolo mondo antico di cui esiste una bellissima pellicola cinematografica,

quei parlamentari che sedevano in queste Aule quando non esistevano i telefonini e avevano la possibilità di studiare un'ora in silenzio in maniera ininterrotta, senza essere frequentemente interrotti, magari dal soggetto criminale. Nelle aule dei tribunali si parla molto di criminali, ma anche nelle Aule del Parlamento probabilmente siamo molto interessati a conoscere, specie grazie ai dossieraggi, quali siano i comportamenti dei colleghi della Lega, che hanno tantissimi beni nascosti e che magari trafficano quantità di valigie di denaro che scorre nelle sedi del nostro partito. Queste fantasie, queste deviazioni, che una parte di servitori dello Stato infedeli pensano di poter continuare a realizzare impunemente in questo Paese, ci portano a riflettere sul fatto che

in modo forse eccessivo. E quando questi giocattoli magari arrivano in mano a qualche soggetto che può essere finito in ruoli apicali grazie ai famosi eventi che conosciamo, come il caso Palamara, è tutto un programma.

sulla quale si usa autorizzare una intercettazione, è pur sempre di base fondata su gravi indizi di reato, e l'intercettazione deve essere assolutamente indispensabile. non capisco quale possa essere l'allarmismo se, dopo quarantacinque giorni, si introduce non un divieto, non un impedimento,

di giustificare, semplicemente adducendo elementi specifici e concreti e una motivazione. Non chiediamo molto e sappiamo bene come nella prassi sarà assolutamente facile dimostrare la sussistenza di elementi specifici e concreti: magari il fatto di aver visto l'indagato uscire più volte da un appartamento o averlo visto transitare in luoghi sospetti rispetto al capo di imputazione che si è formulato.

polizia giudiziaria che dispiegano molte ore di straordinario nelle sedi della procura, per comporre tutto quel quadro indiziario che sarà poi utile a condannare i veri criminali,

immateriale tra persone avveniva saltuariamente con quell'apparecchio, che molti magari non hanno conosciuto, che si usava attivare girando con il dito un quadro con dei numeri, e c'era quella famosa specie di rondella che girava (io l'ho conosciuta), e che oggi non si usa più. La massiva La massiva capacità di comunicare permette, in pochissimi giorni, di avere un quadro completo della potenziale efficienza criminale di un soggetto. E se quell'efficienza criminale supera i limiti della democratica opportunità di tollerare determinati comportamenti, ricordo che una legge - legge che permette, per i più gravi reati, di derogare a quella previsione che stiamo trattando di inserire nell'ordinamento - consente specificamente di ritenere sufficienti dei meri indizi e di giustificare semplicemente la necessità dell'intercettazione. Faccio appunto riferimento all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 che disciplina la lotta alla criminalità organizzata. Quindi, vi è un altro scalino che stavolta, invece, semplifica la possibilità di intervento dell'organo inquirente, allorché la pericolosità sociale di un gruppo di associati che intenda perseguire un'attività criminale sia tale da qualificare il capo di imputazione in qualcosa di ben più grave che non il semplice reato che prevede nel massimo la pena oltre i cinque anni. Quindi, anni. Quindi, non capisco quale possa essere il livello di allarme che i colleghi dell'opposizione ci hanno rappresentato, quando il quadro delle potenziali armi in mano ai nostri uomini delle Forze dell'ordine è tale da garantire un livello di sicurezza eccellente. Quello che non è assolutamente tollerabile sono purtroppo quei casi - lo ricordavo prima - di assoluta indecenza civile e democratica, allorché vi siano dei soggetti deviati

livelli apicali di quella magistratura che noi vogliamo tenere pulita da una serie di soggetti che riteniamo indegni di ricoprire quei ruoli in qualunque nostra sede istituzionale. In questa sede In questa sede noi abbiamo l'opportunità di votare - e anticipo qui il voto favorevole della Lega su questo provvedimento un nuovo modo di calibrare lo strumento dell'intercettazione. E abbiamo l'opportunità di farlo nell'assoluta tranquillità e nell'assoluta garanzia di permettere alle nostre autorità inquirenti di fare bene il loro lavoro. Noi glielo auguriamo e saremo sempre al loro fianco.

Il vostro liceo è intitolato a una vittima della strage di Piazza della Loggia, un attentato terroristico di matrice neofascista. Non so se sapete che in quest'Aula siede il figlio di Giulietta, il senatore Bazoli.

della giustizia di questo Governo e della maggioranza, che segue un percorso coerente. Da una parte ci sono annunci e proclami di rivoluzioni, per rendere - si dice - la giustizia certa e veloce, prevedendo invece giri di vite con l'introduzione di nuovi, improbabili e perfino pericolosi reati che attentano ai diritti e alle libertà individuali delle persone, quello di manifestare le proprie opinioni, come per esempio prevede il disegno di legge sulla sicurezza. Ricordiamo la foresta, la vostra giustizia da palinsesto televisivo, il vostro panpenalismo securitario, come si dice: anti-*rave*, anti-imbrattatori, il decreto Cutro, le pene per manifestazioni e perfino per resistenza passiva nelle carceri, per non dimenticare la non obbligatorietà del differimento della pena per le donne incinte e le madri di bambini fino a un anno di età. Sono cose veramente molto gravi. *(Applausi)*. Altro che garantismo. Voi siete unilateralmente garantisti, solo verso alcuni. Ma in realtà, a partire dal ministro Nordio, siete dei manettari, perché avete istituito più di 30 reati, avete alzato le pene, avete riempito le carceri, anche minorili, con tanti ragazzi. *(Applausi)*. Questo non è garantismo: questo è manettarismo. Vedete: certi reati si affrontano anche penalmente, ma voi non avete proprio nei vostri radar la consapevolezza che molte di queste situazioni derivano dal fatto che non siamo stati, come Paese, in grado di affrontare le sacche di disagio, le grandi questioni sociali, le marginalità che spesso sono legate alla criminalità. Dentro questa strategia - e questa è l'aggravante - c'è anche il tentativo di delegittimare la magistratura secondo un disegno ormai chiaro, quello di minare e colpirne l'indipendenza e l'autonomia, e l'autonomia, cercando di rendere più complesso e tortuoso l'esercizio dell'azione penale, specialmente per alcune fattispecie di reati che nel dibattito corrente vengono spesso chiamati dei cosiddetti colletti bianchi. Non siamo solo noi, forza di opposizione, a dirlo - come

nel *report* sullo Stato di diritto, l'Unione europea si dice molto preoccupata per le recenti riforme della giustizia italiane. Le parole dovrebbero far riflettere. In Italia - scrive l'Unione europea - c'è una nuova legge che abroga il reato di abuso d'ufficio, che limita la portata del reato di traffico di influenza; potrebbe avere anche implicazioni per l'individuazione e l'investigazione di frodi e corruzione. E ancora: le modifiche proposte alla prescrizione potrebbero ridurre il tempo a disposizione per condurre procedimenti giudiziari per reati penali, compresi i casi di corruzione. Non mi soffermo più di tanto sugli attacchi che Governo e maggioranza rivolgono, un giorno sì e l'altro pure, in varie forme, con vari provvedimenti e parole, all'informazione e al giornalismo d'inchiesta, colpiti quotidianamente da attacchi, restrizioni, sanzioni, querele temerarie,

come ha detto il Garante della *privacy* - da quando il ministro Orlando ha riformato le norme, non esistono più. In realtà, voi non volete colpire le gogne mediatiche: voi temete il contropotere della libera informazione. Arriviamo così, all'albero, al disegno di legge Le finalità che voi indicate appaiono deboli e anche ipocrite. Il ministro Nordio, non leggendo evidentemente i rapporti dello stesso Ministero e i dati relativi ai costi, parla di spese insostenibili per le intercettazioni. Sono affermazioni infondate per due motivi. Il primo è che non è vero che le spese di intercettazioni sono aumentate, perché negli ultimi dieci anni esse si sono ridotte. Il tanto vituperato *trojan*, che va usato con moltissima cautela,

Il secondo motivo - come hanno ricordato in diversi - è che, grazie alle intercettazioni, si colpiscono e si scoprono reati. Ma, in seguito a sequestri e confische cautelari, anche definitive, lo Stato italiano, grazie anche allo strumento di indagine delle intercettazioni, rientra in possesso di beni mobili e di beni mobili e immobili frutto di condotte illecite. Il costo delle intercettazioni, che non è quello che si favoleggia anche dal punto di vista finanziario, viene ampiamente ripagato dal fatto che lo Stato, seguendo l'insegnamento di Falcone e la legge Rognoni-La Torre, colpisce

che molti reati corruttivi vengono compiuti da persone della criminalità organizzata che magari prendono un appuntamento, per un caffè in un bar, con un funzionario pubblico per concordare qualcosa e già quella telefonata può essere un indizio di qualche reato che si sta per compiere. E lì l'intercettazione

che non impediscano le indagini, che non le rendano più difficili. Noi temiamo che il risultato, con la vostra consapevolezza e volontà - questo per noi è molto grave - sia di spostare l'esercizio dell'azione penale a favore di una sorta di giustizia per censo, una giustizia di classe, perché i poveri cristi vanno in carcere, che per molti di voi - non voi fisicamente presenti, ma per la vostra cultura - di fatto è una sorta di discarica sociale. Oggi le carceri sovraffollate sono luoghi dove i detenuti sono trattati in maniera disumana. Si tratta di persone che hanno sbagliato e devono anche espiare una pena e pagare un debito con lo Stato. Ma le carceri devono servire a recuperare e a rieducare e una persona rieducata, che può reinserirsi nella società, non torna a delinquere. *(Applausi)*. Investire in carceri umane, nell'articolo 27 della Costituzione,

che impedisce e rende più debole il contrasto ad alcuni reati? Parliamo di reati - è stato ricordato - come l'usura, la bancarotta, gli omicidi, le stragi, la violenza sessuale, ma anche la corruzione, i reati contro la pubblica amministrazione, che vengono derubricati non solo con questo provvedimento, ma anche con gli altri provvedimenti che avete quasi un *optional* il contrasto alla corruzione. E invece la corruzione è molto spesso non solo un reato spia, ma anche l'anticamera di reati che coinvolgono la criminalità organizzata. a proposito di intercettazioni, bisognerebbe investire più risorse in tecnologia: le mafie e la criminalità già investono miliardi nelle piattaforme criptate, anche per penetrare le piattaforme dello Stato, come ci ha ricordato il procuratore nazionale Melillo in un'intervista di ieri al

questa limitazione per le intercettazioni inequivocabilmente rischia di favorire anche i criminali più scaltri, che cercheranno il momento migliore, quando sono scaduti i quarantacinque giorni, per poter esercitare il loro malaffare. La giustizia ha bisogno di ben altro e - come è stato detto, mi pare, dal senatore Scarpinato - la vostra politica della giustizia è una scelta politica, e non una scelta per far funzionare meglio una giustizia, per la ragionevole durata dei processi, ma per riaprire una guerra, con il rischio - mi auguro davvero che non sia premeditato - di fare una giustizia di classe che colpisce soltanto i più disgraziati.

occorreva per delimitare le zone inesplorate dell'Africa, ma che nel linguaggio corrente viene invece ad indicare gli sconfinamenti. Di più, viene ad ammonire il viandante sugli indebiti sconfinamenti e di indebiti sconfinamenti, in Italia, sul territorio delicatissimo della separazione dei poteri, ne abbiamo vissuti purtroppo tanti, troppi. E questi indebiti sconfinamenti sono pressoché sempre avvenuti nel terreno proprio esclusivo del legislatore. Allora, in una cornice di *cupio dissolvi* delle garanzie difensive e lungo un crinale opaco di giustizialismo cieco o talvolta politicamente orientato, è accaduto che la Repubblica abbia talvolta consentito che si facesse strame di un precetto costituzionale, quello dell'articolo 15 della Costituzione, che sancisce la inviolabilità, la libertà e la segretezza della comunicazione in ogni sua forma. È un precetto che, invocando la inviolabilità, riporta all'articolo 2 della Costituzione, cioè a quei diritti assoluti che preesistono agli ordinamenti giuridici perché riguardano le libertà fondamentali. Non vi è dubbio che il diritto tutelato dall'articolo 15 della Costituzione sia quindi un diritto assoluto, inviolabile, intrasmissibile, inalienabile, imprescrittibile, inderogabile, indisponibile. *(Applausi)*. questo specifico diritto e per garantire questo ambito di libertà, il legislatore costituente aveva già all'epoca previsto una doppia barriera, una doppia garanzia: riserva di legge e riserva di giurisdizione. In base alla prima (riserva di legge), mai limitare il diritto di comunicazione se non per atto di legge, con le rispettive garanzie, o, (riserva di giurisdizione), per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Non vi è chi non veda oggi che in tema di intercettazioni telefoniche, telematiche e informatiche, ambientali, tutto questo originario rigore sia andato perduto e come gli interventi legislativi, e di più quelli giurisprudenziali, soprattutto quelli politicamente orientati, abbiano modificato questo contesto, lo abbiano stravolto, lo abbiano mortificato. allora che oggi la disciplina delle intercettazioni sia, nella formula attuale, legata all'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, che prevede che il pubblico ministero che dispone le intercettazioni indichi modalità e durata delle operazioni. La durata delle operazioni dovrebbe essere di quindici giorni, un termine stabilito dal legislatore, che poneva già in equilibrio l'esigenza di riservatezza con la necessità investigativa, e che consentiva, ricorrendone i presupposti e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, di disporre le proroghe. nella criticità della espansione massiva di questo strumento, è accaduto che le proroghe siano divenute di fatto illimitate ed è purtroppo accaduto, nell'ambito di questa deriva, che sia venuto a mancare del tutto il controllo giurisdizionale della riserva di giurisdizione. *(Applausi)*. È inoltre accaduto, e accade sistematicamente nella prassi giudiziaria, che le autorizzazioni, soprattutto in termini di proroga, vengano disposte con formule di stile, senza alcuna autonoma motivazione da parte del giudicante che dovrebbe controllare il pubblico ministero, che dovrebbe controllare la polizia giudiziaria. altresì che si apponga la formula «visto agli atti», che mortifica il ruolo del giudice in un momento di tale invasività nella sfera privata di un soggetto e, purtroppo, la Corte di cassazione, che dovrebbe presidiare, quale massimo organo di legittimità, l'operato delle strutture giudiziarie, ha avallato questa tesi consentendo che si ricorra che si ricorra a motivazioni estremamente succinte, oppure ispirate a criteri di minore specificità. Di qui la necessità di un intervento di riequilibrio che riponga, a presidiare questa libertà, la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. Il disegno di legge si compone che si integrano e si bilanciano tra loro: uno a tutela dei diritti elementari del cittadino, anzi dell'individuo, l'altro complementare, non meno rilevante, a strenua difesa della comunità nazionale. Non vi è dubbio, infatti, che occorra preservare lo strumento investigativo. Non vi è dubbio che lo strumento delle intercettazioni debba rimanere nella disponibilità della polizia giudiziaria per perseguire i reati, non ad uso esplorativo, e che occorra presidiare un ulteriore elemento costituzionalmente protetto e garantito. Il nuovo testo che cosa fa? Stabilisce che il termine della durata ordinaria sia di quarantacinque giorni, cioè il termine originario, con due proroghe successive, ma stabilisce altresì, oltre questo tetto che, qualora ricorrano necessità investigative ulteriori assolutamente necessarie per il proseguimento delle indagini, rafforzate da espressa motivazione e determinate dall'insorgere di elementi specifici e concreti, questo possa tranquillamente essere disposto oltre il limite. Di più, perché il secondo comma, che bilancia il primo, stabilisce espressa deroga a questo regime per i reati di maggiore allarme sociale, per tutti i reati di terrorismo e per tutti i reati di criminalità organizzata in qualunque forma. È chiaro che, soprattutto per i reati di maggiore invasività, lo strumento investigativo della captazione rimane indispensabile e va anzi indirizzato e potenziato presso le due Direzioni distrettuali antimafia, perché è uno strumento eccezionale, indispensabile in quella tipologia specifica di attività giudiziaria. Quindi, tutt'altro che una rinuncia agli strumenti investigativi; al contrario, una puntuale rideterminazione ridefinizione dei confini entro i quali può essere e deve essere applicato. Una norma di mera, ordinaria civiltà giuridica. Signor Presidente, non vi è dubbio che con questo provvedimento non operiamo nessuna rinuncia, nonostante battaglie di retroguardia o culture di oscurantismo. Noi, al contrario, andiamo semplicemente a ridefinire una cornice di garanzie intorno alle intercettazioni e lo facciamo in una visione d'insieme, con provvedimenti già approvati dal Parlamento, che sono quelli che riguardano la tutela dei terzi estranei alle indagini, il divieto di intercettazioni delle comunicazioni tra avvocato e assistito, la procedura di garanzia del sequestro dei dispositivi elettronici. Nessun passo indietro. Noi non consentiamo ad alcuno di sindacare legalità, fermezza, rigore e soprattutto la cura la cura della sicurezza dei cittadini come priorità irrinunciabile. Convincetevene: Fratelli d'Italia è assolutamente questo.

colleghi, «sono grato alla progeria, non la vivo come una condanna, né tantomeno come una punizione divina, non cambierei una virgola della mia vita e so anche perché: perché ho avuto la forza di prenderla per quello che è e renderla unica». Queste parole esprimono la grandezza di Sammy Basso, un ragazzo straordinario un ragazzo straordinario che amava la vita, un esempio eccezionale di coraggio, forza e positività. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Sammy rimaneva immediatamente conquistato dal suo sorriso, dalla sua vitalità e dalla sua gioia di vivere. A me piace vivere e voglio fare più cose possibili, perché dovrei piangermi addosso? Questo era Sammy, un vero e proprio inno alla vita, una persona splendida che ha superato tutti gli ostacoli insieme ai suoi meravigliosi genitori, mamma Laura e papà Amerigo, che lo hanno amato sopra ogni cosa. Vicentino di Tezze sul Brenta, il mio paese, orgogliosamente veneto e cittadino del mondo, Sammy ha insegnato a tutti noi che la vita merita di essere vissuta fino in fondo con sorriso, entusiasmo e passione, da protagonisti e non da spettatori. Perché, come diceva spesso, non serve essere perfetti per fare qualcosa, l'importante è fare e non è mai troppo tardi per fare. Sammy di cose belle e importanti ne ha fatte tantissime, grazie alla sua intelligenza, alla sua fede in Dio e alla sua spettacolare autoironia. È stato scienziato, scrittore, *testimonial* della ricerca scientifica, conosciuto in tutto il mondo, ma la cosa più importante che durerà per sempre è lo straordinario esempio di vita, valori e amore che Sammy ha lasciato a tutti noi. Se i potenti della terra capissero cosa significa lottare per la vita - amava ripetere - credo che non avrebbero il coraggio di fare la guerra. Riposa in pace piccolo grande Sammy e grazie dal profondo del cuore perché hai insegnato a tutti noi il vero senso della nostra

l'ennesimo femminicidio avvenuto questa mattina, alle prime ore dell'alba, nella provincia di Caserta. Ancora una volta una donna uccisa per mano di un marito, un compagno di vita e, ancora una volta, di fronte ai loro figli, a due bambini di quattro Non ci sono parole rispetto a questo dramma quotidiano che stiamo vivendo nella nostra società.

in Italia dall'inizio dell'anno. Sono raddoppiati i maltrattamenti in famiglia, così come sono aumentati ancora di più le violenze e gli abusi sui minori. Se ne consumano 19 al giorno: sono numeri raccapriccianti, a cui - mi permetterete - non credo sia da aggiungere altro. altro. L'appello che rivolgo al Governo e a tutto il Parlamento è non solo quello di non abbassare la guardia, ma di continuare soprattutto a lavorare insieme per cambiare la cultura di questo Paese, per fare davvero un lavoro sui nostri figli, a cominciare dai nostri figli maschi, che abbiamo il dovere di educare al rispetto dell'altro. Lo dico da mamma di un maschio di quattordici anni. È importantissimo continuare a lavorare su questo aspetto. So, signora Presidente, quanto anche lei sia sensibile a questo argomento e quanto

continuando a far crescere il numero degli orfani di femminicidio. Signora Presidente, intervengo in merito alla vertenza Portovesme srl: sostanzialmente è un colpo di grazia che il territorio del Sulcis Iglesiente in Sardegna subisce dopo una serie di pugnalate alle spalle ricevute nella negli ultimi anni. Faccio una sintesi di cosa è successo: Glencore, datore di lavoro in questa vertenza, ha annunciato nelle scorse settimane di voler chiudere anche la produzione zinco. Parliamo di una produzione unica in Italia, di una produzione nazionale strategica. Ebbene, il 24 settembre il ministro Urso ha convocato Glencore al Ministero. C'è stato quindi un tavolo di confronto molto interessante, a cui ho avuto l'onore di partecipare. Erano presenti le rappresentanze

proponendo un'alternativa di cui si conosce veramente poco. Il Ministro ha chiesto a Glencore di illustrare il contenuto di questo progetto nelle giornate dell'8 e 9 ottobre, quindi in questi giorni. Forse questo incontro è ancora in corso. Tramite lei, Tramite lei, Presidente, chiedo al Ministro di aggiornarci prontamente sull'esito di questo incontro, anche perché la proposta avanzata da Glencore avrà sostanzialmente come oggetto il trattamento dei fumi di acciaieria, un'attività che impegnerà circa 250 lavoratori rispetto ai 1.200 attuali. attuali. Ci chiediamo innanzitutto che fine faranno gli altri mille lavoratori, ma soprattutto parliamo di una proposta che stravolgerà completamente l'assetto industriale non soltanto del Sulcis Iglesiente della Sardegna, ma addirittura nazionale. Quindi, rivolgo a lei questo appello: parliamo di 1.250 famiglie che stanno aspettando sono molto preoccupate, deluse e amareggiate, anche perché Glencore non ha mantenuto fede a una serie di promesse fatte. In nome di queste famiglie, chiedo un aggiornamento tempestivo.

La seduta è tolta